Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 747, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge

La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 44, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di organizzazione della pubblica amministrazione, di sport e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica 2025. Fondamentalmente si va a rendere più attrattivo, come da indicazione del Ministero per la pubblica amministrazione, il pubblico impiego e si cerca di far entrare persone competenti nella pubblica amministrazione. Abbiamo fatto tutto? Probabilmente no, ma tutto non si poteva fare. Continueremo? Sicuramente sì. Mi riferisco, tra l'altro, al trattamento accessorio per la valorizzazione dei lavoratori, degli enti di ricerca e dell'aumento del compenso per i vincitori di progetti di ricerca. Questo significa non far andar via dal nostro Paese i cervelli. Cerchiamo di farli restare nel nostro Paese. Penso che questo sia un passaggio di fondamentale importanza, lo è la previsione di un'intensa attività di monitoraggio sulle azioni fondamentali della pubblica amministrazione e la formazione e la valutazione delle *performance* nella pubblica amministrazione. Quanto è importante la valutazione delle *performance* rispetto a qualcosa di pubblico che pagano tutti i cittadini? Per quanto ci riguarda, è molto importante. Per quanto riguarda poi il famoso ricambio generazionale, molte volte ricordato in quest'Aula e non soltanto in quest'Aula, mi limito a due dati: sono previste 3.000 assunzioni straordinarie e saranno assicurate 2.100 assunzioni al comparto sicurezza e difesa. Questo significa avere una visione della pubblica amministrazione, significa immettere nuove risorse e forze fresche. Sarà stabilizzato il personale impiegato negli uffici speciali per la ricostruzione *post*-sisma nei crateri e ancora sono previste stabilizzazioni nelle Regioni, nelle Province, nelle Città metropolitane e nei Comuni del personale già in servizio.

questo sia, per chi governa i territori, un passaggio di fondamentale importanza. Sono tante le sfide che attendono gli uffici pubblici, che da anni ormai si confrontano con difficoltà elevate che incidono spesso sulle direttrici che presentano grosse criticità. Penso al *turnover*, al ricambio generazionale, alla ricerca delle competenze, alla formazione, altro elemento fondamentale. Si è infatti ritenuto, con questo provvedimento, di intervenire anche considerando l'attuale contesto della pubblica amministrazione. Secondo i numeri recentemente illustrati dall'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL), il personale dei Comuni si è ridotto di un terzo negli ultimi quindici anni, passando da 480.000 unità nel 2007 a 315.000 nel 2021. riduzione è frutto del blocco del *turnover* per svariati anni e questo ha portato la pubblica amministrazione ad essere fortemente indebolita e molto fragile. Si è assistito, come abbiamo detto, a un depauperamento delle risorse in termini numerici negli ultimi dieci anni. La nostra pubblica amministrazione si è impoverita di 300.000 unità, ma io mi sento di parlare anche di depauperamento qualitativo: l'età media dei dipendenti pubblici sfiora i

Da qui l'esigenza di iniziare ad intervenire con questo testo per potenziare e stabilizzare organici e portare forze fresche all'interno delle pubbliche amministrazioni. Per tutte queste ragioni, signor Presidente, annuncio il voto favorevole del mio Gruppo al provvedimento in esame.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando il Governo ha annunciato la propria volontà di emanare un decreto riguardante il rafforzamento della pubblica amministrazione, abbiamo sperato in un provvedimento che andasse a potenziare la macchina amministrativa degli enti pubblici del nostro Paese. Abbiamo immaginato un piano straordinario di stabilizzazione delle migliaia di lavoratori e lavoratrici precari che lavorano alle dipendenze della pubblica amministrazione. La riforma della pubblica amministrazione rappresenta un tema fondamentale nel processo di modernizzazione del Paese, soprattutto adesso che dobbiamo affrontare una sfida importante come quella del PNRR, che ci mette a disposizione importanti risorse. È chiaro a tutti noi che che per farlo al meglio abbiamo bisogno di più personale, di persone qualificate, di dare sicurezza e stabilità ai lavoratori e alle lavoratrici della pubblica amministrazione. Ancora una volta, questo Governo ha deluso tutte le nostre aspettative. Questo decreto-legge rappresenta secondo noi un grande fallimento perché la riforma della pubblica amministrazione, quella che ci avete prospettato in pompa magna e che ci aspettavamo, non c'è dentro questo decreto. Non c'è un disegno di rafforzamento della pubblica amministrazione al fine di dare energia a tutti quei progetti che ci possono permettere di realizzare un Paese più innovativo e sostenibile, capace di offrire ai nostri giovani le opportunità che spesso, ormai, tristemente cercano all'estero. Eppure, considerando 300.000 persone che andranno in pensione da qui al 2026, 700.000 nel 2030 - le poche assunzioni che avete scelto di fare riguardano i vertici dell'amministrazione e non la base. Certo, è importante avere vertici all'altezza della pubblica amministrazione, ma soprattutto servirebbe una massiccia immissione di nuove energie,

abbiamo cercato di dare un contributo per migliorarlo; tuttavia, nonostante lo sforzo importante fatto da noi e dalle altre opposizioni per cercare di arrivare almeno alla stabilizzazione di una parte delle migliaia di precari della pubblica amministrazione, non c'è stato alcun cenno di disponibilità da parte della maggioranza. Vorrei ricordare in quest'Aula che le persone che lavorano per la pubblica amministrazione con un contratto precario e non stabile hanno il diritto di immaginare che questo lavoro possa avere una prospettiva e un futuro per loro stessi e per le loro famiglie. inoltre, che senso abbia che lo Stato investa nella formazione di questi lavoratori e lavoratrici se poi decidiamo di rinunciare al loro apporto e li mandiamo a casa una volta formati. Che senso ha mandare a casa queste persone e farne a meno nel momento più importante della vita politica e amministrativa del nostro Paese? Questo è un errore che l'Italia non può permettersi di fare.

decidete di trasformare il presente decreto-legge in uno scontro ideologico con la Corte dei conti. È evidente, infatti, il tentativo di addebitare i vostri ritardi e le vostre incapacità nell'attuazione dei progetti del PNRR, tacciando di iperburocrazia il giusto compito di controllo concomitante della Corte dei conti; il tutto quando proprio pochi giorni fa la Struttura di missione del PNRR ci ha fatto sapere, con

vista. In sintesi, l'idea che il rallentamento sul PNRR sia dovuto al fatto che la Corte dei conti esercita un controllo concomitante, oltre a essere falsa, è pure sbagliata. Mai avremmo potuto pensare che una norma che va a toccare i poteri di un organo costituzionale così importante potesse essere presentata di notte, attraverso un emendamento al decreto-legge, quasi di nascosto per sottrarla al dibattito parlamentare.

con l'intendimento di rafforzare la pubblica amministrazione, ma poi è diventato qualcosa di diverso, un altro decreto *omnibus,* eludendo così anche il richiamo del Presidente della Repubblica, che ha chiesto di limitare la prassi della decretazione d'urgenza,

ciò che manca nel provvedimento è chiarissimo. Serviva intervenire sulla questione dei diritti e dei salari dei dipendenti pubblici, ma avete bocciato tutti gli emendamenti dell'opposizione

che da qui al 2023 mancherà un milione di lavoratori e lavoratrici. Se non interveniamo ora ci ritroveremo con una gravissima carenza di organico e rischiamo il blocco della macchina organizzativa e amministrativa di questo Paese. Rimandando le stabilizzazioni, il Governo si assume la responsabilità di non garantire un potenziamento adeguato della nostra capacità amministrativa e soprattutto spalanca la strada all'aumento delle esternalizzazioni e della privatizzazione di un numero sempre maggiore di servizi della pubblica amministrazione. Per tutti

per l'ennesima volta ci apprestiamo a convertire un decreto-legge senza che uno dei due rami del Parlamento abbia potuto esercitare le sue prerogative. Siamo ormai in un monocameralismo alternato, in cui un ramo lavora e l'altro si limita a una burocratica vidimazione. È una modalità che svilisce la democrazia parlamentare e che la svuota nella prassi. Tuttavia, questa non è l'unica forzatura sul piano del metodo. amministrazione è infatti il primo decreto-legge che arriva dopo l'incontro tra i Presidenti di Camera e Senato e il Presidente della Repubblica. Secondo quanto riportato nelle Conferenze dei Capigruppo di Camera e Senato, l'oggetto dell'incontro è stato il richiamo a non abusare della decretazione di urgenza e a vigilare affinché il vaglio di inammissibilità e improponibilità degli emendamenti, che compete ai Presidenti delle due Camere, impedisse di trasformare i decreti in decreti *omnibus*. Se il Presidente della Repubblica fa un rilievo formale in questo senso, è ancora più singolare che proprio il decreto pubblica amministrazione lo ignori così palesemente. non solo lo ignora, ma addirittura viene proposto immediatamente un secondo decreto-legge, di analogo contenuto. Certamente l'abuso della decretazione di urgenza non è un fatto nuovo, tanto da essere stato oggetto di vigorose critiche proprio da parte di Giorgia Meloni quando era all'opposizione, critiche corredate dalla promessa che avrebbe fatto meglio una volta al Governo. Oggi è al Governo, sostenuta da una maggioranza parlamentare che vanta numeri solidi, tanto alla Camera quanto al Senato, numeri che permetterebbero di votare agevolmente e celermente tutte le norme che il Governo propone, senza abusare della decretazione di urgenza, del monocameralismo di fatto e dei voti di fiducia. Una palese incoerenza, quindi, che ci porta a chiedere se la scelta della decretazione d'urgenza, corredata dal voto di fiducia, dipenda dal timore che la maggioranza non sia così coesa, oppure se si tratti di un disprezzo sostanziale del ruolo del Parlamento. Venendo al merito del decreto-legge, rispetto al quale, essendo stata posta la questione di fiducia, il Gruppo per le Autonomie esprimerà un voto contrario, è deludente anche sul piano del merito, a fronte dell'altisonante obiettivo di rafforzare la pubblica amministrazione, si limita a misure spot ed è, nei fatti, una occasione mancata. Il decreto prevede una mera e limitata serie di assunzioni e di stabilizzazioni in vari settori della pubblica amministrazione. Prevede di incrementare le dotazioni della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo più con la diretta collaborazione, evitando di rendere trasparente per quali tipi di figure e per fare cosa. Il provvedimento, scritto con l'obiettivo di accelerare l'attuazione del PNRR, avrebbe invece dovuto intervenire sul cuore organizzativo della pubblica amministrazione, attuando quei passi avanti già delineati nelle riforme avviate dai precedenti Governi. Alla pubblica amministrazione serviva un intervento davvero utile per la semplificazione amministrativa, per la digitalizzazione, l'ammodernamento organizzativo, la formazione e la valorizzazione del personale tramite percorsi di carriera e retribuzioni. Invece, il decreto è incapace di volare alto, rinunciando alla possibilità di trasformare la pubblica amministrazione e di renderla il motore per una efficace e tempestiva realizzazione del PNRR. Gli unici elementi positivi sono alcune misure a favore delle nuove generazioni, come le facoltà assunzionali di giovani laureati, individuati su base territoriale, nel limite del 10 per cento e per sei mesi con apprendistato, oppure la possibilità di stipulare convenzioni con le università per individuare studenti con meno di ventiquattro anni, che abbiano concluso gli esami, da assumere con contratti di formazione e lavoro. Tuttavia, il decreto-legge in esame resta sostanzialmente vuoto delle riforme necessarie ed è ancorato ad un contesto di pubblica amministrazione che non esiste più. È proprio con riferimento all'orientamento dei giovani verso il pubblico impiego che si delineano timide norme, sottese al pensiero debole, ritenendo ad esempio che basti migliorare la comunicazione, rendendo più accessibili le informazioni sui concorsi pubblici, o che sia sufficiente diminuire i tempi di pubblicazione dei bandi, nonché l'abrogazione di alcuni passaggi tecnici In realtà, oggi non c'è confronto e non c'è competizione tra mercato del lavoro pubblico e mercato del lavoro privato, laddove il secondo è l'unico veramente competitivo, che riesce a riconoscere completamente e compiutamente il merito, anche in termini economici. Per coinvolgere talenti nella pubblica amministrazione, servono orientamento, servizi di *placement*, rafforzamento dei servizi di selezione del personale, opportunità di crescita di carriera e stipendi che premino risultati ed impegno. I limiti di un modello orientato verso le selezioni centralizzate a livello nazionale, rispetto a quelle territoriali, si sono già visti con i *navigator* e con le figure professionali connesse al PNRR. Tali modalità di selezione hanno portato ad un altissimo numero di rinunce, alcune già in fase di prima assegnazione, molte altre solo dopo pochi mesi di lavoro. Anche sotto il profilo della attrattività e della capacità di mantenere la forza lavoro, i segnali sono fortemente contraddittori. Penso al costante ritardo dei rinnovi contrattuali, per cui è diventata la norma il fatto che si approvi il contratto collettivo nazionale di lavoro triennale quando il triennio di riferimento è già decorso, ma penso anche all'introduzione timida e tardiva di elementi di *welfare* aziendale ai continui *stop and go* sullo *smart working*, che dovrebbe invece essere implementato nel rispetto di tutte le regole del lavoro agile. Signor Presidente, per otto mesi avete parlato solo di cambio di *governance* del PNRR, raggiungendo l'unico obiettivo di rallentarne i processi. Avete parlato di rimodulazione dei *target*, senza presentare alcuna proposta in merito. Sostanzialmente si è soltanto perso tempo, ritardando il saldo della terza rata, con un nulla di fatto 27 obiettivi del secondo semestre 2023, che scadono alla fine del mese e la cui realizzazione compete interamente al Governo Meloni. Il PNRR è la più grande opportunità di crescita, di sviluppo, di risoluzione dei problemi strutturali che l'Italia abbia mai avuto e, invece, state riuscendo a trasformare una grande occasione in un problema e in uno scontro politico e di carattere istituzionale. al Governo ci siete voi: portate a casa questi progetti, altrimenti assumetevi la responsabilità davanti al Paese e alle future generazioni.

C'è da riflettere forse su un meccanismo che non funziona più, su un bicameralismo così ingessato che, di fatto, ormai è dato per scontato che un provvedimento che viene assegnato

tanto quasi da non denunciarlo più. Invece noi lo denunciamo con forza, perché era oggetto di una riforma costituzionale che è stata bocciata, anche grazie al voto contrario dell'attuale maggioranza al governo, che quindi mi aspettavo facesse esattamente l'opposto una volta andata al governo. si è tranquillamente accomodata in questo malcostume. Allora, non parliamo più nel nostro Paese di bicameralismo e diamo veramente fuoco alle polveri delle riforme costituzionali in modo serio e completo. fiducia su un provvedimento che francamente non pensavamo arrivasse così. Non pensavamo arrivasse un decreto-legge sulla pubblica amministrazione, dato che è uno dei cardini che abbiamo negoziato con l'Europa per ottenere i fondi del PNRR: una pubblica amministrazione più moderna, efficace e semplice. Forse, quindi, una simile visione non spetta a un decreto-legge, ma più a un disegno di legge, ad una delega al Governo in materia di pubblica amministrazione, anche perché quei criteri di efficienza e semplicità in questo decreto non li vediamo. quel cambio di prospettiva che probabilmente l'Europa ci chiede. La nostra macchina amministrativa è complicata ed è uno dei motivi per il quale facciamo difficoltà a rispettare i bandi di gara, i termini che l'Europa ci dà, la possibilità di spendere le risorse europee. Oggi c'è un tema che voi come maggioranza ponete sul tavolo delle riforme, quello dell'autonomia differenziata, ma siete consapevoli di quanta fatica facciano gli enti locali nel rispettare i termini dei bandi del PNRR? *(Applausi)*. I piccoli Comuni non ce la fanno, non solo per mancanza di numero di tecnici che affrontano i *dossier*, ma perché i *dossier* sono troppo complicati per i nostri piccoli Comuni. Sono complicati per le città metropolitane come Roma, Milano e Torino, figuriamoci per i piccoli Comuni. E voi volete accentrare ancora di più le competenze a livello locale, quando ci aspettavamo, per esempio, che in questo decreto-legge si ponesse l'accento sulla formazione della nuova classe dirigente. Ha ragione il collega Patton che mi ha preceduto: la pubblica amministrazione che voi disegnate in questo decreto è vecchia, non è più attuale, perché oggi c'è maggiore digitalizzazione, perché oggi ci chiedono e si richiedono nuove competenze. Eppure, la formazione di chi va a rivestire il pubblico impiego è esattamente uguale a quella degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta basta, come se fossero l'unico modo per selezionare una classe dirigente competente a dare risposte al Paese. Non ci stupiamo poi che ci vogliano sei mesi per fare la carta d'identità, perché evidentemente tra una pubblica amministrazione che va ancora a timbri e quella che dovrebbe andare con l'intelligenza artificiale tutto si blocca completamente. *(Applausi)*. Io speravo che si vedesse una strada verso quella che in Francia ormai c'è da secoli, con l'*école publique* la formazione del pubblico dirigente, perché la soluzione non è solo nell'aumentare le risorse, ma nel formare veramente. Oggi, nei nostri Ministeri si fa fatica a dare risposta alle domande poste dal PNRR. Noi presentiamo emendamenti e ascoltiamo spesso pareri che - spero mi perdonerà chi mi sta ascoltando - non sono completamente corretti, perché oggi c'è una classe di amministratori pubblici e persone che lavorano nel pubblico impiego anziana, che si è formata secoli fa, che ha una grandissima esperienza sul campo, ma che spesso è lontana dalle nuove regole e ragiona ancora come come quando è entrata a far parte della pubblica amministrazione. Parlo di un Ministero su tutti: il Ministero che fu della transizione ecologica e adesso è dell'ambiente e della

crea una narrazione giusta e positiva di un nuovo tipo di economia. Queste due narrazioni non vanno d'accordo e lo si vede nei pareri dati sugli emendamenti, che dovrebbero andare verso la produzione economica, da una parte, mentre continuiamo a ricevere pareri negativi sulla tutela e sulla "incontaminazione" dell'ambiente, come se nulla fosse scritto nel PNRR in merito alla transizione ecologica. Questo decreto, allora, non è per la pubblica amministrazione; è un decreto che stabilizza una parte dei lavoratori, che dà un piccolo sollievo, non tutto, alle amministrazioni che sono rimaste indietro nel tempo a livello di personale qualificato, ma tutto qui. C'è da dire che, in tema di ritardi del PNRR, uno dei maggiori riguarda proprio la riforma della pubblica amministrazione che dall'Europa si aspettano.

Noi vi abbiamo detto che c'era una parte che riguardava la Corte dei conti già prevista dai Governi Conte e Draghi. Vi abbiamo detto,

per noi era invece un elemento che poteva aiutare la pubblica amministrazione, perché poi è il funzionario che deve firmare e deve essere sicuro

questo decreto "decreto fallimento", perché con esso avreste dovuto potenziare la pubblica amministrazione, mentre avete certificato il vostro fallimento nella gestione del PNRR:

La Corte dei conti ha certificato che dei 32 miliardi del PNRR che bisogna spendere nel 2023 avete speso poco più di un miliardo. Voi cosa avete fatto? Con un *blitz* notturno - come fate spesso - in Commissione alla Camera avete deciso di abolire il controllo concomitante, che è previsto proprio per valutare l'efficienza e l'efficacia dell'uso delle risorse finanziarie. Ma sapete qual è la cosa più surreale? È che negli archivi del Senato c'è ancora il vostro disegno di legge, a firma Fazzolari, un vostro Sottosegretario, che chiedeva di potenziare questo stesso controllo concomitante che oggi state abolendo. questa cancellazione serve per mascherare il fallimento nella gestione del più grande piano di investimenti pubblici che l'Italia abbia mai avuto a disposizione. La dinamica è sempre la stessa: voi non riuscite a fare le cose, voi fallite e la colpa è di qualcun altro. Oggi la colpa è della Corte dei conti; ieri era del presidente Conte e del MoVimento 5 Stelle, che hanno fatto arrivare troppi soldi in Italia. In legge di bilancio, la colpa dell'aumento dei prezzi dei carburanti era dei benzinai e non del fatto che voi non avete rinnovato lo sconto sulle accise. decreto-legge bollette, la colpa era dell'autorità di regolazione per l'energia, quando invece non avete riproposto gli aiuti per le famiglie e per le imprese. Questo vostro fallimento lo si legge anche dai dati macroeconomici, dal quadro più ampio nel quale

l'avete letto, quel documento Istat? Perché non c'è nulla di trionfalistico; anzi, le prospettive economiche per il 2023 2024 sono molto preoccupanti e forse il ministro Giorgetti se n'è accorto, visto che in una nota ieri ha parlato di crescita come un miraggio, quindi si rende conto che in questo momento non possiamo parlare di crescita. Il rapporto Istat dice proprio questo, perché

Il dato più preoccupante di quel rapporto Istat è il crollo della produzione industriale: -7,2 per cento nella produzione industriale ad aprile, che per un Paese manifatturiero come l'Italia è un dato gravissimo. Ma neppure ve ne accorgete. Il rallentamento della crescita è innescato anche dal ridimensionamento delle agevolazioni edilizie, soprattutto del superbonus.

per supportare i cittadini che non riescono più a pagare le rate dei mutui. Quindi, se sapeste leggere quel rapporto Istat, capireste che esso evidenzia che senza il PNRR

A proposito di edilizia, vi chiedo anche di leggere la ricerca che è stata pubblicata, tra gli altri, proprio dal consigliere economico del ministro Giorgetti, secondo cui il superbonus ha avuto un effetto positivo sulla crescita del PIL, sugli investimenti e sulla riduzione del debito pubblico, perché nell'ultimo biennio il rapporto debito-PIL si è ridotto di 11 punti. Questo Questo perché abbiamo capito, a differenza vostra, che se siamo in pericolo di recessione bisogna investire sulla crescita e non tagliare le spese. Voi invece avete scelto l'austerità e avete tagliato i servizi ai cittadini. Avete tagliato *in primis* alla sanità: infatti, in base al vostro DEF, nel 2025 investiremo in sanità il 6,2 del PIL, meno di quello che si investiva prima della pandemia. Ma non avevamo detto che bisognava raggiungere l'8 per cento del PIL? Ma non li leggete gli appelli del presidente dell'Ordine

altro che emergenze inventate. *(Applausi)*. Mettiamo un commissario per le liste d'attesa in sanità e investiamo per assumere personale sanitario. L'allarme lanciato ieri dal presidente dell'Ordine dei medici è che, a breve, altri 10.000 medici lasceranno la sanità pubblica per andare a lavorare nel privato, perché non state facendo altro che gonfiare sempre di più la sanità privata. Evidentemente questo è il vostro disegno: indebolire il servizio sanitario pubblico e incrementare le risorse per il servizio sanitario privato, in modo che chi può pagare mentre chi non può pagare deve aspettare mesi in lista d'attesa e, quando finalmente farà quella visita, probabilmente non avrà più modo di essere curato. Di questo voi siete responsabili. Avete tagliato in sanità, avete tagliato tutti gli investimenti in edilizia e in innovazione tecnologica, avete bloccato la cessione dei crediti, quando gli Stati Uniti hanno appena approvato un maxi-piano di investimenti in transizione ecologica basato tutto sulla cessione dei crediti. Questo, oltre ad essere il decreto fallimento nella gestione del PNRR, è il decreto intolleranza verso tutti gli organi di controllo e le autorità di controllo che garantiscono la trasparenza. Questa è la volta della Corte dei conti; in precedenza vi siete scagliati contro Bankitalia, quando ha espresso dubbi sulle coperture per la legge di bilancio, contro l'ANAC, quando ha manifestato perplessità sul nuovo codice degli appalti, e addirittura contro il Servizio studi e il Servizio del bilancio del Senato, che hanno detto di fare attenzione al profilo economico del progetto di autonomia differenziata. Quando vi abbiamo chiesto un'indagine conoscitiva per presentare i numeri di quel progetto ai cittadini (e non solo al Parlamento), ci avete negato anche questo. Questo è anche il decreto della solita bulimia di poltrone e di potere che avete, perché gran parte delle risorse saranno impiegate per assumere nuovo personale nei Ministeri. Ma io vi chiedo, anche qui: perché volete potenziare ancora di più i Ministeri, se con l'autonomia differenziata gli state togliendo potere? Concentrate le risorse sui territori, sulle amministrazioni locali e solo su quello. Avete anche abolito una legge che avevamo fatto nel 2019 per la la programmazione del fabbisogno di medici specialisti; avete trasformato quella struttura, che era importantissima per programmare gli specialisti che servono in base al fabbisogno di salute, in una direzione del Ministero. Avete commissariato ISMEA e CREA, che sono due enti di supporto importanti per gli agricoltori. Oggi il nostro voto sarà convintamente contrario, perché siamo contrari alla vostra mancanza di visione, alla vostra politica dei bavagli, ai vostri reati creati *ad hoc* per intimorire i cittadini *(Applausi)*, alla vostra politica di spartizione del potere. Però i cittadini se ne accorgendo, perché - come diceva Lincoln - non si possono ingannare tutti per sempre. Se ne stanno accorgendo, perché ci sono i ragazzi nelle tende fuori dalle università, perché ci sono gli ecoattivisti che vi dicono di invertire la vostra strategia climatica, perché - le chiedo solo un minuto, Presidente, e concludo - ci sono manifestazioni in tutta Italia a sostegno della sanità pubblica, perché sabato con noi in piazza c'erano 20.000 persone a chiedere di mettere fine al precariato. E anche quella piazza avete provato a strumentalizzarla, utilizzando parole che erano sulla cittadinanza Proprio voi, che invece parlate convintamente di tasse come pizzo di Stato, di sostituzione etnica, di metadone di Stato riferendovi al sostegno ai deboli. Proprio voi che avete creato il vostro consenso sulla rabbia e sull'odio sociale, alimentando quella distanza, oggi quasi incolmabile, tra istituzioni e cittadini. Voi siete questo. Noi invece siamo quelli che hanno sempre lavorato per il bene comune, che hanno portato il Paese fuori dalla pandemia mettendo assieme tutte le energie positive. Noi vogliamo che i cittadini diventino attori del cambiamento che vogliono vedere. Noi siamo questo e per questo noi votiamo contro con questo decreto

in base a quello a cui pensa e che ritiene pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione infatti è tutto, è qualsiasi cosa, dal livello centrale a quello più periferico, dai servizi più basilari per i cittadini alle cerimonie pubbliche. Tutto è pubblica amministrazione, dalla cosa più fondamentale per la vita quotidiana a quella che magari è distante anni luce dalla vita quotidiana dei nostri cittadini; reazioni positive o molto negative in base alla percezione che ognuno ha dei servizi che ha ricevuto dalla pubblica amministrazione e di quale amministrazione si tratti. Questo provvedimento che è molto eterogeneo e che parla di diverse pubbliche amministrazioni, che quindi che si rivolgono anche a fasce diverse della nostra popolazione e per servizi completamente diversi, ha un obiettivo fondamentale, anche se ovviamente non può risolvere tutti i problemi che sono stati creati soprattutto nell'ultimo decennio abbondante,

Se ci pensiamo, abbiamo vissuto degli anni in cui c'è stata una denigrazione sia della figura del dipendente pubblico sia della figura del politico, inteso come persona che si approfitta dei soldi dello Stato. Ne abbiamo sentite di ogni e non mi sembra il caso di ripetere quello che è stato detto in tanti anni. L'antipolitica e la cattiva immagine della pubblica amministrazione, che ci sono state in certi periodi della nostra storia recente, hanno fatto sì che ci sia stato un allontanamento da parte dei cittadini da entrambe le parti, e quindi nei confronti della politica e nei confronti

Adesso ne subiamo le conseguenze nel momento in cui invece ci serve una pubblica amministrazione, sia centrale che soprattutto periferica, che funzioni bene e dia risposte veloci, anche e soprattutto dopo il periodo pandemico e con il PNRR in corso. Non vi farò un riassunto Non vi farò un riassunto di tutto quello che c'è nel provvedimento perché si tratta di misure completamente diverse le une dalle altre e appare difficile fare un discorso omogeneo. Ci sono però dei punti importanti che secondo me sono da ricordare. per esempio, con un emendamento passato alla Camera, previsto la possibilità di trattenere in servizio il personale dirigenziale in possesso di specifiche professionalità. E ciò è fondamentale soprattutto in questo momento storico, nel quale bisogna avere persone preparate che riescano a gestire la fase del PNRR. Una cosa importantissima di cui si parla poco è la possibilità

individuare studenti di età fino ai ventiquattro anni che abbiano concluso gli esami da assumere con contratti di formazione e di lavoro. Il pubblico si avvicina così al mondo dell'università, si avvicina ai giovani. Non dimentichiamo che l'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione dobbiamo assolutamente invertire la tendenza e fare in modo che sempre più giovani vogliano entrare in una pubblica amministrazione che abbia un modo di lavorare più agevole e più veloce e che lavori anche bene con il mondo privato, perché il connubio pubblico-privato è fondamentale.

della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e anche delle assunzioni straordinarie per i Vigili del fuoco, con un'attenzione particolare per le Capitanerie di porto e la Guardia costiera.

garantire maggiore sicurezza nelle nostre amministrazioni. Mi auguro sinceramente, da sindaco di un piccolo Comune, che questa possibilità venga allargata anche ai Comuni più piccoli, per la sicurezza soprattutto dei nostri agenti di polizia che evitano di impugnare un'arma quando non sono assolutamente nella condizione di emergenza che li obbliga a farlo. Abbiamo previsto anche l'inserimento della carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria con dei concorsi per il reclutamento del personale per il Dipartimento per le disabilità. Ci sono quindi interventi che toccano tanti aspetti e tanti

da quota 100. I piccoli Comuni, che sono il fiore all'occhiello delle nostre pubbliche amministrazioni, sono gli enti percepiti come più vicini al cittadino, per cui i sindaci, gli amministratori, ma anche i dipendenti e i segretari comunali vivono

più risorse per le assunzioni a tempo determinato grazie al PNRR e, dove non fosse stato possibile utilizzare tali risorse in particolare per gli uffici tecnici, resta la possibilità di utilizzare per i Comuni dette somme non spese nel 2022 anche per l'anno

in questo momento sono sempre carenti. Si sta quindi facendo tanto: con questo decreto diamo la possibilità di prorogare anche il tempo di servizio dei vicesegretari comunali, ma è un problema ancora da risolvere con qualche piccolo aiuto anche a livello economico. Ovviamente non entro nel merito di tutti i provvedimenti. Dico semplicemente che come politici abbiamo una grossa responsabilità, perché il danno all'immagine della pubblica amministrazione è stato fatto anche dalla politica.

ognuno si occupa del settore di cui ha più competenza e lavora nelle proprie Commissioni o sul territorio. È importante rivalutare il ruolo della pubblica amministrazione, perché nel momento del bisogno

per le amministrazioni locali e centrali da utilizzare: facciamolo bene, facciamo sempre l'interesse dei nostri cittadini e dei nostri territori. Esprimo quindi il voto favorevole a nome del Gruppo Lega Salvini Premier-Partito

La prima e più grande ragione è che il decreto-legge muoveva dall'intenzione di fare qualcosa di concreto per rafforzare la pubblica amministrazione nel nostro Paese.

con soddisfazione - una soluzione organica dei maggiori problemi che la pubblica amministrazione italiana ha di fronte, ma nemmeno un inizio serio di soluzione. Sarebbe già stato abbastanza e invece non se ne scorge traccia. Il provvedimento appare costituito da una serie di scelte di corto respiro e frammentarie, quando invece sarebbero state necessarie scelte lungimiranti, strutturali e corrispondenti a una strategia

sono nati ieri, ma sono di antica data e sappiamo che i principali hanno a che vedere con una carenza di organico che nel corso degli anni si è fatta molto pesante; un'età media dei dipendenti della pubblica amministrazione troppo elevata; una quantità elevata; una quantità di precari tra le più alte a livello europeo. Io non darò dati da questo punto di vista, perché lo hanno già fatto molto bene ieri per il nostro Gruppo le senatrici Zambito e Furlan, che sono intervenute sul provvedimento. Infine, abbiamo un problema serio di ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro: una situazione che genera incertezza e demotivazione e non mette la nostra macchina pubblica nelle condizioni di svolgere compito nella maniera più efficiente possibile. Ciò, inoltre, non soltanto impedisce alla pubblica amministrazione di affrontare bene gli impegni ordinari - già non sono pochi

Per favorire una buona attuazione del PNRR, cioè per far sì di spendere tutto in tempo e bene, una delle misure necessarie era il varo di un piano straordinario di assunzioni nella pubblica amministrazione; un piano che tenesse conto delle differenze esistenti nel nostro Paese, tra territorio e territorio, tra comparto e comparto. Non si è visto nulla di tutto questo in questo provvedimento, né - mi spiace dirlo - vi sono segnali che vedremo qualcosa del genere in provvedimenti che stanno per arrivare o che sono in fase di concepimento. Una delle cose che io credo debba essere detta in un intervento in dichiarazione finale sul decreto in esame è anche il fatto che in questo Paese, soprattutto nelle ultime settimane, si parla molto di riforme istituzionali. penso che due riforme istituzionali siano tra le maggiori e più necessarie nel nostro Paese. Una è il rafforzamento strutturale della pubblica amministrazione, cioè della capacità dello Stato di spendere bene, di progettare bene, di corrispondere alle esigenze dei cittadini. vediamo che, da questo punto di vista, il Governo fallisce completamente la prova: inanella insuccessi e passi falsi e non riesce a fare niente di concreto. L'altra grande riforma istituzionale della quale avremmo bisogno è quella di ridurre il patologico ricorso alla decretazione d'urgenza per fare legislazione. Io avevo sentito, dai rappresentanti di questo Governo, delle rassicurazioni alle quali ho cercato di credere all'inizio della vita del nuovo Esecutivo. Ci era stato detto più o meno quanto segue: siamo il primo Governo che nasce da una indicazione chiara degli elettori da molti anni a questa parte; anche grazie alle divisioni dei nostri avversari, con poco meno del 45 per cento dei voti abbiamo preso il 60 per cento dei seggi; abbiamo una comoda e larga maggioranza nei due rami del Parlamento; potremo rispettare di più le prerogative del Parlamento, ricorrere meno alla decretazione d'urgenza, ricorrere meno ai voti di fiducia, instaurare finalmente un rapporto più corretto tra Parlamento e potere esecutivo.

più naturale e più spiegabile. *(Applausi)*. Il mio appello è il seguente. Dato che si discute di riforme istituzionali, volete, per favore, dirci quale idea avete per risolvere il problema? volete dirci se lo ritenete un problema? Noi, infatti, non siamo impauriti da una discussione su come si rende più razionale la forma di Governo in Italia. Io, perlomeno, non ho questo timore. però, di poter fare una discussione su come si rende più forte la forma di Governo nel nostro Paese senza discutere di come si ripristina un minimo di dignità del Parlamento nell'esercizio dei suoi poteri legislativi e di controllo è una provocazione. Quale proposta avanza il Governo per ridurre, per esempio, il ricorso alla decretazione d'urgenza? C'è un'idea? C'è un briciolo di idea? Noi non vediamo niente di tutto questo. Aspettiamo fiduciosi, ma con una fiducia decrescente. questo provvedimento merita una forte critica, perché contiene il famoso, anzi famigerato, emendamento che abolisce il controllo concomitante della Corte dei conti per quanto riguarda l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Io non mi soffermerò tanto sul merito tecnico dell'emendamento, perché è già stato detto molto alla Camera. Del resto, questo provvedimento è arrivato qui in Commissione a quattro giorni dai due mesi dalla sua pubblicazione. Non si possono fare molti approfondimenti. Si può però dire che, anche alla luce delle discussioni sulle ultime pseudo-riforme della giustizia, che nelle ultime ore ci stanno impegnando e dividendo, l'emendamento sulla Corte dei conti è rivelatore. Esso rivela due tendenze specifiche, peculiari della maggioranza di Governo e dell'Esecutivo. La prima il tentativo di individuare dei capri espiatori sui quali gettare la colpa dei propri *flop*. C'è un *flop*? Invece di assumersene la responsabilità e di migliorarsi, si cerca qualcuno, possibilmente un'autorità di controllo, su cui scaricare la responsabilità dell'insuccesso che si sta registrando. Questo è vero per la giustizia ed è vero per la Corte dei conti.

l'abbiamo visto con le dichiarazioni sull'ANAC. Credo di poter dire sinceramente che in Italia non c'è bisogno di meno controlli, ma c'è bisogno di meno confusione, di idee più chiare e di maggiore concretezza. C'è bisogno di ricorrere meno a una costruzione continua di propaganda per gettare fumo negli occhi dei cittadini, senza che, dopo tutto questo getto di fumo, resti nelle mani delle famiglie e delle imprese qualcosa di concreto. Infine, dato che bisogna essere conseguenti quando si chiede il potenziamento della pubblica amministrazione, credo si debba dire con forza che potenziare la pubblica amministrazione costa, che servono risorse e senza una politica di sviluppo le risorse non ci sono.

il fronte del recupero dell'evasione fiscale e del potenziamento delle entrate. Da questo punto di vista state facendo, in termini ideologici, dei danni pazzeschi Ne cito soltanto tre: il primo danno è nella legge di bilancio, con i condoni e le sanatorie, ed è la cosa peggiore che si possa fare in termini di danno alla lotta contro l'evasione fiscale. secondo esempio è la dichiarazione in campagna elettorale sul recupero dell'evasione fiscale come pizzo di Stato *(Applausi)*. È indicibile la conseguenza negativa

non pago dei danni fatti con le misure sulla giustizia, che ci metteranno in scontro con l'Europa e paralizzeranno probabilmente l'attività parlamentare per mesi, ci ha fornito la sua idea di come si debba affrontare l'evasione fiscale nel nostro Paese, e cioè non con seri processi contro chi disonestamente ruba risorse a chi paga le tasse, ma con la giustizia conciliativa. Cioè, l'idea geniale è che, verso chi non paga le tasse e non fa il suo dovere, non si deve condurre un'azione di repressione, ma ci si deve mettere d'accordo e si deve venire a patti con la disonestà. Fermatevi, perché questa cosa è dannosa moralmente ed economicamente; farà venir meno tante entrate e, se vengono meno tante entrate, avremo tutti meno risorse per modernizzare il Paese in generale, e anche per modernizzare e potenziare, in particolare, la pubblica amministrazione.

che coinvolge - come dicevo - comparti strategici. Pensiamo al tema della sicurezza urbana: questo è uno dei tanti impegni programmatici su cui stiamo dando quelle risposte per le quali ci eravamo impegnati. Ci sono 2.100 assunzioni nel comparto delle Forze dell'ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Guardia costiera); vi è l'introduzione della carriera di medico nella Polizia penitenziaria, intervenendo su un settore estremamente delicato, sul quale credo che tutti dovremmo impegnarci per un miglioramento e un rafforzamento delle condizioni generali e dell'equilibrio all'interno delle carceri, dando alla Polizia penitenziaria degli strumenti fondamentali, come appunto accade con questo decreto.

fattore secondario, ma è un elemento centrale di tutela dei soggetti deboli, delle persone che meritano di sentirsi sicure all'interno delle loro città e della loro comunità. Viene resa possibile anche l'assunzione dei segretari comunali nei piccoli Comuni: questo è un altro dei temi e delle battaglie su cui ci eravamo impegnati. impegnati. Ovviamente farò solo degli esempi, perché sono davvero tantissimi i settori su cui si interviene: penso al tema dello sport. Viene rafforzato "Sport e salute", dandogli nuove competenze sulla ricerca dei fondi sociali europei, sul lavoro e sugli altri fondi comunitari e naturalmente sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Vi sono importanti interventi sulla pubblica istruzione e sulla mobilità degli organici, che sono stati compiutamente e ampiamente illustrati dai colleghi Melchiorre e Bucalo nella discussione generale: anche questo è un tema fondamentale e strategico. Vi sono nuove funzioni - penso ad esempio a Formez - per assistere i Comuni; abbiamo spesso parlato di come l'Italia profonda, l'Italia delle municipalità, l'Italia delle piazze, dell'Italia dei campanili, l'Italia dei Comuni abbia bisogno di un sostegno reale e il decreto mette in campo strumenti da questo punto di vista. vi è il tema del turismo, la trasformazione di Enit in società per azioni, per attrarre nuovi investimenti, per svolgere un'azione costante di promozione della bellezza italiana, perché sul tema del turismo non c'è nessuno che ci possa fare concorrenza. Sono mancati però negli anni gli strumenti e, quindi, la trasformazione di Enit in società per azioni risponde a questa esigenza, così come la creazione dell'Osservatorio nazionale sul turismo. Poi vi sono fondi - qualcuno la lotta contro i tumori. Almeno su questo tema sono convinto che siamo tutti uniti e che tutte le forze politiche debbano impegnarsi insieme per contrastare una piaga che porta sofferenza in tante famiglie italiane. Nonostante questi e tanti altri interventi, che per brevità non vado a illustrare, in questi giorni la polemica e l'attenzione mediatica sul provvedimento è stata focalizzata sostanzialmente e quasi unicamente su un emendamento del Governo che - lo dico subito - noi sottoscriviamo e condividiamo.

Chiediamo loro dove erano quando i Governi da loro sostenuti affossavano la pubblica amministrazione con il blocco del *turnover* e delle assunzioni, paralizzando la pubblica amministrazione.

per gli amministratori e, quindi, l'esclusione del danno per colpa grave: nello specifico, viene mantenuto il riferimento alla colpa grave con azione omissiva, ma di fatto viene escluso questo tipo di responsabilità per la gestione pubblica di pubbliche risorse. Si tratta sostanzialmente di un'iniziativa sacrosanta - viene prorogata, ricordiamolo, e non introdotta - per ridurre il fenomeno della cosiddetta burocrazia difensiva, meglio noto come la paura della firma. Insomma, per una volta che avevate fatto una cosa giusta e noi l'abbiamo prorogata, avete trovato modo di criticare e dare la colpa al Governo anche per questo. *(Applausi)*. Naturalmente poi c'è il grande scandalo, anche qui richiamato, dell'esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti per quanto riguarda in questo caso specificamente il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ovviamente un tale tipo di intervento non interferisce minimamente con le previsioni dell'articolo 100 della Costituzione, perché rimane assolutamente intatto il controllo di gestione da parte della Corte dei conti; rimane assolutamente intatta la relazione semestrale Grazie a tutti per dieci anni sostanzialmente mai utilizzato visto che, con grande onestà intellettuale, audito alla Camera, lo stesso Presidente della Corte dei conti ha dichiarato che per tanti anni la Corte ha preferito concentrarsi sul più importante e fondamentale controllo di gestione.

sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ci sarebbe molto da dire al riguardo - esercitato nel momento in cui dobbiamo tutti correre per realizzare un obiettivo, che di fatto

il suo controllo e le sue funzioni, ma rinuncerà a uno strumento che - come ho già detto - per tanti anni non è stato utilizzato. Sul Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sarebbe molto da dire: anche chi come il sottoscritto è stato nelle amministrazioni comunali - nel mio caso di Roma -ha visto la fantasiosità di molti progetti messi in campo. Tuttavia, nonostante questo,

per portarlo a compimento e - come detto - riusciranno a farlo. In ogni caso, l'Italia non è di certo in questo momento la retroguardia sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, ma è uno degli Stati dell'Unione europea che lo sta portando avanti con maggiore determinazione. Colleghi, con questo provvedimento segniamo un passo importante verso quel patto che riteniamo strategico e fondamentale tra settore privato e e settore pubblico; per quanto riguarda il settore privato, nelle prossime ore quest'Aula esaminerà un provvedimento molto importante e direi rivoluzionario. Noi vogliamo liberare le energie dei settori produttivi italiani, dell'impresa, delle professioni. Allo stesso tempo, però, vogliamo anche restituire autorevolezza e senso di appartenenza a tutta la pubblica amministrazione: per quest'ultima è finita l'epoca della demotivazione e dell'indebolimento ed è iniziata quella del merito, con l'immissione di forze fresche, di nuove motivazioni e nuove professionalità, anche per essere all'altezza delle sfide del digitale e della modernità e per essere al fianco dei cittadini e non contro gli stessi. Questo è il nostro modello di pubblica amministrazione. Questo è lo stretto legame che mettiamo in campo con i provvedimenti che stiamo portando avanti tra settore privato e settore pubblico. Non si torna indietro: con buona pace di chi rema contro, l'Italia ha ricominciato a correre, come rilevano tutti gli indicatori economico-sociali. Con il provvedimento in esame poniamo importanti basi affinché la pubblica amministrazione sia pienamente coinvolta e attivamente partecipe

di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

chiamato dal senatore Segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza. I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Estraggo ora a sorte

chiusa la votazione. Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 747, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Allegato B).* Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge

Grazie

stato deputato e senatore e, come ricorderete, ha ricoperto per quattro volte la carica di Presidente del Consiglio. Berlusconi non c'è più o forse in qualche modo c'è più di prima. Mettiamo per un attimo nell'angolo odiatori impenitenti anche nel giorno del dolore e facciamo emergere invece il giudizio sulla unicità dell'uomo. Scorrono come in un film le immagini del giovane Silvio che si fa largo nell'Italia degli anni Ottanta, che sogna in grande, che costruisce città avveniristiche che chiama come la sua amata Milano aggiungendovi solo dei numeri (Milano 2, Milano 3), come omaggio a quella Milano che gli resterà sempre nel cuore. Poi, sempre con lo stesso spirito innovatore che lo ha contraddistinto, coglie al volo la nuova possibilità di entrare nel mondo della telecomunicazione e decide di fare concorrenza alla TV di Stato. Non è l'unico a fare questo tentativo, ma è l'unico a capire immediatamente che per fare concorrenza alla TV pubblica occorre avere lo stesso numero di reti che ha la Rai, e realizza questo suo obiettivo anche in questo campo. Nel contempo stringe con i suoi

o quasi tutti - che hanno lavorato con lui a non considerarlo un datore di lavoro, ma qualcosa di molto diverso. volendo innovare e dare il segno del cambiamento che lui imprime, entra in un campo che unisce differenze di classi, di provenienza, di Regioni: il calcio. Anche lì non con mia sempre uguale soddisfazione - ottiene successi di rilevanza mondiale. E tutto procede, innovazione e successo a titolo personale, senza veri contraccolpi, fino a quando - per usare le sue parole - decide di scendere in campo in politica. E sarei poco obiettivo se non ricordassi che a quel punto, accanto ai grandi successi e ai grandi cambiamenti che imprime alla politica (anche lì c'è un prima e un dopo Berlusconi, si impone una sorta di bipolarismo per coalizioni, cambia il rapporto tra elettori ed eletti e soprattutto diventa significativo, per non dire essenziale, il ruolo delle *leadership* e dei *leader* dei singoli partiti), partiti), si crea un problema che egli denunzia come persecuzione e che è un problema non solo giudiziario, ma anche mediatico (a suo avviso), che durerà parecchi anni. Devo però dire che, in questa che lui definisce come persecuzione, non si è mai sottolineato il fatto che Berlusconi un giudice a Berlino lo troverà sempre, se è vero, come è vero, che tutte le accuse più gravi (tranne una, l'unica per cui è stato condannato) cadranno nel nulla. Quello che invece rimane, per esempio, è il suo ruolo in politica internazionale. Quello che avvenne a Pratica di mare rimane un *unicum*: la speranza che gli Stati Uniti e la Russia potessero costruire un futuro di pace insieme porta il nome di Pratica di mare e la regia di Silvio Berlusconi. Nel bene e nel male,

Per quanto egli subisca molti contraccolpi, si può affermare che viene più volte colpito, ma mai affondato.

in ogni modo) e chi ne ha apprezzato, come me, gli enormi pregi, senza però mai fare sconti alle posizioni che risultavano diverse dalle mie convinzioni, ne conserva un ricordo in cui le luci sovrastano di gran lunga le ombre e lasciano solo il posto alla gratitudine per quanto ha fatto e al rimpianto per non averlo accanto in un momento in cui l'Italia, a mio avviso, avrebbe ancora bisogno dei suoi consigli e del suo sorriso ammaliante. Mi consola il generale rispetto - con veramente poche e non lodevoli eccezioni che ha accompagnato la sua dipartita, anche da chi non ha condiviso e non condivide le sue posizioni politiche, che fa onore a chi legittimamente lo ha contrastato in vita, ma si unisce ora a me e a tutti voi nelle sentite condoglianze che rivolgiamo a tutti i familiari, ai tanti che gli sono stati vicino, ai figli, alle persone che lo hanno accompagnato in questi ultimi anni o in tutta la sua vita affettuosamente. Ad essi rivolgiamo le condoglianze più sentite, pregandovi di osservare qualche secondo di silenzio in sua memoria.

Signor Presidente, signori senatori, Berlusconi è stato un grande innovatore

di club (anche io non ho gioito, come il presidente La Russa). È stato un grande uomo di sport e un grande innovatore in politica. Da questi banchi però io voglio ricordare Berlusconi uomo di Governo e uomo di Stato. Uomo di Stato perché ha sempre avuto dell'Istituzione un'immagine di servizio; lo Stato al servizio dei cittadini per dare loro risposte concrete. È quello che ha cercato di fare come uomo di Governo. È stato il Presidente del Consiglio che più di ogni altro nella storia della Repubblica è stato fra questi banchi.

deboli. Anche il più debole per lui era importante come il potente del mondo. Ricordo, appena insediatosi a Palazzo Chigi nel 1994, scendere contro l'opinione generale in mezzo ai minatori del Sulcis-Iglesiente che manifestavano davanti Palazzo Chigi, chiedendo interventi per il settore minerario. Lui andò lì, parlò con loro e si confrontò con loro, cercando poi di dare risposte concrete e così fu in uno dei primi Consigli dei ministri successivi a quella manifestazione. E ricordo un lungo giro a Bari vecchia, qualche anno dopo, dove incontrando

al Consiglio dei ministri successivo decise di proporre l'aumento delle pensioni minime fino a un milione di lire al mese. Di fronte a un'Italia

anche lì lo Stato e il Governo a sostegno di 4 milioni di piccole e medie imprese italiane che danno lavoro a milioni e milioni di nostri concittadini. finalizzato, anche all'azione per ridurre la pressione fiscale, alle grandi opere, all'alta velocità, all'idea di realizzare il Ponte sullo Stretto di Messina, che questo Governo sta realizzando, alla crescita

coloro che intendono uscire da una dipendenza. Lo ha fatto in silenzio e con grande discrezione, utilizzando sempre la fondazione che aveva costituito nel nome del del padre. Un'azione di Governo che ha portato il nostro Paese ad avere una presenza più autorevole, come ricordava il presidente La Russa, sul palcoscenico internazionale. Grazie a quella credibilità siamo riusciti in quegli anni a siglare accordi con i Paesi dai quali provenivano i flussi migratori e l'immigrazione si arrestò.

tanti Paesi del mondo. Le ambasciate erano strumento fondamentale per sostenere il saper fare italiano, per sostenere le nostre imprese nel mondo. Così come guardò

italiani. Tante cose, delle quali forse non si parla abbastanza, hanno caratterizzato la sua azione di Governo: pensiamo all'abolizione della tassa di successione. Ricordava sempre il lavoro e la fatica di ogni italiano che risparmia e investe per lasciare una casa ai propri figli e visto che le tasse le ha pagate per tutta la vita non era giusto che si pagasse una tassa anche nel momento in cui si lascia

al Governo. Ci tengo, in conclusione, signor Presidente, a ricordare Berlusconi combattente della politica, che ha sempre e comunque rispettato tutti gli avversari politici, che nessuno di noi doveva avere dei nemici personali, nessuno di noi che militavamo nel suo partito doveva avere problemi personali con chi non la pensava come noi. Noi difendevamo le nostre idee, ci confrontavamo con gli avversari, combattevamo contro idee e proposte, ma mai contro la persona. Lui ha sempre rispettato tutti gli avversari, pur con la forza e la determinazione del *leader*, del combattente, dell'uomo di Stato che metteva - ripeto - sempre al centro la persona. Un ultimo ricordo, signor Presidente: l'incontro con il comitato di fabbrica della Gilera, società in crisi all'epoca, nel 1994. Ricevette il comitato di fabbrica della Gilera nello stesso salotto e con lo stesso trattamento che riservava ai Capi di Governo, ai grandi *leader* che lo andavano a trovare, proprio perché considerava ogni persona che aveva di fronte un essere umano, un mondo che andava rispettato e che in quel momento per lui era la persona più importante. importante. Durante tutta la sua azione di Governo ha seguito questa linea. Lo ricordiamo e lo ricorderemo come un uomo di Governo e un uomo di Stato, ma soprattutto come

Signor Presidente, non parlerò a braccio e me ne scuso, ma oggi non ne sono capace. L'emozione e la commozione prenderebbero il sopravvento il presidente Berlusconi mi ha insegnato che nelle occasioni solenni bisogna sempre leggere. Questo è un giorno solenne e io, nel dolore, voglio onorarlo come merita, perché il destino ha voluto che toccasse a me. La vita lunga e inimitabile del presidente Berlusconi è talmente densa di fatti che giudicarlo col metro delle categorie comuni sarebbe un esercizio senza senso. Era un genio, già entrato nei libri di storia prima ancora di lasciarci come condottiero delle imprese impossibili. Parliamo di un uomo, di un figlio, di un padre, di un nonno, di un imprenditore, di un *leader* politico straordinario. Straordinario per noi che l'abbiamo amato, seguito, che abbiamo creduto in lui, ma straordinario per tutti, perché era fuori dall'ordinario. Ha rivoluzionato il mondo dell'imprenditoria, il mondo dello spettacolo, il mondo dello sport, quello della politica, ma soprattutto Silvio Berlusconi ha amato gli italiani. Li ha amati così, senza pretendere di cambiarli o impartire loro lezioni, cercando piuttosto di cambiare in meglio le loro condizioni di vita. Voleva cambiare l'Italia e lo ha fatto, eccome, ma mai gli italiani. Per questa profonda sintonia con le persone, per questa comprensione intima del loro carattere, delle loro aspirazioni, delle loro possibilità, Silvio Berlusconi ha amato ed è stato amato. Oggi qui in Senato merita di essere ricordato, però, non solo come l'uomo che monsignor Delpini ha colto nella sua essenza, ma come l'uomo di Stato che gli italiani hanno conosciuto, scelto e amato. Si pensa spesso che essere uomini di Stato abbia a che vedere con il prestigio dell'incarico che si ricopre, ma essere uomini di Stato significa innanzitutto essere uomini, essere persone al servizio dello Stato. Silvio Berlusconi è stato un uomo di Stato, perché sapeva percepire il polso della vita pubblica, sentirne il battito anche sotto i marmi, gli stucchi, le liturgie e il fasto. Uomo di Stato, persona dello Stato è chi non dimentica mai chi sia lo Stato, cioè i suoi cittadini, con la loro esistenza semplice e dignitosa, con le loro ansie, le attese, gli affanni, le gioie. Essere uomini di Stato significa sentire profondamente la voce, la fiducia, il respiro della democrazia. Questo sentimento è quello degli uomini di Stato, delle persone che si sentono parte e non sono solo di parte e che non mettono un diaframma, una distanza tra loro e gli altri, non si proteggono dagli italiani, non ne temono le speranze, non ne evitano il contatto, non ne dimenticano le richieste. Non sono gli incontri con i grandi della Terra o i vertici internazionali a farne uomini di Stato; sono la fiducia e il mandato che i cittadini conferiscono loro. Non è il senso di sé a fare un uomo di Stato, ma il sentimento del «noi», di una forza e di una speranza che ci accomuna; non è la sospensione del giudizio a fare un uomo di Stato, ma la passione civile, non la cautela ma il discernimento, non l'ipocrisia ma il parlare chiaro. Essere uomini di Stato è anteporre sempre il bene del Paese, l'interesse primario e superiore dei cittadini, rinunciando anche a pezzi di consenso, come ha saputo fare lui. Silvio Berlusconi è stato tutto questo. Aveva un dono raro: quella capacità di infondere coraggio nelle persone, di spingerle a superare le sfide più imponenti. La sua *leadership* non ha solo segnato la vita e la carriera di molti di noi, ma ha lasciato un'impronta duratura sulla vita politica italiana e ha davvero cambiato l'Italia. Per me, per noi che siamo sempre rimasti al suo fianco dal primo all'ultimo giorno della sua unica esistenza, con lealtà e coerenza assolute, per quella stragrande maggioranza del popolo italiano che ha riposto in lui ogni fiducia per un futuro all'insegna del riscatto e della dignità, per questa comunità di persone che oggi si ritrova improvvisamente orfana, il presidente Berlusconi continuerà a rappresentare una luce. Lui non sapeva neanche dove fossero di casa l'invidia e l'odio. Non serbava mai rancore. Non conosceva la vendetta, malgrado le ingiustizie subite, risollevandosi ad ogni caduta, lottando fino all'ultimo respiro contro le condizioni avverse, i cattivi presagi, riemergendo, sempre e comunque, grazie a quell'amore innato, folle per la vita, di chi ha sempre tenuto orgogliosamente il sole in tasca. Sapeva trasformare un male in un bene. Ripeteva sempre che una situazione negativa bisognava saperla trasformare, anche con sacrificio, in una nuova opportunità. Lui, vittima di decisioni ingiuste, in questo Senato è tornato da vincitore, con la fierezza e l'orgoglio di chi, anche in questo caso, non si è fatto piegare e con il tributo del Governo in occasione del suo ultimo discorso in quest'Aula. Silvio Berlusconi era, ed è, tutto questo e anche di più. La sua mancanza è un vuoto che sarà difficile da colmare, ma i ricordi e le lezioni che ci ha lasciato saranno un faro che continuerà a brillare e a guidare la nostra rotta. Quindi, grazie, Presidente, per tutto quel che ha fatto per noi, per il nostro Paese, per il nostro futuro. La sua dedizione instancabile, il suo amore per l'Italia, la sua fede nel popolo italiano sono un'eredità preziosa che ci ha lasciato. Il suo spirito continuerà a vivere nei nostri cuori, nelle nostre azioni e in quelli di chi continuerà a lottare per una visione dell'Italia migliore, che lei ha trasmesso a tutti noi. Ci ha mostrato che un futuro più luminoso era possibile e ci ha dato gli strumenti per raggiungerlo. Saremo all'altezza dei suoi sogni, perché non abbiamo altra missione che continuare a lavorare nel solco tracciato da lei, per un'Italia più bella, più forte e più libera. Per questo, al presidente Silvio Berlusconi oggi il suo Gruppo parlamentare, il suo partito, tributano l'onore della memoria e del rimpianto, del rispetto e del cordoglio per il *leader*, per l'uomo, l'imprenditore e il comunicatore, il politico e l'innovatore, per l'uomo di Stato e per l'uomo che è stato per la sua storia italiana. Per me, camminare al suo fianco, caro dottore, apprendere dalla sua saggezza, condividere vittorie e sconfitte, imparare a sorridere e a ridere degli insulti e dei feroci attacchi esterni, raccogliere le sue delusioni, fare tesoro delle sue più intime riflessioni è stato un privilegio assoluto, di cui sarò infinitamente grata alla vita. Ogni momento passato con lei è un ricordo prezioso, ogni lezione appresa un dono inestimabile. Ho potuto conoscere un uomo generoso, che sapeva entrare in sintonia con le persone. Sapeva star loro vicino, nelle gioie e nello sconforto. Sapeva dare sostegno quando ce n'era bisogno. Sapeva essere attento, sempre attento, non solo verso i suoi amici, ma anche a chiunque avesse la fortuna di incontrarlo nella vita. Per concludere, ora lo stiamo commemorando e non sembra neanche vero che al suo posto, al suo banco, non sia seduto lui, ma ci siano questi tulipani, fiori che lui adorava. Il Gruppo Forza Italia al Senato si stringe intorno ai figli, Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, ai nipoti, al fratello Paolo, alla sua Marta, agli amici di una vita, Gianni, Fedele e Marcello. E il nostro pensiero va lassù, dove ha potuto riabbracciare il suo papà Luigi, mamma Rosa, sua sorella Antonietta, Niccolò ed Ennio. Lo vogliamo ricordare così, come sempre diceva: «Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince». Buon vento, dottore. Buon vento, presidente. Buon vento, Silvio Berlusconi! la senatrice Ronzulli, che ha citato Marina, Pier Silvio, Barbara, Eleonora e Luigi, Marta Fascina e il fratello Paolo. Li cito di nuovo perché congiuntamente mi hanno chiesto di ringraziarvi - lo faccio già ora, in anticipo e hanno affidato a Gianni Letta il compito di rappresentarli qui, nel palco a lui riservato. Grazie, Gianni. *(Applausi)*.

Signor Presidente, altri colleghi hanno più titolo e più autorevolezza di me nel sottolineare le luci e le ombre di questa straordinaria personalità che ci ha lasciato. Desidero solo offrire una breve testimonianza personale. Penso che riconoscere che una persona ti ha cambiato la vita, in aspetti importanti, sia il massimo tributo che si possa dare dare a quella persona. Voglio dare la testimonianza, in particolare, dell'influenza che Silvio Berlusconi ha avuto sulla mia vita, introducendomi al servizio alla cosa pubblica. Un rapporto trentennale quello tra il presidente Berlusconi e me, intercorso tra due persone profondamente diverse, oltre che di rilievo ovviamente incomparabile, ma accomunate da due elementi. In primo luogo, avevamo visioni della società e dell'economia abbastanza simili, ma che ancora nella metà degli anni Novanta in Italia erano minoritarie. In secondo luogo, ci saremmo trovati a confrontarci, ma in realtà soprattutto a collaborare, in alcuni momenti drammatici per l'Italia e per l'Europa. Il primo segno di consonanza nella visione fu pronunciato proprio in quest'Aula, il 16 maggio 1994, dal presidente del Consiglio Berlusconi, nelle dichiarazioni programmatiche del suo primo Governo. Qualche giorno prima, sul «Corriere della sera», avevo auspicato che il Governo ispirasse la sua azione a un «liberismo disciplinato e rigoroso», cioè - precisavo - attento al bilancio pubblico, alla concorrenza, ai conflitti di interesse. Nelle sue dichiarazioni, da quel banco, Berlusconi riprese quelle parole, citandone la fonte, e si professò anch'egli «fautore di un liberismo disciplinato e rigoroso». Forse a seguito di quella sintonia, poco dopo il presidente Berlusconi, senza che ancora ci fossimo mai incontrati né parlati, propose la mia designazione a Commissario europeo. Con questa decisione, Berlusconi davvero cambiò la mia vita. Come economista, sentivo la vocazione a incidere sulle cose, a cambiare la realtà, e di Europa ero appassionato fin dall'adolescenza, ma non mi attirava minimamente la vita politica, l'appartenenza a un partito. Per questo avevo declinato negli anni varie proposte di candidatura alle elezioni o di entrare a far parte di alcuni Governi, pur molto qualificati. Quello che mi proponeva Berlusconi era diverso: partecipare al governo dell'Europa - la Commissione - ma senza necessità di far parte di una formazione politica. Per questo accettai volentieri, immediatamente e con Devo dire che Berlusconi fu sempre rispettoso del mio ruolo di commissario, sia allora, sia nella Commissione successiva presieduta da Romano Prodi, quando venni confermato dal Governo D'Alema. Per avermi avviato sulla strada d'Europa serberò per il presidente Berlusconi sempre viva riconoscenza personale. In conclusione, signor Presidente, vorrei oggi esprimere anche una riconoscenza a titolo istituzionale, come presidente del Consiglio che prese da lui il testimone nei giorni difficili che la politica e l'economia italiana attraversarono nel novembre 2011. A differenza che nel 1994, non fu Berlusconi a scegliere la mia persona per quella responsabilità che avrebbe fatto tremare le vene ai polsi a chiunque (e lo fece ovviamente anche a me). Non fu lui, bensì furono il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e il Parlamento con una vastissima maggioranza. Ma Berlusconi non oppose ostacoli; anzi, pur trovandosi in una situazione comprensibilmente molto difficile, con il venir meno della sua maggioranza e consapevole dei gravissimi rischi che incombevano sulla credibilità dello Stato italiano, sull'euro, sulle imprese e sull'economia italiana, contribuì a quella transizione con senso di responsabilità. Con il suo Popolo della Libertà fu anzi partecipante di maggioranza a quell'opera di Governo. Fu un percorso difficile, affrontato con grande senso di responsabilità dal presidente Berlusconi saluto con gratitudine per quella e altre circostanze il dottor Gianni Letta - così come fu affrontato con altrettanto senso di responsabilità dall'onorevole Bersani e dal presidente Casini. Ci furono amarezze da una parte e dall'altra, ma devo dire che il rapporto col presidente Berlusconi, al di là di certe apparenze, è sempre stato di grande lealtà, credo reciproca. In questo momento in cui ci ha lasciato - concordo nel dire che lascia una traccia grandissima e indelebile ho voluto rendergli questo omaggio personale, sicuro che ci ascolta.

Signor Presidente, le sono grato di avermi consentito a titolo personale di rendere omaggio alla memoria di Silvio Berlusconi. Con lui ho condiviso un lungo tratto della mia vita politica. L'ho conosciuto negli anni Ottanta, da giovane deputato della Democrazia Cristiana. Ho partecipato ai momenti fondativi del Polo della Libertà nel 1994. Dalla sua maggioranza sono stato proposto a guidare nel 2001 la Camera dei deputati; tutto questo fino alla rottura del 2008, quindici anni fa, a cui è seguita la mia opposizione al suo Governo nel corso della XVI legislatura. È evidente che le nostre idee non sono state sempre assimilabili, in molti passaggi sono state assai diverse, ma oggi non è il momento di questa contabilità. Oggi è il congedo che amici e avversari, uniti in un'idea civile del confronto politico, rendono al collega senatore. È stato il Presidente del Consiglio più longevo del Dopoguerra: basterebbe questo per capire quanto profonda sia stata la sua sintonia col corpo elettorale, quanto radicata in lui la consapevolezza di rappresentare una parte del nostro Paese. Gli faremmo un torto, però, se in questo momento, sull'onda delle emozioni, non lo ricordassimo per come è stato davvero: un uomo che voleva piacere anche ai più distanti da lui, ma che in molti passaggi della vita repubblicana è stato assai divisivo. Proprio per questo la sua figura ha plasmato il bipolarismo italiano, non solo le coalizioni di centrodestra della cosiddetta Seconda Repubblica, ma indirettamente le stesse alleanze politiche che a lui si sono contrapposte e che, proprio nel nome dell'antiberlusconismo, si sono cementate. Potremmo definirlo per questo il grande alibi, sì, il grande alibi della politica italiana: alibi per la sua coalizione, che spesso ha evitato di fare i conti con le proprie contraddizioni e i propri ritardi, poggiandosi solo sul suo carisma; alibi per gli oppositori, che hanno evitato di compiere scelte più coraggiose, crogiolandosi nel Sacro Graal dell'antiberlusconismo. Per questo oggi siamo più soli, nell'assoluta necessità di fare i conti con noi stessi, evitando la facile ricerca di capri espiatori. Berlusconi ha avuto il merito di favorire l'evoluzione della destra italiana, che ha con Fiuggi e con Fini riconosciuto il valore fondante dell'antifascismo; ha evitato una deriva secessionista della Lega, che è confluita verso un più consapevole federalismo; ha scelto l'Europa, rifiutando la trappola di sovranismi nazionali; ha tentato di associare la Russia all'Occidente e alla NATO, disegno cui tutti abbiamo creduto e che, purtroppo, è stato reso vano dagli irresponsabili comportamenti di Putin. Ha avuto, come tanti protagonisti della vita pubblica, meriti e anche demeriti. A me però piace ricordarlo, in conclusione di questo intervento, il 25 aprile ad Onna, in uno dei suoi momenti più alti cito le sue parole: «L'impegno che ci deve animare è quello di non dimenticare ciò che è accaduto qui e di ricordare gli orrori del totalitarismo e della soppressione della libertà». E ancora: «La Resistenza è - con il Risorgimento - uno dei valori fondanti della nostra Nazione, un ritorno alla tradizione di libertà». Sarà la storia, cari colleghi, come per tutti i grandi protagonisti, a dare un suo giudizio completo. Berlusconi è stato uno dei più significativi interpreti del nostro tempo. Infine, apro una parentesi personale. Alcuni di noi in quest'Aula ne hanno anche conosciuto i tratti umani, capaci di slanci generosi, di autentica amicizia, di sensibilità anche nei confronti delle persone più deboli. Proprio per questo mi unisco alla sua famiglia, ai suoi collaboratori, al suo partito, Forza Italia, esprimendo un sentimento autentico di cordoglio, di amicizia e di solidarietà.

Signor Presidente, colleghi senatori, colleghe senatrici, ringrazio l'opposizione che si è voluta alzare a tributare l'onore al presidente Berlusconi. Non avrei mai voluto essere qui in questo momento, perché è come se con oggi scorressero i titoli di coda; se solo da oggi ci si rendesse conto davvero che il presidente Berlusconi non c'è più. È stato da brividi prima vedere sul *display* che tra il mio cognome e quello del collega Bergesio non c'era più il suo. Ricordare il Presidente in cinque minuti è pressoché impossibile. Nel 2014 ho dedicato alla sua epopea, che ha caratterizzato gli ultimi quarant'anni del nostro Paese, un libro di 576 pagine e sto scrivendo il *sequel*, che non sarà meno copioso. Il titolo originale era «Il cuore oltre gli ostacoli. Nel sogno di Silvio» e credo che il detto popolare «gettare il cuore oltre gli ostacoli» sia l'essenza del berlusconismo, che sia stato il sentimento, lo stato d'animo, l'atteggiamento mentale che più ha caratterizzato Silvio Berlusconi fino all'ultimo respiro e che ci ha uniti in un *idem* sentire che lega indissolubilmente quelli che il Presidente del Consiglio, figli come me - come Matteo Salvini, Matteo Renzi e tanti altri - della Berlusconi *generation*, chiamerebbe gli *underdog*, cioè coloro che, partiti dal nulla, ce l'hanno fatta, in forza del coraggio, del lavoro, di sogni che a volte diventano contagiosi e sono in grado come nel caso del Presidente - di rivoluzionare ogni ambito di un Paese intero. Le meningi diventano le viscere del cuore, perché creare - come diceva Nietzsche - è l'unica liberazione dal dolore. Ecco, per non essere banale tra gli ettolitri di inchiostro versati in questi giorni per il Presidente, credo che proprio Nietzsche mi aiuti a definirlo: lui era l'uomo che parlava al sole, descritto nel libro «Così parlò Zarathustra», il sole in tasca, come ha detto la collega Licia Ronzulli. Zarathustra amava tutti gli animali, non riconosceva valore agli idoli e alla proliferazione delle loro immagini, e lottava dunque per la libertà dell'uomo semplice. Con la sua vita contesa fra storia e leggenda, si dice che nasca ridendo e ad ogni compleanno riderà, il tempo è per lui una danza di costellazioni amiche. Un ex giocatore del Milan ha detto qualcosa di più simile a quello che ho pensato io in questi giorni: l'ha chiamato «immenso Presidente»; lo l'ho chiamato «infinito Presidente», perché il suo modo di essere non è finito con la vita terrena, perché dal suo caos e dalla sua energia creatrice è scaturita la stella danzante e abbiamo ballato tutti insieme - l'economia, la politica, lo sport, le istituzioni, Paesi interi, l'Italia intera - un tango con lui di passioni assolute e contrastanti. Si dice che il suo lascito in politica sia l'unità della coalizione e l'invenzione del bipolarismo. Io credo che il suo lascito più grande sia la fede nella speranza, che la politica dovrebbe sempre ingenerare e di cui l'umanità, in un'epoca di relativismo valoriale e culturale, di solitudine, sente un grande bisogno. E credo che lui stesso incarnasse il bipolarismo in grado com'era Grazie a tutti poteva cambiare la storia di un Paese stanco, riverso su se stesso, dal quale esalava un'ansia di rinnovamento. Silvio Berlusconi ha sfidato i confini dell'ordinario, creando una narrazione epica che ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana e che l'Italia gli ha riconosciuto con una commozione profonda, con un funerale degno di un padre della Patria come è stato lui; non Presidente della Repubblica con i galloni istituzionali eletto dal Parlamento, ma dal cuore degli italiani. Un'amica d'infanzia che non c'entra nulla con la politica e che però è la cifra degli italiani ieri mi ha detto: l'Italia sembra orfana senza di lui; c'è un vuoto abissale che fa paura, come se fosse venuto meno un un punto di riferimento. È quello che proviamo tutti noi che abbiamo avuto l'onore di viverlo nella sua grandiosità e nella sua complessità. Lui era quello che una volta si sarebbe chiamato un condottiero: trascinava le folle con un carisma inconfondibile, incarnando l'essenza del *carpe diem*. Le sue parole, sempre affabili ma dirette, erano capaci di trafiggere le convinzioni

o quasi. Silvio Berlusconi è stato un eroe moderno. Come ogni grande protagonista, ha lasciato un'eredità complessa e duratura, una storia scolpita nella pietra del tempo. Come state capendo, ci sto girando intorno, perché in realtà affondare nei miei ricordi personali - tanti - fa molto male. Quello descritto fin qui è il Berlusconi pubblico, quello per lo più che si troverà sui libri di storia. Ma c'è un Berlusconi privato che ho avuto la fortuna di vivere e, con Frattini, è stato la mia famiglia. Quindi comprenderete che per me, a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, è un dolore difficile da tradurre. Mi ero voluta autoconvincere in quest'ultimo anno che il Presidente, al quale, nonostante la confidenza e la vicinanza ho sempre dato del lei per il rispetto che nutrivo nei suoi confronti, mi fosse uscito dal cuore. Ma non era affatto vero. Tra gioie e dolori, tra epiche baruffe e slanci da affetta assoluto, tra rabbia infinita e profonda gratitudine, la sua morte è stata come un soffio di respiro fuggito via, di quelli che fermano il cuore, che rimbombano nel silenzio, che ti tagliano le gambe. Ho conosciuto Silvio Berlusconi a Macherio: mi mandò a chiamare tramite Sandro Bondi perché voleva conoscere quella ragazza che - mi disse - aveva tinto d'azzurro l'Alto Adige italiano. Lo aveva raggiunto l'eco delle mie vittorie nel segno del berlusconismo più ortodosso. Trovai un Presidente molto diverso da quello che immaginavo: depresso, giù di morale per le tante cause giudiziarie, ma soprattutto perché, leggendo i giornali, credeva di non essere compreso dagli italiani, in tutto lo sforzo e il sacrificio che ci metteva alla guida del Governo. Ma quando uscii da lì, dopo che punto su punto rintuzzai le sue errate credenze e dicendogli che io sentivo la pancia della gente, perché ero sempre per strada anticipando la stagione dei gazebo, aveva un sorriso a trentasei denti. Io e lui insieme ai bei tempi, quando potevamo, eravamo come la nitro e la glicerina, un'esplosione di lucida follia. Dopo quell'incontro voleva nominarmi portavoce nazionale del partito, perché secondo lui avevo presenza e passione. Ma io declinai la proposta perché non mi sentivo preparata. Lui rimase colpito dal mio diniego, perché tutti andavano da lui solo per chiedergli posti e incarichi, mi disse. Da allora ci siamo fusi in un abbraccio costante e travolgente. Non feci il portavoce ufficiale, ma sono stata sempre in trincea e in prima linea per lui su tutte le reti televisive e tv, su tutti i media possibili e immaginabili, a cuore aperto, senza paura, difendendolo da accuse infamanti e ricevendo minacce di morte e insulti di ogni tipo, pagando con la mia stessa salute. Ma non me ne sono mai pentita. Capisco che c'è poco tempo. Voglio semplicemente dire che nel 2013 gli scrissi una *mail*, quando si formò il Governo Letta, dicendogli... *(Il vado a finire, Presidente - ...che sarebbe stata la cronaca di una morte annunciata, vedendo le persone che aveva indicato in quel Governo. Qualunque persona probabilmente si sarebbe adirata e mi avrebbe come dire - sbattuto la porta in faccia; invece lui mi nominò Sottosegretario, ruolo dal quale mi dimisi proprio in protesta di quella sentenza del 1° agosto 2013. Quel Natale c'ero io accanto a lui e e lo trovai con le mani nel volto. Mi chiese perché gli stavano facendo questo, perché quel torto, dopo che aveva dato tutto se stesso per questo Paese. Ebbene, io non seppi dargli una risposta, ma oggi spero che chi è stato reo di quel dolore, che lo ha portato a non essere più il Presidente con il sorriso che abbiamo tutti conosciuto, si batta il petto, perché, con molta probabilità, è stato anche concausa del suo dispiacere e della sua salute. Voglio solo ricordare - e concludo, Presidente - una giornata in cui era presente anche il dottor Letta, per me preziosa, che è stata l'ultima che abbiamo passato insieme a Merano, in cui, come due matti, io, lui e sua figlia... PRESIDENTE. Siamo in diretta televisiva e la prego di rispettare ...abbiamo passato una giornata straordinaria. Concludo veramente, Presidente. Lo dico perché quel giorno è stato un Berlusconi che si è offerto... *(Il microfono ...con tutta la sua generosità, come sempre. e voglio ringraziare l'Italia intera per la commozione che gli è stata tributata e per la vicinanza, che risponde più di mille parole a quelli che non hanno saputo capire chi era Silvio Berlusconi e quanto era stato amato.

Signor Presidente, ricordiamo oggi un uomo e un *leader* politico che, senza dubbio, è stato per lungo tempo tra i principali protagonisti della vita pubblica di questo Paese; un uomo politico che è stato anche, per la sinistra italiana, non solo un avversario, ma il principale avversario nell'arco di molti decenni. È giusto farlo, naturalmente. Ma, seppure penso che anche il giudizio più critico debba sempre pagare un tributo al turbamento della morte, non credo sia utile da parte mia limitarmi al solo cordoglio e alle condoglianze alla sua famiglia e alla sua comunità politica, che pure ovviamente rivolgo sentitamente, a nome mio e del Gruppo che rappresento. Farò oggi anche qualche considerazione più politica, a maggior ragione perché ritengo - e lo dico senza ipocrisie e spero con serena chiarezza - che non sia stato affatto giusto e nemmeno accettabile trasformare i funerali di un *leader* dichiaratamente di parte, la figura più divisiva forse di ogni epoca della Repubblica, in una cerimonia di santificazione quasi pagana, usata per celebrare ed esaltare, attraverso il *leader* scomparso, i suoi eredi politici oggi al Governo. È per questa ragione che abbiamo considerato inopportuna la proclamazione del lutto nazionale. La storia la scrivono i vincitori, come sempre. Eppure, io penso che cose del genere non debbano succedere in una democrazia compiuta. Come penso non possa succedere - come invece è stato - che la televisione pubblica si sia piegata così clamorosamente a una narrazione di parte, suggerita e alimentata dalle leve del potere politico. Da Silvio Berlusconi ci divideva tutto e io non voglio nascondere ora, nel momento di un lutto che pure ovviamente rispetto, quello che ho sempre pensato e che ho sempre detto. Ci divideva tutto, perché consideravamo e consideriamo Berlusconi portatore di un disegno politico regressivo, un disegno potente e seduttivo, fondato sulla cultura del mercato, che ha egemonizzato e trasformato la società italiana, chiudendo definitivamente l'epoca delle conquiste sociali, dei movimenti, del Sessantotto. Avevamo visioni della società opposte. Berlusconi credeva nelle magnifiche sorti del mercato e contrastava qualsiasi forma di regolamentazione. credo invece che, nell'assoluta libertà del mercato, non ci sia nessuna saggezza e senza un intervento regolatore, a pagare i prezzi sono sempre i più deboli. Avevamo concezioni della politica totalmente divergenti. Berlusconi, abilissimo comunicatore, ha svolto un ruolo impareggiabile nel potenziare l'aspetto pubblicitario e propagandistico della politica. E anche questo ci divideva. Quel modello egemone, perché rapidamente adottato anche da molti dei suoi avversari, a nostro parere ha grandemente impoverito la cultura politica di tutti, della destra come della sinistra. Questa distanza incolmabile non ci impedisce tuttavia di riconoscerne la sua centralità non solo come imprenditore, ma anche come *leader* politico. In questi giorni molte figure che pure lo avevano combattuto hanno riconosciuto le sue doti umane, la capacità di empatia, per esempio. Hanno fatto bene perché neppure la più radicale contrapposizione dovrebbe accecare e spingere a demonizzare l'avversario. Berlusconi ha creato una destra politica che prima di lui non aveva mai avuto ruoli rilevanti. La destra che oggi è al potere del nostro Paese non è stata e non è la destra liberale nella quale molti all'inizio hanno sperato; non poteva esserlo perché non si può svolgere contemporaneamente il ruolo dell'uomo di affari che tutela il proprio interesse innanzitutto e quello del politico liberale. Sino all'ultimo Silvio Berlusconi è rimasto prima di tutto un uomo d'affari, senza che il suo conflitto di interessi peraltro fosse risolto anche per responsabilità della sinistra politica, proiettando questa sua caratteristica sul mutamento sociale e democratico del Paese. La sua destra non è stata tuttavia animata da uno spirito sovranista. Non era comunque poco e io mi auguro davvero che i suoi eredi non lo tradiscano proprio su questo punto. Sarebbe ipocrita smussare adesso le critiche che gli abbiamo sempre rivolto, i legami opachi, i rapporti a volte innominabili, le amicizie imbarazzanti, la legittimazione della mercificazione dei corpi delle donne. Sarebbe per me sbagliato non sottolineare che oggi l'Italia non è certo un Paese migliore di trenta anni fa. per me altresì ipocrita non vedere che spesso gli avversari lo hanno combattuto con argomenti che hanno fatto, a loro volta, danni alla nostra cultura politica. Invece di contrastare le politiche di Berlusconi e della sua destra, si è scelta per troppo tempo una scorciatoia, peraltro inefficace; forse perché nella pratica si adottavano invece le sue stesse formule politiche, subendo l'egemonia di quel pensiero liberista che ha goduto di un sostegno trasversale ben oltre i confini delle sole destre politiche. Ci siamo raccontati che l'affermazione della destra fosse conseguenza solo delle capacità seduttive del suo *leader* o del controllo delle sue televisioni. tutte cose - sia chiaro - che io penso abbiano giocato effettivamente un ruolo. Ma Berlusconi ha dato anche risposte, per noi sbagliate naturalmente, a esigenze che invece erano reali. Senza quella sintonia, non sarebbero bastate le doti di comunicatore e nemmeno le televisioni. Penso allora che il compito di chi lo contrastava a viso aperto avrebbe dovuto essere sempre quello di non limitarsi all'anatema, ma di capire quelle domande per offrire diverse risposte, anche opposte. un'ultima considerazione: Berlusconi - credo questo gli vada riconosciuto - non era un imprenditore della paura, uno dei tanti cioè che montano emergenze inesistenti per poi lucrare politicamente sui timori irrazionali. La sua propaganda era opposta: faceva leva sulla speranza e sull'ottimismo, anche se questo spesso strideva con il Paese reale e le sue condizioni. In ogni caso, però, raccoglieva consenso non agitando lo spettro di un futuro peggiore, ma promettendone uno migliore. Questa, dal mio punto di vista, è una differenza non certo secondaria tra la sua destra e quella oggi al Governo, perché la politica deve saper far leva sulle speranze e sui sogni e non invece sulle paure e sugli incubi.

Silvio Berlusconi è stato senza dubbio uno dei grandi protagonisti della vita politica e sociale di questo Paese. La sua costante presenza ci faceva quasi credere che fosse immortale. Anche se tutti sapevamo dei suoi problemi di salute, la notizia della sua morte ci ha colti di sorpresa. Oggi siamo qui per commemorarlo, ma non siamo in un luogo di culto: siamo in Parlamento, il che impone di deviare dal *de mortuis nihil nisi bonum* per esprimere sincere considerazioni politiche. Io devo ammettere che nel mondo tedesco non era facilmente comprensibile che una figura come Berlusconi sia riuscita per quattro volte a fare il Presidente del Consiglio. Nella nostra concezione, il privilegio di guidare un Paese si accompagna alla necessità assoluta di affrancarsi dai propri interessi economici per perseguire solo il bene pubblico: cosa che di Berlusconi, con tutta la buona volontà, non si può dire. Dai politici di alto livello si pretende che siano un modello nel rispetto delle regole: Berlusconi non lo era. Diceva di essere un liberale, ma temo che questo per lui significasse soprattutto non attenersi alle regole, perché c'era ben poco di liberale nella sua impostazione sui diritti civili e su una politica economica che invece era caratterizzata dal protezionismo di certe categorie. La riprova sta nel fatto che nessuno ricorda una grande riforma nata nei suoi dieci anni di Governo. Dov'era allora il segreto di Berlusconi che riusciva a farsi perdonare dagli italiani gli errori, le promesse non mantenute e soprattutto le minacciose esternazioni contro giudici e giornalisti sgraditi? La spiegazione non può essere solo il suo potere mediatico e le sue sconfinate possibilità economiche. Mi convince la spiegazione che nella prima Repubblica i *leader* politici ambivano a mostrarsi migliori dei cittadini che andavano a rappresentare. Berlusconi invece si è mostrato come uno di loro, o meglio come uno che loro volevano essere. Ha in qualche modo umanizzato la politica, ma l'ha spinta anche verso un populismo dall'alto che poi ha fatto da modello a figure come Trump. Poi quelli che lo conoscevano di persona lo descrivevano come uno molto empatico, sempre attento, generoso, che dava a ogni interlocutore la sensazione di essere importante come pochi altri. Questo però non toglie che fosse una persona divisiva come poche altre. Anche dopo la sua morte, il Paese rimane spaccato tra berlusconiani e anti-berlusconiani e ci vorrà una generazione di storici per trovare un'inquadratura che metta tutti d'accordo. Come femminista non posso non ricordare che con il suo approccio patriarcale, le sue esternazioni e le sue cosiddette cene eleganti abbia fortemente danneggiato l'immagine della donna italiana.

Per quel che riguarda il rapporto con le Autonomie speciali, la testimonianza più autorevole è quella del nostro longevo presidente di Provincia Luis Durnwalder, che dice che da Presidente della Provincia ha incontrato 17 Presidenti del Consiglio e Silvio Berlusconi era il più divertente. Ricorda che diceva sempre di sì, che si parlasse di concessione della A22 piuttosto che di finanza locale o delle competenze delle Regioni; tanto che quando tornava a Bolzano aveva l'illusione di aver ottenuto risultati importanti. Ma capì che si sbagliava: alla nostra autonomia non ha tolto, ma non ha neppure dato niente.

l'adesione totale ai valori del popolarismo europeo e il suo costante impegno a tenere il centrodestra ancorato allo schema europeo. Io non l'ho mai conosciuto personalmente *(Commenti)*. Ma, Ma, se c'è un'altra cosa che ho apprezzato, è stato il suo amore per gli animali: vederlo circondato dai suoi tanti cani mi ha sempre fatto tenerezza. Eravamo abituati a un Berlusconi che dopo ogni caduta si rialzava. Purtroppo questa volta non sarà così e allora non ci resta che rinnovare il nostro cordoglio alla famiglia, ai suoi cari e al suo mondo politico.

Signor Presidente, non è possibile avere un giudizio uniforme e condiviso della figura storica di Silvio Berlusconi. è un dato di fatto di cui dobbiamo prendere atto ed è anche la grandezza di una persona che ha segnato la vita politica della Seconda Repubblica come nessun altro. La sinistra, sia quella che lo ha contestato, sia quella che lo ha odiato, deve riconoscere in Silvio Berlusconi un *unicum* nell'edilizia, nell'editoria, nella comunicazione, nella televisione, nello sport, nelle forme della politica; nel fatto che egli è stato - come veniva ricordato anche prima - il Presidente del Consiglio più longevo della storia repubblicana

Dall'altro lato, però, questo tratto di unicità porta anche la destra a dover fare i conti con una vera e amara realtà: il dibattito sull'eredità di Silvio Berlusconi non ha senso di esistere. Proprio per le sue caratteristiche di unicità, non c'è un erede possibile per Silvio Berlusconi. Egli ha degli eredi, i figli, cui rinnovo la mia e nostra solidarietà, vicinanza e il sentimento di condoglianze. Silvio Berlusconi ha un grande lascito anche nel mondo professionale: Mediolanum, Mondadori, Mediaset. Pronuncio i nomi delle principali aziende perché sono per noi un patrimonio nazionale e ai *manager* va l'augurio di buon lavoro, nel solco di una complessa situazione. Tuttavia, togliamoci dalla testa che qualcuno possa raccogliere l'eredità politica, perché Berlusconi era più grande dell'eredità politica che qualcuno vuole raccogliere. Se vogliamo essere coerenti con un dibattito politico vero, anziché fare ciascuno una sfilza di ricordi che sono comprensibili e umani e che naturalmente fanno bene al cuore e all'anima, ma che non colgono il punto politico - mi rivolgo al ministro Salvini, al ministro Salvini, che interverrà, e al presidente del Consiglio Meloni, che è intervenuta - se vogliamo davvero cogliere l'eredità politica di Berlusconi ricordiamoci che nel 1998, in un momento di sua difficoltà, quando ha perso le elezioni ed è oggettivamente l'uomo che prima le ha vinte, anche su un'alleanza complessa al Nord e al Sud con due forme di coalizione diverse, in quel momento sceglie la strada del popolarissimo europeo. Lo fa insieme a Kohl e ad Aznar, con la con la regia di un giovane spagnolo che si chiama Alejandro Agag; lo fa facendo arrabbiare tutti noi - guardo qualche amico - che stavamo nel Partito Popolare Italiano, perché lo sposta a destra, ma entra in una grande famiglia europea. Secondo me questo è un punto politico sul quale dovreste riflettere da qui al 2024. Ha un senso l'esperienza della destra in questo Paese se è collocata in una grande famiglia europea. Dall'altro lato, vedo che c'è una gara a inaugurare opere e infrastrutture. Credo che Berlusconi lo apprezzerebbe molto per quello che l'ho conosciuto, che sia il Ponte sullo Stretto, un aeroporto o una via. C'è però un dato di fatto: intestategli un grande risultato nella prossima legge di bilancio, ossia l'abbattimento delle tasse. Berlusconi ha sempre teorizzato una rivoluzione liberale, anche in questo caso innovando nelle forme e nei contenuti della politica rispetto alla tradizione italiana, ma non sempre è riuscito a raggiungere i risultati. Di conseguenza, se volete davvero tenere alto il ricordo di Silvio Berlusconi, fate una legge di bilancio che abbatta le tasse come egli, per una intera esperienza di vita, ha voluto e ha cercato di fare, e in alcuni casi lo ha fatto, ma non sempre, anche se era il vero cardine della sua rivoluzione liberale, insieme alle battaglie sulla giustizia, sulla libertà e a quello che sappiamo. Questo è il modo per ricordare Silvio Berlusconi, la cui eredità è, per chi lo ha conosciuto, anche un elemento personale. Io venivo da un'esperienza in cui il mio rapporto con Berlusconi era traviato dal fatto che avevo iniziato a fare politica contro Berlusconi e il berlusconismo. Io venivo da un'esperienza politica nella quale Berlusconi era il nemico, l'avversario. Conoscendolo, mi sono reso conto che alcune delle cose che noi utilizzavamo contro di lui erano false, erano banali. Gli dicevamo che il suo sorriso era di plastica, un sorriso non vero, un sorriso ipocrita. Quante volte abbiamo accusato Berlusconi di avere un sorriso televisivo? Conoscendolo, nel bene e nel male, scoprivi che Berlusconi era un uomo che aveva voglia di sorridere. C'è un'immagine, quella di una campagna elettorale difficile, del 2013. Berlusconi la perde per un soffio, ma per poco non riesce a fare il miracolo di pareggiarla, se non di vincerla. della cosiddetta non vittoria del Partito Democratico nel 2013. In quel passaggio lì, Berlusconi fa un capolavoro mediatico, andando in una trasmissione televisiva che lo detesta e pulendo con uno straccio la seggiola di un giornalista che aveva parlato prima di lui. Partono i fischi dello studio. Tutti iniziano a fischiare. Berlusconi si gira e prima si arrabbia, poi si gira e, con grande teatralità, dice che non sanno neanche sorridere. C'era gusto per la vita, per la provocazione, per l'ironia, per il piacere, qualche modo anche di provocare, che è un tratto caratteristico che Berlusconi aveva. Ma chi lo ha conosciuto, ha visto anche, in alcuni momenti, un tratto, che definisco non di depressione, perché non sarebbe corretto, ma di grande tristezza. Nei cosiddetti giorni del Nazareno, Berlusconi viveva un momento personale molto difficile. Tu parti dal presupposto che l'altro sia un avversario, quasi un nemico, e poi vedi quella persona vivere un momento di difficoltà e di complessità. Poi, però, lui usciva, naturalmente, con entusiasmo da tutti gli incontri e comunque, alla fine, non è il caso di parlare del patto del Nazareno: mi ha fregato lui, ma questo lo sappiamo tutti. Il punto vero è che non importava nemmeno non crederci, perché la grandezza di Berlusconi, quando raccontava una cosa che non era del tutto vera, non era quella di farla credere a te, ma che anche lui credeva nella bugia che raccontava quando te la faceva credere. In questo, era un fuoriclasse assoluto.

poi andavi a vedere e agli incontri Berlusconi arrivava con gli appunti sottolineati, contestando il singolo punto, l'articolo X o un emendamento. Questo perché, evidentemente, avendo anche avuto tutto dalla vita, aveva la voglia di mettersi in gioco. Berlusconi è stato un uomo che è stato capace anche di commuovere e far commuovere, sia gli avversari che gli amici, anche in alcuni momenti personali. A me ha colpito, signor Presidente, quando è entrato in Aula nei primi giorni di questa legislatura. Lo abbiamo visto tutti, è inutile fare grandi giri di parole: camminava male, non camminava più come prima, non era il Berlusconi dell'inizio della sua vita o dell'inizio della sua attività politica. Ha raggiunto il suo banco, il banco dove oggi ci sono i tulipani e le rose, con un po' di fatica, quasi incespicando: Eppure, quando ha preso la parola e tutti noi ci aspettavamo l'*incipit*, anche perché si era a distanza di qualche anno dalla nota vicenda della legge Severino, egli ci ha un po' stupiti, nel dirci quasi saltellando, che era appena nato il suo diciassettesimo nipotino. Ecco, in questo senso, forse forse dovremmo tutti fare uno sforzo per accogliere l'altro, che sia avversario, che sia compagno di strada, che sia nemico, che sia amico. Dovremmo cioè capire che dentro l'altro c'è una dimensione di umanità, che talvolta, anche complici le esagerazioni di Silvio Berlusconi, ma in larga parte anche per effetto della polemica *ad personam* che gli è stata lanciata contro, noi non abbiamo colto della sua esperienza di vita. A me questo viene in mente pensando al mio incontro con lui, il primo,

umano e politico di grande importanza come Silvio Berlusconi: puoi dire tutto quello che vuoi, puoi avere tutti i lussi che vuoi, puoi avere tutti i patrimoni che vuoi, ma - come diceva un grande scrittore francese - il più grande lusso della vita sono i rapporti umani. È questo che io mi porto dietro di Silvio Berlusconi: uno statista, ma soprattutto un uomo capace di rapporti umani.

Signor Presidente, mi spiace che non tutti prendano la parola in quest'Aula, però è il bello della democrazia.

vado a braccio quando parlo di tutto, ma quando ci sono questioni affettive e personali è meglio scrivere quello che la mente ti ha portato a

ne hanno comunque dovuto riconoscere la rilevanza epocale, tanto che nei libri di storia si parlerà certamente di un'era berlusconiana, di un prima e di un dopo Berlusconi, tale e a tal punto profondo è stato il suo impatto sulla società italiana e sull'immaginario collettivo in tutti i campi: l'audacia, la passione, l'Italia è il Paese che amo, l'energia, la tenacia, la speranza e il sole in tasca. Ci sono, in particolare, tre concetti che ho provato a riassumere e che illustrano, a mio avviso, la sua vicenda umana e politica, unica e irripetibile. Il primo concetto è la libertà. Questa parola, a lui tanto cara, assume diverse sfumature, armonicamente collegate. Innanzitutto c'è la libertà economica, che il Berlusconi imprenditore ha incarnato perfettamente. Un uomo che, grazie alla propria iniziativa e alla propria determinazione, rischiando e mettendosi in gioco, riesce a costruire un impero industriale a partire dal nulla. Per redistribuire la ricchezza, prima bisogna crearla e penso che Berlusconi sia stato un esempio

contro i dogmi del pensiero unico e il monopolio della televisione pubblica. Oltre la libertà, voglio citare anche il concetto di normalità. Parlare di normalità a proposito di un uomo eccezionale e unico, come Silvio Berlusconi, sembra strano, eppure l'ho sentito anche da qualcuno prima di me: la sua capacità unica di entrare in sintonia con le persone comuni, di parlare un linguaggio che tutti potessero capire è stata una delle sue grandi forze, una forza che, non a caso, certa sinistra, intrisa di ideologia, non ha mai capito, ha sempre disprezzato e non ha mai compreso. Pur avendo raggiunto successo, ricchezza e poteri globali, Berlusconi non ha mai dimenticato le sue origini, non ha mai perso il contatto con la realtà, coi ceti popolari, con la casalinga e con l'operaio, che qualcuno invece ha perso di vista negli ultimi anni. Silvio li amava veramente, non li analizzava come una realtà da sondaggio, ma li sentiva. terzo concetto, dopo la libertà e la normalità, è il sogno. La politica è concretezza, è l'alta velocità, il Brennero, la TAV, il Ponte, la Napoli-Bari, la Brescia-Vicenza, ma è anche sogno. Silvio Berlusconi è stato un rivoluzionario capace di ispirare più generazioni.

a misura d'uomo e a misura di bambino, che è ancora lì da vedere. Ha inventato il centrodestra, ha inventato il bipolarismo. Ricordo ancora - me la sono riletta - la prefazione che Berlusconi scrisse all'«Elogio della follia» di Erasmo da Rotterdam. «Ad affascinarmi fu, in particolare, la tesi centrale della pazzia come forza vitale creatrice», ed è vero. «L'innovatore è tanto più originale quanto più la sua ispirazione scaturisce dalla profondità dell'irrazionale. L'intuizione rivoluzionaria viene sempre percepita al suo manifestarsi, dapprima come priva di buon senso, addirittura assurda». Solo in un secondo momento «si afferma, viene riconosciuta, poi accettata, perfino propugnata da chi prima l'avversava». Il sogno è qui. Ovviamente da Ministri abbiamo il dovere di sognare e di realizzare, associando speranza e concretezza. Il sogno è qui, nella sua irrazionalità, ma anche nella sua concreta potenza creatrice. La grandezza di Silvio Berlusconi non è disgiungibile dal suo tratto umano: ne hanno accennato in tanti. Irripetibile il legame per la sua mamma, per la sua famiglia, per la sua Milano, per il suo Milan. Lascia a tanti un grande vuoto. Ci mancheranno il genio, la guida, i consigli, il sorriso e i rimproveri. Tuttavia, il nostro dovere è portare avanti la sua straordinaria eredità di valori. L'Italia e il mondo di oggi non sono quelli della fine del secolo scorso, ma sono l'Italia del 2023, con altre sfide. La nostra epoca, purtroppo, è tutt'altro che pacificata. Berlusconi seppe ai suoi tempi, in politica estera, unico e ultimo, applicare quella flessibilità che è caratteristica dei *leader* autentici. La foto con Bush e Putin è qualcosa che rimane nei libri di storia, anche se c'è qualcuno che ancora ultimamente non ha capito l'approccio di Berlusconi, che era uomo di pace. Ho sentito dire anche qua che era divisivo. Le grandi personalità al mondo sono divisive, solo gli "amebi" mettono d'accordo tutti. Berlusconi voleva la pace, a costo di far passare se stesso e la sua comunità politica come l'esatto contrario. È nostro dovere, come Governo, perseguire ogni via che porti alla pace. Noi dobbiamo proseguire nella linea da lui tracciata, lo faremo come azione di una squadra di Governo che lui ha voluto, ha costruito e di cui era orgoglioso, fino all'ultima telefonata del sabato sera. Quindi, difendere la casa, frutto dei risparmi di una vita, difendere il diritto a una pensione dignitosa è quello per cui abbiamo lavorato con Silvio Berlusconi fino a pochi giorni prima del suo saluto. Io lo immagino quella stessa mattina, quello stramaledetto lunedì 12 giugno, col fascicolo in mano, col *dossier* sull'Europa, sulla Cina, sulla casa, sulle pensioni, sul lavoro, domandare: Matteo, cosa state facendo al Governo? Mi raccomando, avanti, fino all'ultimo secondo. Amava la vita in modo eccezionale. Difendere il lavoro e difendere i confini, lottare contro un fisco nemico,

una riforma che va fatta tutti insieme, perché ancora oggi troppi italiani innocenti pagano per errori, lungaggini e sciatterie giudiziarie di cui nessuno alla fine paga il conto. Su questo la riforma della giustizia va fatta per il bene non della politica, ma delle famiglie, degli imprenditori e dei cittadini italiani in genere, di qualunque idea politica. Sempre dalla parte dell'Occidente e delle democrazie liberali, per una politica aperta a tutti che parte dal basso. Da *leader* della Lega mi interessano poco le analisi di quel che sarà dopo. Coltivo ancora il presente, l'istante, quel che ancora c'è a tener viva non la memoria, ma quel mazzo di tulipani: mai mollare, mai arrendersi fino alla fine. Quindi, anch'io mando un abbraccio forte e sincero a tutta la sua famiglia, ai figli, ai nipoti, a Marta a tutta la comunità di Forza Italia che ha tutta la mia vicinanza. Nei Nei discorsi non si dovrebbe ripetere quello che ha detto qualcun altro, ma oggi non penso che sia una giornata di politica e vorrei ripetere quello che ha detto la senatrice Ronzulli nel suo intervento. Nella vita, anche se magari qualcuno ne sorriderà, ponetevi sempre dei traguardi ambiziosi ed elevati: «Chi ci crede combatte. Chi ci crede supera tutti gli ostacoli. Chi ci crede vince». Ciao Silvio, onore a te, grande italiano, amico mio.

Signor Presidente, il ricordo del senatore Silvio Berlusconi, imprenditore, per quattro volte Capo del Governo italiano, per il Partito Democratico non è una commemorazione formale, una commemorazione da lasciare ai verbali dell'Assemblea. La sua scomparsa, signor Presidente, chiude un lungo ciclo politico durato quasi trent'anni. Oggi è il giorno del ricordo, verrà di nuovo il tempo della polemica, del contrasto e dello scontro in Parlamento; dello scontro su leggi non condivise, dello scontro anche sull'agenda politica di questo Governo, che noi contrastiamo e che in questi giorni ha utilizzato anche storie del passato per rivendicare proposte delle quali oggi non parliamo, signor Presidente. Oggi, a nome del nostro Gruppo qui in Senato e dell'intero Partito Democratico, esprimiamo vicinanza e cordoglio alla famiglia, perché Silvio Berlusconi, oltre a essere un uomo politico, era un padre ed era un nonno. Comprendiamo il vuoto che lascia in chi gli ha voluto realmente bene, innanzitutto le persone nelle quali il profondo affetto, accompagnato al grande dolore, c'era e resterà per tutta la vita. Esprimiamo solidarietà alle migliaia e migliaia di cittadini che gli hanno sempre manifestato il consenso politico e che hanno creduto nel suo impegno, solidarietà che indirizziamo ovviamente ai colleghi senatori di Forza Italia, all'intero partito e alla coalizione della quale Silvio Berlusconi è stato fondatore e protagonista. Pur non condividendo la sua visione politica, sarebbe lunare non riconoscergli un ruolo di primo piano sulla scena politica e istituzionale italiana, sin da quando nel gennaio del 1994 annunciò il suo impegno politico. Una vita politica tra alti e bassi,

Berlusconi ha contribuito a costruire il centrodestra italiano, ma non è riuscito, com'è venuto fuori anche dagli interventi di altri colleghi dell'opposizione, a modernizzare l'Italia come avrebbe voluto e come aveva promesso. Ha indirizzato varie correnti del pensiero conservatore della destra italiana verso una cornice istituzionale, presidente La Russa, che ha trovato per il suo partito un ruolo importante di governo in Europa - richiamavano il senatore Monti e il senatore Casini - ma non per la sua coalizione, che in Europa resta divisa in tre blocchi contrapposti e rappresenta ancora oggi la maggiore contraddizione valoriale, in un contesto di politica estera che ha assunto, non i tratti della diplomazia tradizionale - lo ricordiamo tutti - in cui la forma coincide spesso con la sostanza, ma caratterizzata da una figura intesa nel suo insieme di legami stretti e personali. Non abbiamo dimenticato il suo impegno internazionale, i successi e i fallimenti, ma Pratica di Mare costituisce senz'altro un momento importante nel dialogo tra Est Abbiamo contrastato Silvio Berlusconi e la sua idea di Paese, la destra che ha costruito, la sua forza negli anni del consenso: lo abbiamo fatto quando era al suo apice, ma mai perdendo il rispetto dell'avversario e dell'Italia che ha rappresentato e rappresenta. Nel 1994 aveva annunciato la rivoluzione liberale che non si è mai realizzata. La coalizione costituita era partita prima dalla Lega secessionista al Nord - lo ricordava prima il senatore Renzi - e dagli eredi del Movimento sociale italiano nel Centro-Sud; poi negli anni ha prodotto un liberismo all'italiana e ha determinato oggi la nascita del Governo più a destra della storia repubblicana. Il fatto che la sua lunga parabola, quella di una destra che si professava liberale, moderata e conservatrice, si sia risolta oggi nel Governo più a destra della storia repubblicana non è un argomento polemico, signor Presidente. Sarebbe inopportuno e sbagliato oggi, ma è una riflessione che consegno a voi, alla destra che siede in Parlamento, perché con questa riflessione dovrete fare i conti voi almeno quanto dovremmo farli noi. Il liberalismo, oltre a sostenere la libertà individuale come principio fondamentale, professa l'importanza dello Stato di diritto in cui tutte le persone, compresi i governanti e soprattutto i governanti, sono soggetti alle leggi e non sono mai al di sopra di esse. Questo garantisce l'uguaglianza di fronte alla legge e il rispetto dei diritto fondamentali di tutti i cittadini. Il liberalismo, signor Presidente, promuove la tolleranza il rispetto delle diverse opinioni, culture, credenze; rispetta la diversità e la pluralità delle idee. Ciò si traduce innanzitutto nel rispetto dei diritti di tutti, non solo di pochi. Il liberalismo teorico, professato a piene mani nelle istanze programmatiche, si è tradotto alla fine in un liberismo a volte senza regole, a volte con regole personalizzate. Il rispetto che in questa sede desideriamo manifestare nei confronti Silvio Berlusconi non deve farci dimenticare che noi la pensiamo diversamente su molte Crediamo che lo Stato di diritto significhi pari condizioni di partenza per tutti e non l'esaltazione, nella legge fatta su misura, del più forte; e che le fragilità della nostra società debbano essere sempre compensate da un'azione vigorosa delle politiche pubbliche. Crediamo che pagare le tasse non sia un «pizzo di Stato», ma un atto di cittadinanza. Pensiamo che nessuno sia al di sopra della legge e che la magistratura debba agire sempre con l'autonomia garantita dalla Costituzione, fondata sul sangue della Resistenza. Quello che Silvio Berlusconi lascia sarà sicuramente un vuoto all'interno della vita pubblica italiana: di questo...

e a tutto il partito di Forza Italia auguriamo di proseguire nel suo cammino. Oggi è il giorno del ricordo e da avversari tributiamo l'ultimo saluto politico all'uomo che ci ha lasciato. Lo facciamo con rispetto, ma anche con la considerazione che l'idea di società che vogliamo è molto diversa dalla sua. Abbiamo molto apprezzato l'omelia dell'arcivescovo di Milano, signor Presidente; c'è chi l'ha percepita come un elogio di Berlusconi e chi l'ha percepita come una critica. Io mi ritengo, come tanti, un credente in cammino con molte fragilità, ma una cosa ho capito: quell'omelia vale per tutti, vale per tutti, per ognuno di noi. La vita ci fa andare per mille sentieri, ma poi alla fine ci porta al compimento del giudizio di Dio. Dio accoglie tutti noi peccatori, quelli che in vita hanno ceduto a scorciatoie o, come ha detto... hanno goduto il bello della vita. Per questo, dinanzi alla scomparsa di Silvio Berlusconi, pur ribadendo il nostro stare dall'altra parte, voglio concludere ponendomi e ponendoci umilmente in silenzio davanti al giudizio della storia,

Signor Presidente, è un momento che non avremmo mai voluto vivere quello di dover commemorare Silvio Berlusconi, del quale si potrebbero dire mille cose, ma in questo momento bisogna limitarsi ad alcune, ad alcune, tralasciandone tantissime altre: episodi, detti, ricordi. Berlusconi è stato un innovatore, prima ancora di essere un imprenditore; è stato naturalmente un un innovatore come imprenditore nei tanti campi in cui si è cimentato ed è impossibile citarli tutti. Nell'edilizia aveva una nuova idea di città: non i casermoni fatti per moltiplicare il numero di unità abitative a scapito dello stile di vita, ma il contrario. È stato un innovatore nelle televisioni, in modo straordinario e sconvolgente, tanto da sovvertire tutti i pronostici. È stato innovatore nel calcio,

servizi e idee: ad esempio, con le sue televisioni, servizi ai cittadini, cui forniva nuovi contenuti, come servizi agli inserzionisti, dando nuove opportunità ad essi e in particolare a quelle tante medie e medio-piccole aziende - la grande forza dell'Italia - che nel regime di di monopolio precedente avevano enormi difficoltà o erano impossibilitate ad ottenerle. Ha costruito la sua fortuna imprenditoriale grazie alle sue capacità di innovazione e non, come altri hanno fatto magari nei decenni, grazie a sovvenzioni e a prebende sotto vari aspetti. No, sempre e solo con le forze sue e dei suoi tanti collaboratori. Poi c'è stata la discesa in campo, la ragione per cui abbiamo avuto l'onore di averlo come collega qui al Senato, e di vederlo ricoprire cariche importantissime più a lungo di qualunque altro nella storia della Repubblica italiana. La sua discesa in campo fu dovuta a una straordinaria intuizione, a un'innovazione. Egli intuì e capì che c'era un popolo che si riconosceva in determinati valori, in determinati principi, in determinate idee e anche umori, che era compatibile con un'ampia area degli italiani. Capì che non era né giusto, né ragionevole non far partecipare gli elettori di destra, di quel Movimento Sociale che si stava trasformando in Alleanza Nazionale,

La stessa cosa capì che valeva per gli elettori della Lega, all'epoca presente solo nel Nord Italia. Anch'essi meritavano la possibilità, insieme ai tanti elettori del partito che lui fondò e che in due mesi portò a risultati straordinari (Forza Italia), (Forza Italia), di gareggiare per il Governo e più volte di arrivarci. Berlusconi è stato Presidente del Consiglio per tre volte. Ha guidato quattro Governi, ma dal 2001 al 2006 c'è stata continuità. E queste tre volte, guarda caso (sembra scontato, ma non lo è stato in molti altri casi), hanno coinciso con tre chiare vittorie elettorali, cosa che non è avvenuta per altri. Oltre a queste tre vittorie, c'è stata anche la vittoria del settembre scorso. La vittoria dell'attuale coalizione che ora vede al Governo il presidente Giorgia Meloni è è frutto dell'intuizione di Silvio Berlusconi, fondatore e *leader* a lungo del centrodestra, di questa idea del centrodestra. può essere portata anche a livello europeo. Se altri *leader* in Europa avessero avuto le stesse idee, le stesse intuizioni e la stessa capacità di amalgamare, ci sarebbero stati forse meno partiti estremisti e meno divisioni inutili anche in altri Paesi, con beneficio di tutti, non soltanto delle parti moderate, di centro destra e conservatrici (a seconda di come possono essere chiamate nei vari Paesi). Tutto questo, che è solo una piccola parte di ciò che si potrebbe dire, dice poco per i tanti di noi che abbiamo avuto la fortuna e l'onore di conoscere personalmente Silvio Berlusconi, perché il vuoto che lascia, lo straordinario messaggio e lo straordinario ricordo che lascia in ciascuno di noi non è solo negli straordinari traguardi che ha raggiunto nella politica, nell'imprenditoria e nello sport, ma il suo ricordo è soprattutto per la sua umanità, per la capacità - anche questo è stato detto, ma è giusto ripeterlo, perché evidentemente abbiamo un sentire comune su questo su questo - di mettersi in sintonia con ciascuno. Uno degli uomini di maggiore successo in assoluto in così tanti campi sapeva essere in sintonia con i Capi di Stato da una parte, ma anche con la gente più comune. Sapeva mettersi nei loro panni, sapeva lavorare con loro, sapeva capire le loro esigenze. Per questo molti, pur non avendolo conosciuto da vicino, l'hanno amato, perché comprendevano questa sua empatia e questa straordinaria umanità che ha sempre espresso. Ci mancherà moltissimo il presidente Berlusconi. Ci lascia però moltissimo, non solo l'eredità politica di cui ho parlato, ma un grande esempio, quella capacità di essere allo stesso tempo un combattente strenuo dal primo all'ultimo giorno del suo impegno politico e, dunque, all'ultimo giorno della sua vita, senza senza mai però avere parole di odio per nessuno, neanche contro coloro che l'hanno espresso, anche fin troppo recentemente, nei suoi confronti. il Gruppo Fratelli d'Italia si stringe ai colleghi e agli amici di Forza Italia, alla famiglia, a tutti coloro che sono stati vicino a lui, ai suoi tantissimi collaboratori e cito perché presente, uno per tutti, il dottor Gianni Letta. Aggiungo ancora un pensiero: grazie, presidente Berlusconi, per quello che hai fatto, per come sei stato, il tuo ricordo ci darà ulteriore forza nel lavorare per il bene dell'Italia che tu hai tanto amato.

Grazie a tutti per la compostezza e per i toni usati in questa commemorazione. Il Senato ha dato ancora una volta prova della propria natura. Grazie a tutti A tal fine per la seduta di oggi non è stabilito orario di chiusura. L'ordine del giorno della seduta di domani prevede la discussione del decreto-legge in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro. Dopo la discussione generale la seduta sarà sospesa, su richiesta del Gruppo Partito Democratico, per riprendere alle ore 13 con le votazioni degli emendamenti al decreto-legge. Per la seduta non è fissato orario di chiusura: tuttavia le votazioni potranno proseguire, ove necessario, nella seduta di giovedì 22 giugno. Il calendario dei lavori della prossima settimana reca invece la discussione dei seguenti argomenti: decreto-legge su amministrazione di enti pubblici e società, termini legislativi e iniziative di solidarietà sociale; ove richiesto dal prescritto numero di senatori, risoluzioni approvate dalla 3a Commissione sulla partecipazione dell'Italia a missioni internazionali; ratifiche di accordi internazionali; documenti definiti dalla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Come già stabilito, mercoledì 28, alle ore 15,30, si svolgeranno le comunicazioni del presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023.

proseguiranno nella seduta di martedì 4 luglio; diversamente, se cioè concludessimo tutti gli argomenti previsti, la settimana dal 3 al 7 luglio

la mozione sull'attuazione degli impegni previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e resilienza ha raccolto più di un terzo delle firme dei senatori e delle senatrici

e Sinistra abbiano deciso di trasformare la richiesta di chiarimenti fatta più volte al ministro Fitto nei mesi scorsi in un atto di indirizzo politico che non lasciasse spazio ad interpretazioni, che di solito vengono date - non me ne voglia il ministro Fitto - su impegni che quasi sempre coincidono con scadenze comunitarie. Siamo stati costretti, senza attendere la relazione semestrale, sull'esame della quale ci rivedremo sicuramente nelle Commissioni e in Aula nelle prossime settimane, perché riteniamo che, ad alcune settimane dalla scadenza che ci avvicinerà alla data del 31 agosto, le nubi siano aumentate e la piena attuazione del PNRR, che rappresenta anche per il Documento di economia e finanza una condizione per il rispetto dei numeri che caratterizzano le ipotesi di crescita del Paese, è ormai una chimera. Questo per le ragioni che lo stesso Governo ha dovuto ammettere nei dibattiti delle settimane scorse. È una chimera perché, vista l'impossibilità di poter intervenire direttamente su alcuni ambiti, il Governo ha deciso di smontarne la *governance* e di rimontarla senza aver ancora attivato

Nella mozione che abbiamo presentato, facendo riferimento espresso anche alle criticità sottolineate dalla Corte dei conti lo scorso 28 marzo, abbiamo messo in evidenza come quelle criticità

alcuni *target* rispetto alle *milestone* a cui il Governo avrebbe dovuto associare strutture e interventi (quindi la correlazione con i diversi livelli istituzionali coinvolti) non sarebbero state in grado di garantire i risultati attesi.

la correlazione esistente tra quell'intervento della Corte dei conti e la reazione che c'è stata successivamente da parte del Governo danneggiato ulteriormente non solo i rapporti istituzionali, ma anche la credibilità del Governo su questi temi. Ciò che vogliamo sottolineare in apertura (poi i miei colleghi interverranno successivamente) è che probabilmente il ministro Fitto, che con tutto il suo Gruppo parlamentare non ha votato il PNRR quando è nato in Europa nel 2020 e nemmeno nei passaggi successivi,

per intervenire sulla riduzione delle stesse, per intervenire sulla sanità e sulla scuola pubblica, sui servizi alla persona, per garantire il trasporto pubblico locale, per intervenire a favore del Mezzogiorno, delle aree interne, delle aree più disagiate delle aree di montagna, per garantire una transizione ecologica e una transizione digitale. Ancora oggi, noi non sappiamo se, su alcuni territori, alcuni provvedimenti e alcuni interventi sono garantiti. In maniera abbastanza generica, il ministro Fitto ci ha fatto sapere, attraverso il dibattito pubblico, che il Governo Meloni non crede nelle case di comunità; quindi, non crede alla nostra idea di sanità pubblica, basata su una rigorosa prevenzione territoriale e su una presenza della stessa sui territori. Lascerò ai miei colleghi la descrizione puntuale degli impegni che chiediamo al Governo. Nel testo 2, che abbiamo presentato alcune ore fa, abbiamo sottolineato due aspetti per noi fondamentali. Il primo è l'impegno del Governo a non utilizzare utilizzare il PNRR per armi e munizioni, un impegno che il ministro Fitto aveva già assunto in un *question time* qui al Senato, come lo stesso presidente Meloni in diverse occasioni pubbliche. e ambientale; 10) a trasmettere alle Camere, in tempo utile e comunque non oltre il 30 giugno, le schede descrittive di revisione del PNRR e del nuovo capitolo dedicato al REPowerEU, al fine di consentire alle Commissioni parlamentari competenti di presentare la relazione all'Assemblea per la conseguente deliberazione parlamentare di indirizzo; so che c'è un impegno del Governo. Gli altri punti restano per noi punti aperti e dirimenti rispetto alla possibilità di condividere la maggior parte degli impegni con un voto comune di tutta l'Assemblea. *(Applausi).* PRESIDENTE.

io illustrerò innanzitutto le ragioni per le quali, come Terzo polo, abbiamo deciso di approcciare questa discussione con una piattaforma a sé stante,

richiesto come essenziali alla buona canalizzazione e anche al cambiamento di alcune impostazioni derivanti dal passato. Il PNRR è una grande occasione per il Paese, ma è anche una grande occasione per consolidare un atteggiamento dell'Europa che, di fronte a grandi crisi, si muove compatta, agisce sulla base di un'impostazione solidaristica e lo fa con un atteggiamento in grado di valorizzare le singole peculiarità dei Paesi che utilizzano le risorse. Quindi, la sconfitta del nostro Paese sul tema del PNRR sarebbe la sconfitta non soltanto dell'Italia e della credibilità del Paese, ma anche dell'intera Europa e di quella visione solidaristica cui facevo accenno. Ed è la ragione per la quale noi non ci accoderemo mai alle file di chi spera nel tanto peggio tanto meglio e alle file di chi, magari, pensa di ricavare politicamente un qualche vantaggio dall'insuccesso del Paese. Lo dico sinceramente: in questo senso, noi siamo diversi da tutti. Siamo diversi anche dalla forza principale dell'opposizione del Governo Draghi, attualmente forza principale del Governo in carica, che, sul PNRR, ebbe un atteggiamento ben differente dal nostro. Quando c'è in gioco la credibilità del Paese, il Terzo polo fa la propria parte. Fa la propria parte con un atteggiamento magari critico, ma in grado di andare a individuare singolarmente le modalità con le quali migliorare la situazione. È questa la ragione per la quale abbiamo apprezzato la disponibilità al dialogo del ministro Fitto, che ribadisco in quest'Aula. Abbiamo apprezzato la correzione del ministro Fitto su alcune impostazioni a dir poco incredibili, come l'utilizzo delle risorse del PNRR per gli stadi, cosa che ha immediatamente corretto e reimpostato nella maniera giusta. Abbiamo anche apprezzato uno stile di dialogo,

all'interno del PNRR, magari virate verso obiettivi diversi, ma anche nel cercare di definire assieme una nuova impostazione di PNRR, nei tratti in cui il PNRR ha battuto la fiacca. Dico anche, con altrettanta franchezza, che non apprezziamo che, ogni volta che il Governo approccia al tema del PNRR, voglia marcare la differenza con il Governo precedente e magari attribuire, attraverso alibi, le responsabilità

recentemente con un voto di astensione il nuovo approccio sul PNRR e anche in questa occasione ci accingiamo a fare delle proposte di merito. Le proposte di merito che facciamo che facciamo sono due. La prima è quella di vedere un coinvolgimento attivo del Parlamento in tutte le fasi di redazione della nuova impostazione del PNRR e dei decreti conseguenti, puntualmente anche le Commissioni. Su questo siamo stati molto precisi, perché ovviamente teniamo al fatto che questa discussione sia fatta nel modo più consapevole, puntuale e coinvolgente, da parte del Parlamento. La seconda proposta è che gran parte di queste risorse vengano ridefinite e riallocate nei seguenti temi. Il primo è quello del dissesto idrogeologico e abbiamo più volte detto che, assieme a risorse nuove sul tema del dissesto, serve anche un'organizzazione nuova, che peraltro nuova non è, ma qualcosa di antico conserva, ed è quella del piano ItaliaSicura. Noi teniamo molto a un utilizzo di queste risorse per il tema dell'energia. Pensiamo che il piano Industria 4.0 abbia segnato una positività nel nostro Paese e debba essere rilanciato all'interno del nuovo PNRR. Ciò comporta un coinvolgimento maggiore di aziende di Stato, di privati e di soggetti che possono contribuire a migliorare la spesa? Se sì, ben venga, perché da parte nostra non c'è alcuna limitazione in tal senso. Anzi, pensiamo che la parte positiva del Paese debba essere tutta impegnata a cercare di garantire la cosiddetta messa a terra e la capacità di spesa di queste risorse. Termino sul tema delle armi. Al riguardo voglio dire una cosa di chiarezza in quest'Aula. Ho letto la mozione del Partito Democratico e quel punto è già stato discusso anche a livello parlamentare, quindi c'è qualcosa di già consolidato e non mi stupisce che che sia stato scritto così. Voglio però sottolineare una certa ipocrisia in quel punto, che oggi magari non sarà la partita divisiva tra noi perché, quando una decisione è già stata presa, è inutile incaponirsi. Di recente il senatore Spagnolli è stato in visita all'arsenale militare di La Spezia e magari continueranno le visite della sua Commissione in quello di Taranto e in altre realtà. Quando si fa un investimento in un arsenale militare o in un'azienda che ha una produzione armiera o che produce macchinari di grande capacità innovativa sul piano della difesa

per la tenuta e il mantenimento della democrazia in Europa. Quindi, fare una distinzione sull'utilizzo in Ucraina o meno è pura ipocrisia utilizzata sul piano politico per marcare una differenza, quando questa differenza - ripeto - è del tutto sbagliata e del tutto irrilevante. Lo diciamo per amor di verità e lo dico perché qua dentro - a mio modo di vedere - le battaglie in qualche modo ambigue non dovrebbero essere combattute. Lo dico perché da quello che capisco questa opinione accomuna la destra di Governo e la sinistra. Ecco, fatemi dire che scrivere una cosa del genere è davvero del tutto irrilevante e del tutto ambiguo rispetto agli obiettivi che noi ci diamo anche di lotta contro le autocrazie.

del Governo, qual è lo stato dell'arte. Una cosa è certa: molti degli obiettivi che ci si era posti non siamo oggi in grado di onorarli. In sostanza, basti pensare che la Corte dei conti dice - quindi non io, non noi noi - che nei primi cinque mesi del 2023 è stato speso un miliardo, portando la spesa complessiva a 25,7 miliardi di euro, appena il 13 per cento dei fondi previsti da qui al 2026.

il senatore Boccia nella sua illustrazione - noi abbiamo avuto risorse maggiori degli altri per affrontare i problemi della disuguaglianza tra Nord e Sud del Paese dentro le stesse realtà, ovviamente su alcuni temi importanti,

porta nella situazione in cui le disuguaglianze aumentano e i costi aumentano, anche da un punto di vista economico. Questo è il dato su cui il Governo ci deve dire problema che noi denunciamo - vorrei ricordare che lo facciamo anche nel Documento economico finanziario - è il seguente: quando avete modificato la *governance*, avete portato tutto al centro, escludendo il coinvolgimento di Comuni e Regioni. Posso testimoniare che nella mia realtà, nella Brianza in cui vivo, certamente chi sta spendendo le risorse sul PNRR sono i Comuni. Ad esempio, nel mio piccolo Comune si sta rifacendo

se ci sono delle correzioni da apportare. C'è chi dice che bisogna rinunciare a un pezzo di risorse, c'è chi dice che bisogna spostarle, ma qual è la ragione? Perché? Se non si ha il quadro preciso, non si può ragionare. Infine,

se oggi siamo qui a discutere ancora una volta di PNRR è perché continuiamo ad assistere a comportamenti schizofrenici, che impongono dovute riflessioni. «Non disturbare chi vuole fare» è il motto di questo Governo, annunciato dalla Meloni e, dopo otto mesi, siamo ancora a chiederci: «Ma a fare cosa?». Registriamo non solo le continue uscite dei Ministri, che mettono quotidianamente in dubbio la riuscita della spesa dei fondi del PNRR. Accertiamo che ad oggi l'unica certezza è la vostra incapacità.

dei servizi al cittadino. Ho parlato di comportamenti schizofrenici, come il tentativo di imbavagliare la Corte dei conti sull'attuazione del PNRR: l'ennesimo tentativo di trovare un capro espiatorio per mascherare il fallimento nella gestione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questo solo basta a preoccuparci e dovrebbe preoccupare tutti, poiché non esiste ad oggi alcun atto, alcun documento e alcune analisi che attesti che il controllo concomitante rallenti l'attuazione dei progetti del PNRR. Eppure, si vuole limitare il controllo della Corte dei conti e questo è molto pericoloso, colleghi, perché certifica il non riconoscimento da parte del Governo del ruolo fondamentale delle autorità di controllo indipendenti, il non riconoscimento dell'equilibrio tra controllori e controllati, tra sistemi di gestione e sistemi di controllo, la cui assenza svuota di significato la parola democrazia. D'altronde, però, cosa aspettarsi da chi dichiara che le tasse sono un pizzo di Stato o che è onesto chi non paga le tasse? Nei novi punti della mozione chiediamo serietà di approccio, chiarezza istituzionale e trasparenza: caratteristiche richieste anche a livello europeo. Già, perché la Corte dei conti - questa volta però quella europea - ha rivolto alla Commissione europea nei giorni scorsi cinque raccomandazioni, tutte accolte senza riserve e alcune di queste riguardano proprio l'Italia. In cima ai rischi ci sono il mancato rispetto dei tempi e la mancata messa in opera delle riforme necessarie, secondo le scadenze previste e concordate. Viene considerato anche il nuovo codice degli appalti,

riducendo la concorrenza e sollevando dubbi sulla trasparenza, due pilastri delle migliori pratiche internazionali, signor Presidente. Ecco però il ministro Giorgetti esternare alla festa de «Il Messaggero» che quelli europei sono dei tecnici burocrati cavillosi. invece di perdere tempo per evitare i controlli, non sarebbe meglio impiegare questo tempo per capire come spendere i 209 miliardi che vi siete casualmente ritrovati a gestire? Del resto, vi sarà difficile mettere alla Corte dei conti europea lo stesso bagaglio che avete messo alla Corte dei conti italiana. Presidente, abbiamo assistito a uno sforzo di questo governo nell'eliminazione dei più gravi reati di corruzione dal novero dei reati ostativi, dall'abuso d'ufficio al taglio delle intercettazioni telefoniche; uno sforzo notevole, come a dimostrare che il concetto di spesa dipende dall'indebolimento degli anticorpi dello Stato contro la criminalità. Lo diciamo con chiarezza, signor Presidente, con le parole del collega Silvestri non vi lasceremo trasformare il sogno del PNRR a servizio degli italiani in un incubo, quella che per il nostro Paese doveva essere un'alba in un definitivo tramonto. *(Applausi)*. Signor Presidente, con il Piano di ripresa e resilienza, che ha l'obiettivo di sostenere i Paesi dell'Unione europea e a ripartire dopo gli enormi danni economici, ma anche sociali, causati dall'emergenza sanitaria da coronavirus, si vuole contribuire anche a rendere le economie dei Paesi più eque e sostenibili, resilienti, preparate alle grandi sfide che stiamo affrontando e alle opportunità della transizione ecologica che noi sosteniamo, ovviamente equa e giusta, e a quella ovviamente digitale. Si è trattato di fatto del primo importante segnale, da parte delle istituzioni europee, di effettiva solidarietà nel contesto dell'Unione dell'Unione europea, che finalmente si occupa non solo di norme, direttive e regolamenti vincolanti e spesso lontani dalle priorità dei cittadini, ma anche di risorse da usare in prospettiva come investimenti intelligenti e strategici in settori che non possono più essere sottovalutati. La crisi sanitaria e il mutato scenario geopolitico in seguito alla guerra in Ucraina sono stati un risveglio molto, molto duro per Bruxelles. Ci si è accorti che parte delle industrie strategiche avevano una produzione fuori dai confini europei; che filiere di approvvigionamento energetico dipendevano da alcuni Stati ostili e che, a causa di una miope visione, negli anni precedenti si era preferita una rigidità di regole ferree a una flessibilità che avrebbe stimolato la crescita e agevolato gli imprenditori a rimanere all'interno dei confini dell'Unione. Si tratta di errori che, pian piano, si incominciano a riconoscere e che noi della Lega da anni denunciamo, nel silenzio di chi all'epoca aveva paura di difendere l'interesse nazionale, delle nostre imprese e dei nostri imprenditori. Ora alcune cose stanno migliorando, certamente, ma molta strada deve essere ancora fatta. Sicuramente il capitolo REPowerEU tocca un settore strategico come quello energetico e mostra due vie maestre sulle quali è necessario investire: sicurezza e indipendenza energetica, due carte fondamentali sia per la questione economica che per quella geopolitica. Ora, dopo essersi resi conto che non potevamo essere dipendenti dal gas russo, è necessario fare tutto il possibile per evitare di passare da una dipendenza ad un'altra, ed è necessario indirizzare gli investimenti per sottrarsi a quella dipendenza dalle tecnologie cinesi che rischia di minare il nostro futuro e legarci inevitabilmente mani e piedi a Pechino. Grazie a questo Governo, che senza paura e senza soggezione alcuna sta facendo emergere questi argomenti e vuol rilanciare la competitività dell'Italia nel contesto europeo e globale attraverso progetti seri e credibili di infrastrutture, sanità, ambiente e tecnologie, ma anche istruzione e ricerca, il nostro Paese sta dimostrando serietà e autorevolezza. Il ruolo protagonista dell'Italia nel contesto europeo è innegabile da parte e di tutte le parti in causa. Inoltre, molto è stato fatto per rispettare gli impegni, le scadenze e il perimetro entro il quale il nostro Paese intende operare e negoziare con l'Unione europea. Voglio inoltre ricordare che la modifica della *governance* non ha assolutamente portato alcun rallentamento o interruzione della fase di esecuzione del Piano, ma anzi ha dato continuità e rafforzato l'operatività. Per questi motivi, chiediamo al Governo di continuare nell'attuazione delle riforme e degli investimenti previsti con il PNRR, come aggiornato anche con l'inserimento del REPowerEU, e ad elaborare una proposta di aggiornamento del Piano stesso che si focalizzi specificamente su misure che hanno registrato un notevole ritardo nella fase di avvio o un rilevante incremento dei costi, evidentemente a causa dell'inflazione, della mancanza di materie prime, ovvero di altre circostanze oggettive e non preventivabili. Concludo, signor Presidente, ricordando un breve aneddoto. Nel mio mandato precedente come europarlamentare ho partecipato a diversi incontri e riunioni, e c'era anche il ministro Fitto, sempre estremamente operativo e competente. Assieme ai colleghi abbiamo discusso di PNRR, ma poche volte, se non forse nessuna, ho sentito deputati europei di altre Nazioni parlare male del proprio Paese o cercare di mettere i bastoni tra le ruote al proprio Governo. Anche se all'opposizione, quando si parlava di questioni strategiche e di interesse nazionale, tutti erano presenti. Vivendo un momento particolarmente sensibile da un punto di vista sia economico che sociale, auspico davvero che tale maturità possa venire anche dalle nostre opposizioni. L'interesse nazionale va difeso sempre e non solo quando si è al Governo. Questa è la maniera di fare quel sistema Paese di cui tanti si riempiono la bocca, ma di cui poi, per meri calcoli di politica interna, qualcuno dei banchi dell'opposizione si dimentica immediatamente.

la modernizzano, garantendo in questo modo un futuro migliore per tutti gli italiani. Si tratta di un'occasione senza precedenti, che ci potrebbe consentire di affrontare le grandi sfide del nuovo secolo, a cominciare dai cambiamenti climatici e dall'abuso del suolo, riducendo le diseguaglianze sempre più profonde nel nostro Paese. Ecco perché sulla piena attuazione del PNRR (oltre 191 miliardi di euro) l'Italia si gioca la sua credibilità e la sua affidabilità internazionale. E ripeto credibilità e affidabilità. Fallire la realizzazione del PNRR equivarrebbe a dare una testimonianza di inefficienza e inaffidabilità dell'Italia nel contesto internazionale. Riteniamo davvero molto preoccupanti le parole del Governo delle ultime settimane, che prefigurano come l'Italia potrebbe anche rinunciare al conseguimento conseguimento di una parte degli obiettivi previsti dal Piano; una visione sbagliata, che il Partito Democratico contesta alla radice. Non si può oggi alzare le mani per incapacità o, peggio, perché si ritiene che poi a tutta questa modernizzazione possiamo anche rinunciare, che - tale visione è sostenuta anche dal ministro Fitto - queste riforme avrebbero ricadute negative per l'Italia, qualora dovessimo rivedere il Patto di stabilità. Se così fosse, rappresentanti del Governo, avreste già clamorosamente fallito la vostra missione. Quindi, prendete atto della vostra clamorosa incapacità. Non può l'Italia, non potete voi della maggioranza avere incertezze, perplessità o tentennamenti davanti a questa straordinaria occasione. Le vostre incertezze e le vostre indecisioni possono rivelarsi fatali e già stanno compromettendo il raggiungimento di diversi obiettivi. Sarebbe imperdonabile indietreggiare. Invece tutti gli ultimi atti e pronunciamenti di questo Esecutivo ci fanno tremendamente preoccupare. Dovete dirlo e dirlo ora se non condividete gli obiettivi del Next generation EU. Chiediamo trasparenza e sincerità. Abbiamo sotto gli occhi l'esempio del MES: per la vostra chiusura ideologica, l'Italia sta accumulando un ritardo sempre più ingiustificabile di fronte a tutti gli altri Paesi, unica tra i venti dell'eurozona che ancora non ha ratificato la riforma del regolamento. Il *premier* Meloni pronuncia la parola «stigma» come una formula magica e intanto l'Italia è isolata. Gli investimenti nelle infrastrutture procedono a rilento e lo stesso succede ai piani per le rinnovabili e il lavoro, per non parlare di quelli legati al trasporto pubblico locale, alla scuola, all'università e alla sanità. Per noi migliorare la sanità pubblica è un obiettivo prioritario irrinunciabile, perché noi siamo dalla parte dei cittadini, di tutti i cittadini. Sento parlare meno di come queste risorse dovranno trasformarsi in opportunità concrete per il Paese di rilancio economico e soprattutto di cambio di passo sull'inclusione sociale e sulla sostenibilità. Come non affrontare il tema dell'occupazione femminile. Come non sottolineare che stiamo rischiando di spaccare il Paese perché vi state dimenticando del Mezzogiorno? Ecco perché siamo preoccupati. Davanti a tutto questo ci si aspetterebbe dal Governo un impegno eccezionale e straordinario, quasi dovesse diventare - e giustamente - una ossessione quotidiana su cui coinvolgere pienamente tutte le parti sociali, i territori, le categorie economiche, i sindacati, il terzo settore, le università, i centri di ricerca. Di tutto questo abbiamo perso le tracce. Non vediamo impegnate le energie che questa impresa impresa necessita e risulta davvero incomprensibile questa resa. Ma come: avete già annunciato che alcuni obiettivi non saranno realizzati? Qualcuno dice anche apertamente di restituire delle risorse, per poi magari - come già è stato fatto in altre occasioni - scaricare la colpa su altri se non si centra

tutte le risorse che l'Europa ci ha messo a disposizione, tirate le conclusioni e ammettetelo, senza incolpare altri al posto vostro. Ma c'è una cosa che sarebbe ancora più grave dell'incapacità, e cioè il fatto che non volete utilizzare le risorse del PNRR perché siete contrari al modello di sviluppo che quel Piano indica. Siete Siete ancora per il motore a scoppio e per le fonti energetiche fossili. Negate i cambiamenti climatici. Non volete i progetti di transizione economica. È un oscurantismo anacronistico che combatteremo sempre, egregio collega Dreosto. Vi chiediamo una cosa sola, non fare perdere all'Italia questa straordinaria opportunità, questa occasione di ripresa e di riscatto, che può rappresentare e già rappresenta la più eccezionale occasione per modernizzare l'Italia e ridurre le disuguaglianze tra territori e

rappresentante del Governo, il Governo Meloni è entrato in carica il 23 ottobre scorso. A quella data erano stati raggiunti appena 25 dei 55 obiettivi stabiliti per il secondo semestre, cioè meno della metà. entro il 31 dicembre, questo Governo ha conseguito i restanti trenta traguardi. Successivamente è stata inoltrata alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza *tranche* del valore di 19 miliardi. A differenza degli altri Stati membri, l'Italia ha puntualmente presentato le richieste di pagamento entro i termini stabiliti. Il nostro Paese è stato uno dei pochissimi, su un totale di 27, ad aver inviato alla Commissione europea ben tre richieste di pagamento e questo nonostante il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano presenti un numero significativamente maggiore di scadenze totali e la percentuale più alta di indicatori relativi ai risultati utilizzati per valutare il raggiungimento degli obiettivi. Desidero precisare che ad ottobre scorso si è cercato di diffondere una narrazione distorta riguardante il ritardo dell'Italia nell'attuazione del PNRR. In particolare, si è tentato di attribuire ritardi al nostro Governo, mentre la realtà dei fatti dimostra chiaramente la sua abilità nel gestire e adempiere agli impegni assunti. Nel frattempo il nostro Governo è attivamente impegnato nella rimodulazione degli obiettivi del PNRR, la cui prima stesura risale a quando l'Europa era impegnata nella gestione della pandemia da Covid-19 alla luce dei cambiamenti nella geopolitica globale conseguente l'invasione della Russia in Ucraina. In tal senso il capitolo aggiuntivo riguardante il REPowerEU mira a coordinare e allineare i quadri programmatici delle diverse fonti di finanziamento sia europei che nazionali, al fine di garantire una gestione più efficace ed efficiente. Questo permetterà di affrontare, in maniera mirata e con soluzioni adeguate, le sfide legate all'aumento dei costi energetici e alla necessità di costruire passo dopo passo una maggiore indipendenza nazionale dalle fonti energetiche straniere, fornendo un supporto concreto alle imprese e alle famiglie in difficoltà. La quota italiana dei fondi REPowerEU ammonta a 2,7 miliardi di euro, a cui si può aggiungere fino al 7,5 per cento dei fondi della politica di coesione relativi alla programmazione 2021-2027. Pertanto, è fondamentale che il capitolo REPowerEU del PNRR italiano includa riforme e investimenti realizzabili entro il periodo del dispositivo di ripresa e resilienza, contribuendo concretamente al raggiungimento degli obiettivi di diversificazione dell'approvvigionamento energetico, riduzione dei combustibili fossili e aumento della resilienza, sicurezza e sostenibilità del sistema energetico italiano. Nonostante qualcuno stia alimentando una narrazione fuorviante, l'Italia non è in ritardo nella riprogrammazione dei fondi europei e della coesione. Secondo il Regolamento europeo il termine per definire la riprogrammazione è il 31 agosto; ciò significa che mancano ancora più di due mesi. Solo 8 Stati membri hanno già presentato le modifiche con l'inserimento del nuovo capitolo del REPowerEU all'interno del PNRR. pertanto dimostra coerentemente di essere in linea con le modalità e i tempi del dibattito in corso. Il Governo ha avviato interazioni costanti con la Commissione europea riguardo all'aggiornamento del PNRR e al capitolo REPowerEU. Lo scopo di tali interazioni è proprio quello di concordare preventivamente i contenuti, i tempi e le modalità di presentazione della riprogrammazione entro il termine del 31 agosto 2023, previsto dai regolamenti europei. Nella cabina di regia del PNRR del 31 maggio scorso è stata poi approvata la terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR. La relazione, trasmessa al Parlamento il 7 giugno 2023, ha tutti i contenuti preliminari del Capitolo REPowerEU del PNRR italiano. Sono descritte le macrotipologie formulate formulate dalle amministrazioni per la modifica del PNRR, tra cui la rimodulazione delle *milestone* e dei *target* a causa dell'aumento dei prezzi o di altri fattori oggettivi; la rimodulazione delle scadenze delle *milestone* e dei *target* intermedi senza che vengano modificate le *milestone* e i *target* finali; la previsione dei meccanismi di verifica per chiarire gli obiettivi e le revisioni connesse alle criticità nel contesto attuativo e la riallocazione delle risorse per l'utilizzo più efficiente. La mozione di oggi ha l'intenzione in quest'Aula di impegnare il Governo a continuare nell'implementazione delle riforme e degli investimenti previsti dal PNRR, incluso il capitolo REPowerEU, adottando tutte le misure necessarie per garantire il raggiungimento tempestivo delle *milestone* e dei *target* entro il 2026, mantenendo il Parlamento informato sullo stato di attuazione del PNRR, sugli investimenti e sulle riforme incluse nella propria proposta di aggiornamento. Si chiede poi il coinvolgimento attivo delle principali società a partecipazione pubblica statale, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e degli enti locali per riformulare insieme l'aggiornamento del PNRR nel capitolo REPowerEU italiano. Si richiede inoltre di includere nel capitolo REPowerEU del PNRR italiano proposte di investimento e riforme coerenti con gli obiettivi e le condizioni stabilite a livello europeo. Queste proposte dovrebbero riguardare principalmente la modernizzazione delle reti di trasmissione e distribuzione di energia, la promozione delle energie rinnovabili e la riduzione della domanda energetica e la sua transizione verso fonti rinnovabili. Al fine di garantire il completo successo del PNRR e il raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti, chiediamo al Governo di elaborare una proposta di aggiornamento al Piano focalizzata innanzitutto sulle misure che hanno subito ritardi significativi nella fase di avvio e hanno registrato un aumento dei costi a causa di fattori come l'inflazione, la mancanza di materie prime o altre circostanze oggettive e imprevedibili. Parliamo di interventi che, qualora esclusi dal PNRR, dovranno essere protetti attraverso altre fonti di finanziamento nazionali o mediante un utilizzo diverso delle risorse provenienti dalla programmazione 2021-2027. L'aggiornamento del PNRR e del capitolo REPowerEU italiano dovranno determinare un miglioramento tangibile e duraturo per l'Italia. e attenzione con le quali sta affrontando questa tematica così importante e strategica per l'Italia. Caro Ministro, Fratelli d'Italia e tutta la maggioranza sono compatte e coese con lei. Continui su questa strada e ci vedrà sempre al suo fianco.

portare un contributo di chiarezza su alcuni aspetti che evidentemente vengono rappresentati in modo difforme da quella che è la realtà dei fatti. Io ho il dovere di iniziare in questo modo perché ho ascoltato con molta attenzione gli interventi di tutti coloro i quali hanno portato il loro contributo e devo dire che su alcune questioni ci sono dei dati che oggettivamente non corrispondono alla realtà dei fatti. Io, più che una replica di carattere generico su molte critiche altrettanto generiche che ho ascoltato, cercherò di riportare la discussione in modo specifico sulle singole questioni per poter dare una risposta diretta anche rispetto alle critiche che vengono avanzate. Diversamente, rischiamo di sollevare una discussione che ci allontana dal merito delle questioni. E penso che su un argomento così rilevante ed importante sia indispensabile parlare del merito delle singole questioni sollevate sia nella mozione, sia nel dibattito parlamentare. Ho seguito con molta attenzione gli interventi dei senatori che hanno portato il loro contributo e devo partire da alcune valutazioni di carattere generale. Le discussioni e i ritardi che vengono indicati e che accompagnano ogni intervento dovrebbero essere dettagliati, nel senso che sarebbe opportuno indicare in modo specifico la ragione e la responsabilità del ritardo, quando quest'ultimo è stato effettuato, con quali motivazioni e quale proposta si porta per modificarlo. Procedendo

nella ricostruzione dei fatti si tenti di attribuire queste responsabilità all'attuale Governo: è un paradosso che sinceramente non possiamo in alcun modo accettare. *(Applausi)*. Dettaglierò le questioni. Il Governo si è insediato alla fine di ottobre 2022; gli obiettivi da raggiungere per poter ottenere la terza rata erano 55. Abbiamo trovato - è un fatto ufficiale - 25 obiettivi raggiunti a quella data, abbiamo predisposto tutti gli atti collegati per il raggiungimento degli altri 30 obiettivi mancanti per arrivare a 55 obiettivi.

tradizionalmente una fase abbastanza lunga e complessa con tutti gli Stati membri, non con l'Italia. È così complessa perché per la prima volta il nostro Paese si trovava con la terza rata non solamente ad avere il maggior numero di obiettivi (55), ma anche una valutazione di merito sulle *milestone* e che interveniva sugli obiettivi fisici, nel senso che per la prima volta si passava dall'approvazione di documenti e norme alla verifica dell'inizio della spesa delle risorse. Vi era quindi una fisicità degli interventi diretti che andava verificata. Abbiamo aperto questa fase di verifica, che è in via di conclusione, nella quale abbiamo recepito molte indicazioni. Non voglio aprire il tema del perché, del come e di quali atti abbiamo modificato; andiamo recepito molti suggerimenti che hanno cambiato profondamente alcune scelte e che sono anche oggetto di un'analisi all'interno della relazione semestrale che è stata già depositata in Parlamento e che sarà oggetto del confronto che avremo nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.

la relazione della Corte evidenzia le incapacità di questo Governo. Questo è ciò che noi ascoltiamo. Ebbene, la relazione della Corte dei conti

distruttive importanti, ma che in due mesi abbiamo creato le condizioni per tutto lo scatafascio che viene rappresentato sinceramente lo trovo abbastanza imbarazzante dal punto di vista della critica. a questo vorrei evidenziare un approccio differente che io mi auguro ci possa essere sul tema del PNRR. Penso infatti che l'approccio aggressivo, critico a prescindere, con l'idea di individuare le responsabilità per forza in capo a questo Governo

penso che sia importante dire le cose come stanno, ma non con critiche generiche dicendo che abbiamo tolto il controllo alla Corte dei conti perché viviamo nella illegittimità e quindi vogliamo fare chissà che cosa. Rimettiamo in ordine le situazioni: il controllo della Corte dei conti rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza è previsto nel decreto-legge n. 77 del 2021 che è previsto come *milestone* all'interno del programma con la Commissione europea. Quel decreto-legge è stato votato da tutti i partiti che sostenevano il Governo Draghi ed è stato sostenuto perché regola il controllo conseguente, non il controllo consultivo preventivo concomitante, così come è stato indicato successivamente. Basta leggere la delibera.

ma non prevede il richiamo alla legge prevista specificatamente per il controllo sul PNRR. Prova ne sia che la Commissione europea, rispetto a quello che noi abbiamo determinato come motivo di modifica rispetto al controllo della Corte dei conti, non ha potuto sollevare nulla, ma ha condiviso, per il semplice fatto che noi siamo

erariale, che è stata approvata dal Governo Conte 2, prorogata una prima volta dal Governo Conte 2 e prorogata dal Governo Draghi. Quando, però, la proroghiamo noi, si crea un dibattito che, sinceramente, è abbastanza singolare. Io ritengo che su questi temi, andando nel dettaglio di merito dei provvedimenti, vi sia bisogno di affrontare le questioni in modo chiaro. Diversamente, costruiamo una narrazione che non corrisponde alla realtà dei fatti. Vengo al tema della quarta rata, che prevede ventisette obiettivi al 30 giugno di quest'anno; obiettivi sui quali, evidentemente, c'è la necessità di intervenire per correggerne e modificarne alcuni. Qui voglio fare due esempi concreti. Il primo è quello relativo alle colonnine dell'idrogeno all'interno

la domanda è: c'è un tema che riguarda una incapacità di questo Governo, che nulla c'entra rispetto a tutto questo percorso? O vi è l'esigenza di adeguare e modificare il *target* di riferimento, perché evidentemente esso non può essere raggiunto, per dati oggettivi? quando parliamo del tema degli asili, evidentemente, nella costruzione del percorso dei bandi, dal punto di vista dei tempi e del merito una serie di difficoltà, che verificheremo nel dettaglio, perché porteremo all'esame anche il dettaglio di quello che sto per dire. Quando noi lavoriamo con la Commissione europea per modificare questo obiettivo intermedio, lo facciamo per quale ragione? Perché vogliamo, come viene detto, cancellare gli asili nido? O perché vogliamo correggere un *target* intermedio per raggiungere l'obiettivo finale, realizzando gli asili, che sono l'obiettivo finale, visto che l'obiettivo intermedio non lo si può raggiungere per un dato di fatto oggettivo?

è stato fatto un lavoro dettagliato per ridefinire la *governance* del PNRR e della coesione. Dirò qualcosa di più preciso anche su questo tema, che prevede, dal punto di vista delle scelte, una organizzazione che rafforza, da una parte, la struttura di missione in capo a Palazzo Chigi e, dall'altra, l'ispettorato in capo al Ministero dell'economia e delle finanze e della Ragioneria generale dello Stato, perché questi sono due strumenti fondamentali che devono interagire. La validità e la credibilità di questo decreto sta nel fatto che, come ho detto già in altre circostanze, contro i Comuni e nessuna posizione contraria al sistema di autonomie locali. Fino a prova contraria, infatti, questo decreto-legge è stato approvato in Conferenza unificata, col parere favorevole dei Comuni, delle Regioni e delle Province. Sono fatti, non sono opinioni. Sono fatti, che io voglio riportare alla vostra attenzione per provare a riportare il dibattito sul giusto canale, sul giusto binario, perché noi abbiamo bisogno, in questo momento, di avere un approccio un approccio su questo tema che sia coerente. Il senatore Magni ci invitava a fare attenzione, perché le strutture di missione presso i Ministeri si stanno indebolendo, dal momento che il personale non è stabilizzato. Ma nel nostro decreto-legge abbiamo stabilizzato quel personale che non era stabilizzato prima. Lo abbiamo fatto noi, basta leggere il decreto-legge, per trovare una risposta in quella direzione. Quindi sono tutti elementi che testimoniano in modo concreto il lavoro che si sta portando avanti e anche il fatto che, rispetto a questo lavoro, non possiamo immaginare che ci sia un tentativo di narrazione negativa a prescindere, quando un un elemento di comparazione con il resto d'Europa ci aiuta a comprendere la situazione. Vogliamo parlare dei presunti ritardi della terza rata? Quanti Paesi in Europa hanno chiesto la terza rata? Sono

Questo è il quadro della comparazione, nel contesto europeo, sulla terza rata. Allo stesso modo, rispetto al tema della richiesta della modifica del piano, integrato con il regolamento REPowerEU, vorrei ricordare, per amor di verità, quando qualcuno ha parlato nel Paese, dopo l'invasione dell'Ucraina, molti mesi prima che ci fosse l'attuale Governo, della necessità di modificare il piano in funzione delle nuove esigenze, allora non lo si poteva dire. Non lo si poteva dire, perché il piano non si poteva modificare. Oggi tutti discutiamo, per fortuna, dell'adeguamento del piano sulla base di quello che ha deciso la Commissione europea, con l'approvazione del regolamento REPowerEU, che prevede una serie di interventi in questa direzione, che però ci portano anche qui, se vogliamo fare una comparazione, ad avere solo paesi che hanno già presentato il piano modificato con il REPowerEU e due Paesi che hanno presentato delle singole modifiche senza il REPowerEU. Il termine è il 31 agosto. Se è vero, come è vero, che abbiamo il piano più importante nel contesto europeo, è anche vero che è un po' più complesso rimodellare e riorganizzare questo piano, rispetto a quanto si faccia in altri Paesi, visto che stiamo parlando di una cifra molto rilevante. per un chiarimento, perché spesso, anche alla Camera dei deputati, viene ribadito che avete lasciato in eredità un piano così importante, grazie al lavoro fatto, e noi non siamo capaci di spenderlo. Questo è un po' il messaggio che si prova a dare. Vediamo però quali sono i criteri in base ai quali abbiamo ottenuto queste risorse.

*(Applausi)*: la dimensione della popolazione, la mancata crescita del PIL durante la fase Covid e la mancata crescita dell'occupazione. Essendo questi dati tra i più negativi in assoluto - i nostri dati erano tra i peggiori, in quella circostanza - abbiamo avuto un parametro che ci ha consegnato 68 68 miliardi di euro a fondo perduto. Poi, dopo, c'è stata la scelta di prendere per intero, come la Grecia e la Romania, la quota a debito, per arrivare ai 122 miliardi di euro a debito, più i 30 miliardi di euro di Fondo complementare nazionale. Questo è il quadro nel quale ci stiamo muovendo e in questo quadro sinceramente

per evidenziare negativamente il lavoro del Governo, invece è proprio il contrario, perché se leggiamo le raccomandazioni della Commissione europea, al netto di qualche titolo, ma leggendole una per una - non solo quella dell'Italia, ma anche quelle degli altri Paesi - vediamo c'è una prima raccomandazione che parla della necessità di andare velocemente e di fare rapidamente nell'azione di modifica e spesa del piano, che troviamo nelle raccomandazioni rivolte a tutti i Paesi. Addirittura in alcuni Paesi, anche impensabili, la troviamo rafforzata e ancora più critica rispetto a questo tema. Poi troviamo una seconda raccomandazione, che è quella del rafforzamento della capacità amministrativa, soprattutto nei confronti dei Comuni e degli enti territoriali, cosa che nel decreto-legge n. 13 abbiamo iniziato a fare e nel decreto-legge sulla pubblica amministrazione abbiamo confermato e stiamo portando avanti ulteriormente: è un dato oggettivo. La terza questione che viene indicata è una questione della quale questo Governo fa un punto - se mi consentite - anche di orgoglio, perché è stata una scelta lungimirante del presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quando al momento dell'insediamento di questo Governo, nell'organizzazione delle deleghe, ha messo insieme il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le risorse della coesione, che è la terza raccomandazione che qualche settimana fa la Commissione europea ha fatto agli Stati membri, quella cioè di raccordare l'utilizzo di queste risorse. Noi lo abbiamo immaginato all'inizio della legislatura, lo abbiamo inserito nelle deleghe del Governo e lo stiamo praticando in un lavoro coerente con ogni singola Regione rispetto all'utilizzo delle risorse della Anche qui, c'è grande polemica, ma la polemica secondo me viene spazzata via dai numeri e dai fatti. Viene spazzata via, per esempio, dai dati Istat dei giorni scorsi, che ci raccontano di quanto sia stata inefficace la spesa delle risorse europee della coesione dal punto di vista della capacità capacità di incidere positivamente sui meccanismi e sui numeri economici del Mezzogiorno d'Italia e dell'Italia. Sono fatti, non dati che noi portiamo come opinione. Su questo è altrettanto importante immaginare che l'azione coordinata delle risorse della coesione con il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha un doppio obiettivo strategico: il primo è evitare che ci siano due programmazioni, una molto grande, ma l'altra altrettanto grande, perché la coesione 2021-2027 complessivamente ha oltre 40 miliardi di risorse europee, più la quota di cofinanziamento nazionale, più il fondo di sviluppo e coesione (quindi cifre rilevanti ed importanti), che operano sullo stesso Paese, sullo stesso territorio, in contraddizione con quanto previsto dal PNRR. Questo era il rischio e l'aver voluto, invece, una visione unica e d'insieme di questa programmazione ci consente di guardare con chiarezza anche a delle scelte strategiche. Soprattutto, la seconda riflessione positiva è che ci consente di utilizzare, nella valutazione specifica dell'attuazione del PNRR, anche quei progetti che sono critici. Sì, critici. Ogni volta solleviamo un problema: siamo a giugno del 2023 giugno 2026 è fra tre anni. Dobbiamo portare una dose di realismo nel nostro dibattito: la coesione ha una scadenza al 31 dicembre del 2029 e può essere l'occasione per coordinare la differenza dei finanziamenti all'interno del rapporto fra i due programmi. Questa cosa va detta con molta chiarezza, soprattutto rispetto ad un'altra questione. La critica è: voi pensate di utilizzare i soldi della coesione per finanziare dei progetti già esistenti. prendiamo i numeri della coesione 2014-2020; il Governo ha predisposto un monitoraggio attento su questo, una relazione che è stata oggetto di approvazione in Consiglio dei ministri e di discussione nelle Commissioni parlamentari congiunte. Sulla spesa 2014-2020, su 126 miliardi di euro, dopo nove anni, la percentuale di spesa è del 34 per cento: questo non lo diciamo noi, lo dicono i dati della Ragioneria generale dello Stato. Qualcuno magari li potrà criticare, ma deve darmi un riferimento più credibile dei dati della Ragioneria generale dello Stato o della relazione sulla coesione della Corte dei conti, visto che viene richiamato spesso questo organo, o dell'ottava relazione sulla coesione della Commissione europea. Possiamo richiamare degli elementi oggettivi che ci spiegano quanto sia complesso il tema dell'utilizzo di queste risorse e quanto sia fondamentale non solamente avere insieme la politica del PNRR e quella della coesione, perché non c'è solamente un tema della quantità della spesa, che resta il tema principale, ma c'è anche un tema della qualità della spesa, che deve essere efficace e introdurre meccanismi virtuosi e positivi rispetto alle questioni di fronte alle quali ci troviamo. Questo è il quadro di fronte al quale ci stiamo muovendo ed è per questo che riteniamo che, a partire - come veramente auspico - dalla discussione che avremo sulla relazione semestrale nei prossimi giorni, ci possa essere un dibattito propositivo che non sia quello di chi immagina di scagliarsi contro presunte responsabilità che non vengono mai circostanziate, ma che si basi invece su un confronto vero che porti alla modifica del PNRR, con il REPowerEU, che sicuramente è uno strumento fondamentale per dare una risposta alla crisi energetica del nostro Paese; non solo, sulla base delle indicazioni della Commissione europea, anche alla possibilità di utilizzare, all'interno della riverifica e del monitoraggio del PNRR, il cambio di alcuni interventi che non dovessero riuscire ad essere spesi entro il giugno del 2026. Questo lavoro giungerà in Parlamento, visto che la mozione lo rivendica, quando gli elementi sui quali stiamo lavorando saranno dettagliati, e giungerà nei tempi previsti che rispettano la tempistica indicata dai regolamenti europei. Avremo poi un dibattito parlamentare. Io sono venuto in Parlamento diverse volte e ci ritornerò con piacere ogni volta che verrà chiesto. Devo dire che

per allargare la partecipazione decisionale in quel contesto; lo abbiamo fatto e lo vogliamo fare anche in momenti di confronto parlamentare come questo. Per questo, nell'ambito di questo dibattito, posso esprimere

in sede parlamentare e come abbiamo ribadito in più circostanze, se può essere utile a chiudere una discussione sulla possibilità che il Governo Meloni abbia preso in considerazione

che sui passaggi successivi, che non mancheranno anche nell'immediatezza, ci possa essere l'occasione per entrare nel merito delle questioni e, soprattutto, per poter discutere realmente di un percorso che non sarà breve.

per la modifica di alcuni obiettivi, che non sono solo quelli della quarta rata, ma che saranno quelli di tutte le scadenze che ci accompagneranno al giugno del 2026 e la rimodulazione ha l'obiettivo di dare una risposta organica in questa direzione, cogliendo le opportunità che vengono date dalle stesse decisioni assunte a livello europeo: penso, per esempio, al Consiglio europeo dello scorso febbraio, quando è stata data un'indicazione molto chiara sulla flessibilità flessibilità dei programmi di intervento. Questa è stata una proposta del Presidente del Consiglio italiano, condivisa da tutti i Primi Ministri in quel consesso e questo è un aspetto molto importante. Al tempo stesso, penso che sia altrettanto rilevante e utile cercare di costruire, nell'ambito del percorso che ci accompagnerà alla fase di realizzazione, delle scelte che siano coerenti anche con il cambio di scenario che abbiamo di fronte. Infatti i fattori dinanzi ai quali ci siamo trovati non sono di di poco conto. Ritengo che, quando fu scritto il famoso articolo 21, che prevedeva la modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza rispetto a condizioni oggettive prima della guerra, chi ha scritto quell'articolo mai avrebbe immaginato che lo stesso potesse essere utilizzato un domani per una guerra al confine con l'Europa e in Europa. Credo che questo un tema su cui riflettere, che ha cambiato molto le priorità, insieme ad una serie di fattori di carattere internazionale, penso all'Inflation reduction act messo in campo dal governo americano e alla necessità di dare una risposta adeguata su questo fronte. Il Governo sta lavorando seriamente con spirito costruttivo in questa direzione. Mi auguro che, oltre a questo dibattito parlamentare, ne avremo degli altri e che l'approccio possa essere positivo e propositivo. Questo è ciò che noi vogliamo portare avanti e questo è il lavoro che faremo.

essendo qui oggi, dimostra attenzione nei confronti del Parlamento e di un Piano che, come ha dichiarato nella sua replica, è lo strumento fondamentale per la crescita della nostra Nazione. Con la mozione di maggioranza presentata oggi, sottoponiamo all'Esecutivo precise e puntuali richieste che ci arrivano, ad esempio, dai territori, quindi *in primis* dai Governatori regionali, dagli amministratori locali, dai cittadini, dalla società civile e dalle nostre imprese.

dipenderà lo sblocco della terza rata del PNRR, da 19 miliardi di euro. Com'è noto e lo dicono i fatti, questo Governo ha lavorato bene proprio per raggiungere questo obiettivo, che siamo sicuri arriverà nei tempi previsti e dovuti. Il centrodestra alle chiacchiere preferisce il linguaggio del fare. Sono i numeri a dircelo: l'Italia ha raggiunto 55 obiettivi entro il 31 dicembre 2022 per avere la terza rata. Il Governo, come ha ricordato anche lei prima, signor Ministro,

ad aver presentato alla Commissione tre richieste di pagamento. I numeri sono complessi: 527 scadenze da rispettare, un numero superiore a quello di altri Paesi (Spagna, Francia, Polonia e Grecia), che come noi beneficeranno di risorse simili in termini economici. C'è un dato però su cui vorrei porre l'attenzione. I costi stimati inizialmente dalla Commissione europea per il *recovery* erano agganciati a tassi di interesse più contenuti rispetto a quelli attuali, ma i tassi sono aumentati dopo i rialzi i rialzi decisi dalla BCE. Bruxelles aveva stimato un costo del denaro pari all'1,1 per cento per finanziare il *recovery*, mentre oggi è al 4 Non solo: è cambiato anche il quadro socioeconomico oltre a quello geopolitico, poiché sul fronte internazionale è scoppiato purtroppo il conflitto in Ucraina, con le ripercussioni che esso ha avuto su tutto il vecchio continente, Italia compresa. Sul fronte socioeconomico, la crisi energetica è stata come una miccia: ha fatto scoppiare l'ondata dell'inflazione, con un aumento generalizzato dei prezzi che ha colpito le fasce sociali più deboli della nostra popolazione e contro cui, non a caso, nella scorsa manovra abbiamo investito due terzi di tutta la legge di bilancio. I frutti di questi primi 250 giorni di Governo e di centrodestra alla guida di Italia si stanno vedendo: sia l'Istat che Bankitalia hanno rivisto al rialzo le stime di crescita del PIL: +1,3 per cento. È il segno che questo Governo sta lavorando bene e con concretezza. Ma, onorevoli colleghi, non siamo abituati a gioire, non ne abbiamo il tempo né la voglia. Sappiamo che le prospettive di crescita della nostra Nazione, come ci ha ricordato qualche giorno fa l'OCSE, dipenderanno dalla capacità del nostro Paese di mettere a terra le risorse europee del Next generation EU. Questo obiettivo sarà essenziale per una crescita duratura e concreta. Ecco perché oggi siamo qui. Siamo qui perché come maggioranza chiediamo, alla luce del nuovo quadro socio-economico, di tenere conto del nuovo contesto e quindi di condividere il percorso di revisione del Piano con il Parlamento, aggiornando lo stesso Piano con l'inserimento del capitolo del REPowerEU. Come noto, infatti, il Parlamento europeo e il Consiglio del 27 febbraio 2023 hanno approvato le modifiche al regolamento istitutivo del PNRR. Al momento solo otto Paesi su ventisei in Europa, tra cui l'Italia, hanno presentato una modifica al PNRR. Di questi otto Paesi, due non prevedono il REPowerEU, ma modifiche più semplici. Il 18 maggio è iniziato il confronto tra Governo e Commissione europea proprio su questo punto: parliamo di investimenti che aiutano imprese, famiglie e territori a far fronte, ad esempio, al caro energia. Sono convinto che il metodo messo a punto dal ministro Fitto sia quello giusto: è il linguaggio della concertazione, del dialogo e del confronto con i rappresentanti dei territori, a partire appunto dalle nostre Regioni e dai nostri governatori. Questo metodo lo condividiamo, perché il PNRR non è un obiettivo o una partita di destra o di sinistra, ma una sfida che appartiene a tutto il Paese e a tutta l'Italia. Non solo. Questo Governo ha fatto un'altra scelta, che noi condividiamo e accogliamo con favore: ha deciso di mettere insieme il PNRR con i fondi con i fondi delle politiche di coesione, per utilizzare al meglio le risorse europee e per salvaguardare l'organicità dei progetti previsti proprio dal PNRR. Si tratta di una scelta che è esattamente in linea con le raccomandazioni dell'Unione europea, che ha chiesto agli Stati membri di sviluppare un raccordo operativo tra le risorse ordinarie e quelle del PNRR. L'obiettivo è fare velocemente e bene. Questo è un obiettivo che tutti dovremmo avere a cuore. Entro il termine del 31 agosto verranno fatte le modifiche concordate preventivamente con la Commissione. È chiaro che il capitolo del REPowerEU all'interno del nuovo PNRR dovrà essere oggetto di un esame approfondito da parte del Parlamento, che è quindi centrale in questo passaggio. Non a caso - mi avvio alla conclusione - con la mozione condivisa da tutte le forze politiche della maggioranza di centrodestra abbiamo chiesto di elaborare una proposta di aggiornamento al piano europeo, che focalizzi l'attenzione su quei progetti su quelle misure che hanno registrato ritardi o un rilevante incremento dei costi a causa dell'inflazione. Oggi siamo qui in Aula per chiedere il massimo impegno affinché questo piano, che è il più grande piano di investimenti pubblici del nostro Paese degli ultimi decenni, dia le giuste risposte che servono a tutti gli attori coinvolti, puntando sul rafforzamento dell'autonomia energetica e sul sostegno delle attività produttive alle nostre imprese e alle nostre famiglie). Proprio per questo motivo, il Gruppo Civici d'Italia-UDC-Coraggio Italia-MAIE voterà convintamente a favore della mozione condivisa da tutta la maggioranza.

ribadire qui le ragioni per le quali io e il mio Gruppo riteniamo vitale per il nostro Paese raggiungere in tempo utile gli obiettivi fissati dal PNRR. Ce lo siamo detti tante volte. Prima la pandemia e poi ovviamente la crisi energetica conseguente al conflitto in Ucraina hanno determinato una situazione che conosciamo bene, di cui abbiamo spesso parlato e che naturalmente ci preoccupa moltissimo: l'aumento esponenziale delle disuguaglianze, il divario che è cresciuto, la condizione sociale di milioni di persone che è peggiorata in maniera profonda. Qui voglio soltanto citare i dati sulla sanità pubblica, che la dicono lunga sullo stato in cui versa il Paese

Le liste di attesa sono infinite. Ci sono ormai tantissimi casi di rinuncia alle cure. La diseguaglianza tra Nord e Sud - lo dico a lei, Ministro, che è un uomo del meridione - è aumentata ed è cresciuta senza precedenti. In Italia finanche l'aspettativa di vita delle persone cambia a seconda di dove si ha la fortuna di nascere; e cambia di alcuni anni, non semplicemente di dettagli. Il Servizio sanitario nazionale arretra, il privato avanza; ci sono diverse inchieste della stampa, anche recenti, a tale riguardo. Sappiamo bene però che la sanità pubblica, che è una conquista sociale dal nostro punto di vista irrinunciabile, ha profondamente a che fare con il livello di salute e di benessere della popolazione, ma anche con la crescita economica del Paese. C'è un nesso molto forte e studiato tra la condizione di crescita di un Paese e il livello di salute e di benessere dei suoi cittadini. Dentro questo quadro, già di per sé drammatico, aggiungiamo anche che negli ultimi dodici mesi più di quattro italiani su dieci non sono riusciti a risparmiare, schiacciati dal peso delle bollette, dell'inflazione e dei rincari,

delle società energetiche. Tutto questo lo dico semplicemente per capire qual è il contesto politico, economico e sociale all'interno del quale si cala la nostra discussione. Nel 2022 l'inflazione ha raggiunto il suo *record*

i famosi 190 miliardi messi a disposizione dal PNRR sono totalmente irrinunciabili. Vorrei dire che in una condizione come quella in cui siamo, difficile e complessa, ci si aspetterebbe dal Governo - da qualsiasi Governo - che davvero venissero messe in campo tutte le forze e tutte le energie per raggiungere tempestivamente gli obiettivi fino al 2026, anche perché a me preoccupa molto che in qualche modo possa essere reso vano il risultato politico che dal mio punto di vista fu assolutamente straordinario. Non fu infatti una cosa normale che il Governo Conte II, del quale noi avemmo la positiva possibilità di far parte, riuscisse a strappare quei fondi in Europa. Non era scontato che ci fosse quel tipo di chiave di lettura in quel momento; non era nemmeno scontato che il PNRR in qualche modo rompesse una lunga stagione europea, segnata invece dalle politiche dell'austerità. Penso che il Governo dell'epoca fece un eccellente lavoro su questo, soprattutto nella fase più difficile e più acuta

davvero con una certa incredulità a quello che sta accadendo in questi mesi; alle incertezze, alle titubanze, anche alle scelte sbagliate che ci sono state, che io penso possano davvero porre a rischio il raggiungimento degli obiettivi previsti per l'anno in corso e quindi, come è stato ricordato anche nella mozione che abbiamo presentato e nella discussione di oggi, il conseguimento della terza e della quarta rata spettante all'Italia per i complessivi 35 miliardi di euro. Francamente il fatto che si inizi già a parlare di possibili rinvii delle prossime scadenze mi lascia perlomeno perplesso. A certificare questi ritardi nell'attuazione degli obiettivi richiesti, come sappiamo - anche di questo abbiamo, nelle ultime ore, lungamente discusso - la Corte dei conti per aver esercitato il proprio ruolo di controllore è stata sanzionata con un provvedimento *ad hoc*

sono le sorti del Paese e della popolazione impoverita dalla crisi, da anni di politiche sbagliate. Le numerose criticità evidenziate lo scorso 28 marzo dalle sezioni unite unite in sede di controllo della Corte nella terza relazione semestrale sullo stato del PNRR impongono al Governo, ma in realtà a tutti noi, un vero e proprio cambio di rotta. Credo che in questo contesto sia indispensabile rafforzare la collaborazione e lo scambio di informazioni con la Commissione europea. È necessario e indispensabile che il Governo ponga in essere un dialogo molto più forte di quello che c'è stato finora con il Parlamento, innanzitutto garantendo informazioni e trasparenza, fornendo le relazioni, le schede di progetto che rendano chiare le prospettive del Piano. considererei invece particolarmente sbagliato un non sufficiente coinvolgimento del Parlamento né sulle modifiche che il Governo potrebbe apportare al PNRR, né tantomeno sull'inserimento di un apposito capitolo dedicato al Piano REPowerEU che lei stesso ha citato, adottato a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e che ha come obiettivo rendere l'Europa indipendente dai combustibili fossili russi prima del 2030. Chiedo con forza la collaborazione con la Commissione europea attraverso uno scambio costruttivo e continuo. Penso sia necessaria un'informazione efficace e completa che permetta di dare soluzione al ritardo nel pagamento della terza rata in tempi rapidi e utili. Credo che il Governo - come dicevo poc'anzi - debba mantenere sempre informato il Parlamento

in qualche modo abbia finalmente assunto una centralità e abbia convinto anche altre forze politiche della giustezza di questa argomentazione.

il Governo a fare del suo meglio per realizzarlo. Signor Ministro, è il sistema Paese che realizza il PNRR, non il Governo da solo, e del sistema Paese fanno parte anche il Parlamento con le opposizioni, nonché gli enti locali che poi materialmente realizzano i progetti. Devo dire in sincerità che, quando si prova a esprimere qualche critica a come viene portato avanti il PNRR, dalle risposte del Governo sembra che questo Piano sia una sorta di incombenza posta sul vostro tavolo Grazie a tutti

per aumentare la competitività del sistema produttivo e per sciogliere i ritardi e i nodi strutturali del Paese. Il problema, ministro, ha riguardato soprattutto la comunicazione: voi siete al Governo da ottobre prima avete detto che il PNRR non si toccava; poi che bisognava rinunciare a una parte dei fondi; poi che bisognava darli ai territori che li sanno spendere; poi che i fondi restavano ma il Piano andava rivisto. Questa, almeno, è l'impressione che se ne è avuta. Pertanto, vorremmo finalmente capire esattamente di cosa si tratta. Lei oggi è stato

parte del sistema Paese. Gli apparati dello Stato non sono qui per scaricare ad altri la colpa di ciò che non va, ma sono qui per fare sintesi e per coordinare il Paese a raggiungere gli obiettivi stesso modo è inaccettabile prendersela con la Corte dei conti e con quanti stanno evidenziando le difficoltà di far andare bene le cose. Questo è da evitare e, se traspare, è perché qualcuno lo dice.

dobbiamo sbloccare il più rapidamente possibile la terza e la quarta *tranche.* Ci vuole chiarezza col Parlamento e con il Paese sui termini della revisione del Piano e ciò - da un lato - aiuterebbe anche il confronto con l'Unione europea, ma - dall'altro lato - aiuterebbe a portare il confronto interno sul piano dei contenuti e non su quello delle chiacchiere. Il terzo punto riguarda i contenuti: se si deve mettere mano al piano, lo si faccia in un'ottica di rafforzamento delle politiche per la transizione ambientale, per la protezione del territorio e - come è stato detto quasi da tutti - di lotta al dissesto idrogeologico. Il PNRR, signor Ministro, appartiene a tutti gli italiani. Cambiate passo. Fate del Parlamento il luogo della discussione e del confronto. Create le condizioni affinché attorno a questa sfida possa costruirsi uno spirito di unità e di impegno condiviso. Un fallimento del PNRR non sarebbe solo vostro, ma sarebbe il fallimento di tutti noi. Pertanto dobbiamo portare a casa

Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, la nostra posizione sul PNRR è presto detta: per noi è la prima preoccupazione. Questo perché abbiamo la consapevolezza che dalla realizzazione e dalla messa a terra degli investimenti e dall'approvazione delle riforme collegate al PNRR non solo dipendono il superamento dei divari tra Nord e Sud, la crescita del Paese, la qualità della vita dei cittadini e la modernizzazione; ma anche perché, fra un consenso facile e la consapevolezza che le sfide ineludibili che il Paese ha davanti passano dal PNRR, noi scegliamo di affrontare, anche dai banchi dell'opposizione, queste sfide. Quali sono tali sfide? Il superamento dell'inverno demografico; la denatalità; affrontare in maniera seria e compatibile con il mantenimento delle filiere produttive i cambiamenti climatici, che ci sono; le transizioni, quella ecologica ma anche quella digitale. Insomma, sono tante le sfide ineludibili che passano dalla realizzazione del PNRR. Quindi, non sentirà mai il Terzo polo inveire contro il Governo e strumentalizzare il tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza per attaccare il Governo. Non è la nostra postura, non è il nostro modo di intendere il ruolo di opposizione.

dalla nostra capacità di affrontare la sfida del PNRR dipende anche una nuova visione d'Europa. E noi vogliamo essere, come Paese, molto ambiziosi, nel delineare un'Europa che deve essere non la sommatoria dei singoli nazionalismi, ma un'Europa capace di traguardare il futuro e di andare verso gli Stati Uniti d'Europa. *(Applausi)*. Fare questo significa avere la consapevolezza che il nostro debito è arrivato a 2.800 miliardi, che il rialzo dei tassi mette sempre più in difficoltà la nostra economia. Quindi, bisogna essere seri e responsabili, anche perché non possiamo restare indietro. Un grande Paese come gli Stati Uniti ha varato l'Inflation reduction act e, attraverso un *booster* che vale tre volte Next generation EU, prova a dare un sostegno forte a quella economia. Noi sappiamo bene che fallire la sfida del PNRR significherebbe lasciare i Paesi soli davanti ai rischi della globalizzazione. E di fronte alla sfida della competizione globale noi ci sentiamo rassicurati dal fatto che, invece, sia l'Europa a favorire le condizioni di una crescita, di una ricetta industriale, di una capacità di affrontare i temi economici. Pertanto, fra chi sceglie la piazza, addirittura evocando l'utilizzo del passamontagna, e chi ha chiaro cosa voglia dire riformismo ed europeismo, noi scegliamo questa seconda strada. Lo facciamo, però, senza fare sconti al Governo, Vengo, quindi, al tema della *governance*. Lei lo ha spiegato prima e noi, signor Ministro, le diamo atto di avere imboccato una strada. Avremmo preferito una continuità con il precedente Governo, e non per una questione di appartenenza o di partigianeria, ma perché forse si sarebbe perso meno tempo. Al tempo stesso, però, noi abbiamo ben chiaro che questo è un Governo politicamente legittimato dal consenso e che ha compiuto una scelta diversa. È una scelta che noi non osteggiamo, perché osteggiarla significherebbe da un lato - non fare l'interesse del Paese e - dall'altro - aiutarvi ad avere degli alibi, che noi non vogliamo darvi. Avete fatto la scelta di un cambio di *governance*? È assolutamente legittimo. Prendetevene le responsabilità fino in fondo e fate quello che avete promesso, ovvero mantenete le scadenze. Il problema, signor Ministro, non è la terza rata; probabilmente è la quarta. È lì che ci sarà un vero banco di prova rispetto a ciò che il Governo è in grado o non è in grado di fare. oggi l'atteggiamento del Terzo polo è di chi è consapevole che avevate tutte le facoltà di scegliere una diversa *governance*. Lo avete fatto. La cosa importante è che non si disperdano queste risorse, che si rispettino le scadenze. E, a riprova della nostra buona fede, sicuramente non possiamo essere annoverati fra coloro che hanno fatto polemiche attorno ai controlli concomitanti della Corte dei conti. Carlo Calenda, da un lato, e Matteo Renzi, dall'altro, sono stati molto chiari nel dire che non si può nemmeno eccedere con i controlli e concorrere in questo modo a rallentare il piano. I controlli vanno fatti, ma noi dobbiamo dimostrare, come Paese, e non solo voi come Governo, che siamo all'altezza della sfida, che rispettiamo le scadenze e che l'Italia, con la schiena dritta, si presenta in Europa con i compiti fatti. *(Applausi)*. Quello che le chiediamo è che ci sia un coinvolgimento importante del Parlamento e anche delle opposizioni. Su questo mi permetto di dire che anche il precedente Governo, che era di unità nazionale, ha dato spazio al Parlamento e ha provato a condividere una discussione fra maggioranza e opposizione. Le scadenze che avete davanti sono molto ravvicinate; si parla del 31 agosto, e quello che ci auguriamo è che tale scadenza sia il momento nel quale anche l'opposizione - magari un po' prima di Ferragosto ditecelo - sappia cosa intendete fare e quali sono le modifiche che intendete portare avanti per realizzare il PNRR. Pensiamo che sia importante coinvolgere il Parlamento e metterlo a conoscenza di quei cambiamenti, magari necessari, magari suggeriti anche dalle Regioni o dagli enti locali, che vanno assolutamente condivisi. Sicuramente non giochiamo, come ha detto anche prima la collega Paita, al gioco del tanto peggio, tanto meglio, ma vogliamo che le cose vengano fatte nel migliore dei modi. Abbiamo alcune preoccupazioni e abbiamo alcune ragioni che vogliamo esprimere all'interno di questa Assemblea. La prima preoccupazione riguarda la sanità, signor Siamo molto preoccupati, perché avete scelto di non ratificare il MES e quindi, a dicembre, avete perso un'opportunità, che secondo noi era quella di utilizzare quelle risorse. Avete fatto una scelta diversa quello che ci preoccupa è che la guerra - da un lato - e l'emergenza energetica - dall'altro lato - hanno distolto lo sguardo dalla causa scatenante di Next generation EU, che è l'esigenza di adeguare il sistema sanitario nazionale non solo al tema delle pandemie, ma banalmente a far fronte all'invecchiamento della popolazione. Su questo il PNRR non basta, perché possiamo ragionare delle case di comunità, possiamo cambiare quell'impostazione, ma alla fine, signor Ministro, mancano gli infermieri, mancano i medici e c'è un problema gigantesco di liste d'attesa Non è che ve la cavate con il PNRR, perché purtroppo quei problemi necessitano di un investimento maggiore, che va trovato. Accanto a questo abbiamo avanzato due proposte ed è la ragione di una riscrittura della nostra mozione. Sono due proposte che avevamo già presentato anche precedentemente. La prima riguarda ItaliaSicura, ovvero la necessità di un'unica unità di missione per affrontare il dissesto idrogeologico. È una proposta di buonsenso, contro la burocrazia, che viene dal basso e che ci auguriamo voi possiate accogliere. Al tempo stesso, c'è una richiesta forte che Carlo Calenda porta avanti da tempo, e noi con lui, che è quella del ripristino di Industria 4.0 *(Applausi)*. Ci auguriamo che una delle misure con cui reimpiegare i fondi del PNRR non spesi possa essere Industria 4.0. Lo diciamo perché siamo favorevoli alla transizione ecologica, perché vogliamo assolutamente che l'Italia imbocchi la via della transizione. Ma, al tempo stesso, abbiamo ben chiaro che la tutela delle nostre filiere produttive e dei nostri posti di lavoro passa anche dalla difesa degli interessi nazionali. Le nostre imprese hanno bisogno di Industria 4.0, hanno bisogno di alcuni correttivi in Europa rispetto alla posizione di Timmermans, che non corrisponde agli interessi delle imprese italiane. Su questo, ci auguriamo che il presidente Meloni faccia sentire la propria voce, ma porti a casa dei risultati. La transizione ecologica deve essere compatibile con la difesa dei ceti produttivi, con la difesa delle nostre filiere, in particolare quella dell'auto, e con la difesa degli interessi nazionali. Chiudo dicendo che il compito della politica non è solo quello di rallegrarsi dei risultati raggiunti. Il primo trimestre 2023 - è vero - ha fatto segnare all'Italia una crescita superiore alle attese. Voi avete provato ad intestarvi questa crescita, ma vi ricordo che è il frutto del lavoro nel settore del turismo e dei servizi e anche dei molti incentivi che sono stati dati all'edilizia. Quello che resta però è che il settore della manifattura e dell'impresa ha delle criticità e rispetto ad esse mi auguro che la riscrittura del PNRR vada ad intercettare le esigenze. Noi preferiamo questo modo di fare opposizione, perché non possiamo permetterci il lusso di sprecare la straordinaria occasione del PNRR, un Piano che riguarda non una forza politica o un Governo, ma il Paese. Ecco perché non smetteremo di incalzarvi, di pretendere il rispetto delle scadenze, di invocare la collaborazione e di entrare nel merito. Questa è la ragione per cui chiediamo che la votazione delle mozioni, proprio perché sia fatta sulla base non delle bandiere ma dei contenuti, venga effettuata per parti separate.

I Piani nazionali di ripresa e resilienza sono la conseguenza di una crisi economica causata da una novità assoluta per il panorama internazionale: la pandemia da Covid-19. Le conseguenze della stessa e il modo in cui la si è affrontata a livello mondiale sono state una diminuzione della crescita economica e del benessere in tutto il mondo, Europa compresa. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza italiano è stato approvato dall'Unione europea a metà del 2021, con la previsione di una cadenza di attuazione degli interventi che arriva a metà del 2026. Il Governo Meloni, che si è insediato nel novembre del 2022, oltre due anni dopo, ha dovuto quindi prendere atto di quanto si era fatto e di quanto si è dovuto realizzare. In questo va ricordato che il PNRR italiano prevede 132 programmi di investimenti e 63 riforme, che vengono adottate oggi e che saranno strutturali. Le risorse - lo sappiamo - sono tante: 222 miliardi complessivi, ai quali si aggiungono i quasi 31 miliardi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. È evidente quindi che le risorse vanno spese molto bene, ottimizzando il risultato. Va ricordato che, quando si è insediato il Governo Meloni, erano stati centrati 25 dei 55 obiettivi da raggiungere entro la fine dell'anno del 2022; gli altri 30 li ha ottenuti questo Governo. Va evidenziato che ora l'incasso delle rate successive alla terza è legato soprattutto alle fasi di attuazioni concrete degli investimenti che sono stati programmati e all'entrata a regime delle riforme approvate. Ecco perché è necessario un monitoraggio attento e soprattutto l'adozione di atti, azioni e soluzioni che portino alla piena realizzazione di quanto proposto, che rispettino le scadenze previste. Per queste ragioni a gennaio è stata adottata una riorganizzazione della *governance* del PNRR, rafforzando il sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio. Allo stesso tempo, sono state rafforzate la risposta degli enti interessati al Piano e la loro capacità amministrativa, così come sono state semplificate le procedure, con lo scopo principale di rispettare i tempi di realizzazione degli investimenti. Il passaggio dalla *governance* iniziale, prevista a maggio del 2021, al nuovo modello disegnato a gennaio del 2023, non ha implicato rallentamenti, in quanto si sono rafforzate le strutture iniziali e si è reso più coerente e razionale il coordinamento. Nel frattempo, si è purtroppo verificato un altro evento ancora più eccezionale, il conflitto in Ucraina, che ha avuto un impatto enorme sul costo dell'energia, dei materiali da costruzione e delle materie prime, e ha modificato l'impatto delle importazioni e delle esportazioni a livello mondiale. La crisi economica che ha colpito l'Europa ne è l'evidente conseguenza. Il lievitare dell'inflazione ha inciso e incide anche su molti progetti *in itinere* legati al piano italiano. Per questo il Governo Meloni, attraverso il ministro Fitto, ha messo in moto una serie di verifiche tra attività programmate in precedenza e la loro effettiva realizzabilità. Si aggiunge a questo che l'Europa ha inserito a febbraio di quest'anno il capitolo REPowerEU proprio per affrontare il tema della resilienza e dell'indipendenza energetica dell'Unione europea, oltre che della sostenibilità delle fonti. A questo capitolo viene collegata la possibilità di utilizzare anche la parte di fondi di programmazione europea 2014-2020 a sostegno delle piccole e medie imprese e delle famiglie bisognose. Di fronte a questi nuovi fatti concreti il Governo Meloni ha approvato la terza relazione al Parlamento sul PNRR, in cui vengono ridefiniti e rimodulati alcuni termini e scadenze. La mozione di maggioranza prende atto dei fatti oggettivi e impegna il Governo a proseguire nell'azione già intrapresa, che può comprendere anche le necessarie variazioni ai termini del Piano, al fine della sua completa e piena attuazione. Lo scopo è quello di utilizzare al meglio le risorse, che sono importanti, che vanno investite con oculatezza e serietà, accompagnando la crescita economica italiana e la modernizzazione del Paese attraverso l'articolata attuazione delle riforme programmate. Per noi di Forza Italia è stata una settimana terribile, ma, nonostante le varie Cassandre che si sono susseguite, noi siamo uniti e compatti. Noi di Forza Italia a testa alta continueremo a sostenere il Governo di centrodestra, quel centrodestra inventato, creato e voluto dal nostro Silvio Berlusconi, così come abbiamo fatto ieri e faremo domani. Noi di Forza Italia continueremo il percorso tracciato dal presidente Berlusconi, con i piedi ben piantati nella storia di questi ventinove anni e lo sguardo rivolto al futuro.

dalla conferma della disponibilità del MoVimento 5 Stelle a contribuire affinché il Governo porti a compimento, durante il suo mandato, il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Questa disponibilità è stata

emergerà anche dal mio intervento, nel quale vi posso assicurare che non parlerò di Corte dei conti, di danno erariale o di interventi divisivi o che possano in qualche modo essere di solletico ad alcune parti politiche, ma che credo non rilevino rispetto all'impianto complessivo del Piano. Con questo approccio, però, ribadisco un altro elemento. Io ritengo che su alcuni temi, in particolare quando il Presidente del Consiglio del nostro Paese partecipa a consessi europei, si tratta del Presidente del Consiglio italiano e quindi avere il massimo supporto delle forze politiche, a tutela degli interessi nazionali del nostro Paese in Europa. Questo, signor Ministro, è stato ribadito anche da lei nel suo intervento e per noi vale,

rispetto al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla necessità che l'Europa facesse qualcosa che non aveva mai fatto prima, ossia intervenisse con un debito comune in aiuto dei propri Paesi membri e si comportasse veramente per la prima volta, non mi sembra che chi in quella fase era all'opposizione del Governo Conte abbia supportato il nostro Paese nella tutela degli interessi nazionali.

per dire la verità molto limitati - non contribuiscono al modo con cui noi approcciamo il tema del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Si è detto che 25 obiettivi sono stati raggiunti dal Governo precedente e 30 dal Governo Meloni, ma faccio l'esempio del bando agrisolare:

fatto detto esempio e lo citerò più volte, anche per capire quali sono le modalità con cui si vuol modificare il Piano. In realtà il centro vero della discussione di oggi, al di là delle mozioni delle forze di opposizione, era stimolare un dibattito rispetto al come si vuole intervenire sul Piano, e non sul se. Su questo, però, vedo ancora che non c'è molto. molto. Oggi mi aspettavo una mozione di maggioranza che impegnasse il Governo, nelle modifiche necessarie al Piano, ad avere dei paletti, dei recinti e un perimetro chiaro sul come ci si muove anche sulle singole missioni e sui singoli interventi. È questo che ancora non abbiamo capito, al di là del fatto che la maggioranza e il Governo

dichiarato sul PNRR: la frittata ormai è fatta, sono soldi che non bisognava prendere. Non mi sembra che questo sia l'approccio di tutto il Governo e di tutta la maggioranza. Questa confusione nel dibattito non l'abbiamo

giugno 2023, dicembre 2023 o giugno 2024, e quindi tara nuovamente il *target* per non cambiare l'obiettivo finale. Va benissimo, ma è solo questo ciò che si proporrà? Una rifasatura temporale delle missioni, dei singoli obiettivi e dei singoli *target* del Piano? Parliamone. Si stralciano alcune parti di Piano? Quando sento autorevoli esponenti del Governo dire che nel Piano bisogna dare i soldi alle partecipate di Stato, chiedo: in che modo? Per fare cosa?

Senza alcun tipo di volontà di rivangare dibattiti rispetto alle cessioni, al superbonus e quant'altro - non è questa la sede e non voglio farlo che quello della cessione del credito sia uno strumento fondamentale di sostegno agli investimenti privati per mobilitare il capitale privato delle imprese è una realtà oggettiva. Vogliamo discutere quindi se, attraverso una rimodulazione del Piano, possiamo incrementare quella parte di crediti di imposta e di cessione di crediti che stimolano gli investimenti privati dormienti nelle imprese italiane? facessimo un accenno a questo dibattito, a questa discussione, un po' più nel merito delle cose che vogliamo chiedere all'Europa. Vogliamo chiedere il REPowerEU? Benissimo: come? Altro tema: terza raccomandazione della Commissione rispetto alla compenetrazione di utilizzo di fondi e di risorse diverse per i vari strumenti di sostegno che ci sono. Mi riferisco ovviamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con all'interno anche la parte del Piano nazionale complementare, e ai fondi strutturali FSC. Il principio di quella raccomandazione è sempre stato di non duplicare gli interventi,

le finalità dei fondi strutturali FSC vengano stravolte dall'utilizzo di quelle risorse rispetto alle necessità del nuovo Piano di ripresa e resilienza modificato, senza conseguire gli obiettivi fissati con i fondi strutturali FSC. Se oggi c'è un problema di capacità di spesa - come è stato più volte evidenziato quali sono gli strumenti e qual è la strada per potenziare quella capacità di spesa? Non mi piace il ragionamento secondo il quale, siccome non c'è capacità di spesa, non vengono dati i soldi. Siccome non c'è capacità di spesa, ti aiuto ad averla. Questo deve essere l'obiettivo con cui si affronta il tema. quindi questo momento di confronto e siamo disponibili a farlo in qualsiasi sede e in qualsiasi forma Ci sono le mozioni sul tavolo. Annuncio ovviamente il voto favorevole alla mozione del Partito Democratico, del MoVimento 5 Stelle, dell'Alleanza Verdi e Sinistra e delle altre forze di opposizione.

mozione della collega Paita, perché nello stesso punto vengono messi assieme la riformulazione della struttura di missione ItaliaSicura e il 4.0. Ovviamente siamo totalmente a favore di un potenziamento di Transizione 4.0, ma non tornerei a Industria 4.0. 4.0. Industria 4.0 prevedeva piani di ammortamento che tagliavano fuori totalmente il comparto agricolo e tutte le imprese italiane che non fanno il bilancio, che sono sempre di più. Io tornerei a rafforzare Transizione 4.0, cioè un sistema di credito d'imposta che ha funzionato tantissimo e su cui abbiamo messo 24 miliardi. Continuare a dire di voler rifare Industria 4.0 con gli strumenti dell'ammortamento credo sia profondamente riduttivo del modo in cui andiamo a incidere sui sistemi produttivi italiani in fatto di micro imprese, che molto spesso hanno dei sistemi forfettari, non fanno bilanci e non fanno ammortamento. anche sulla mozione della collega Paita chiediamo un voto per parti separate.

l'impressione che abbiamo nell'affrontare questa dichiarazione di voto sulle mozioni che sono sul tavolo è che la discussione sul PNRR venga portata all'attenzione dell'opinione pubblica da una parte dell'opposizione - non da tutta l'opposizione - soprattutto per cercare di fare polemica e attaccare il Governo e non invece con quella critica costruttiva che meriterebbe un Piano così importante (a detta di tutti). Alla fine si vede, nel dibattito politico quotidiano, che tutte le volte che si parla di PNRR ci sono sempre lo scontro e la polemica, L'ultima di queste polemiche è stata la questione legata ai famosi controlli concomitanti della Corte dei conti.

inserendo di fatto un passaggio ulteriore. È un po' una contraddizione; vogliamo accelerare, ma nello stesso tempo introduciamo un passaggio in più sapendo come funziona

successivo, come si evince dall'articolo 103, comma 2, della nostra Costituzione. Si parla di controllo di legittimità, fatte salve le competenze del giudice penale. Quindi il controllo di legittimità successivo è una cosa, i controlli di legalità sono un'altra. Chi è parlamentare questa differenza dovrebbe un minimo conoscerla; Tenuto conto poi che, a detta di alcuni costituzionalisti (qualcuno è stato anche Presidente della Consulta, come Sabino Cassese), sostanzialmente i controlli preventivi e concomitanti spesso sono inefficaci e servono a soddisfare il desiderio dei controllori di aumentare la propria sfera di influenza, come accade purtroppo spesso. Con ciò massimo rispetto del lavoro che fa la Corte dei conti, anzi l'invito al Governo - mi sembra che sia questo l'intento - è quello di lavorare

l'Italia cresce maggiormente rispetto a tutta l'eurozona e quando c'è stata l'emissione dei BTP Italia c'è stato un successo straordinario che testimonia che l'affidabilità e la credibilità a livello internazionale l'Italia ce l'ha *(Applausi)*, nonostante tutti i gufi e tutti gli scenari catastrofici auspicati già dai tempi della campagna elettorale. Polemiche incentrate anche sul fatto che dobbiamo essere più trasparenti, che ci vuole un maggiore coinvolgimento, che si vuole avere l'aggiornamento del Piano nei dettagli. Ecco, intanto mettiamo in evidenza il fatto che in questo momento il Governo ha aperto e sta

ci potrebbe essere un'oggettiva difficoltà nel realizzare determinati nostri intenti o desideri. Sinceramente, poi, tutta questa trasparenza, tutto questo coinvolgimento a noi sarebbe piaciuto vederli anche quando ha avuto origine il Piano di ripresa e resilienza nel nostro Paese, non solo adesso. Ricordo, infatti, che quando fu redatto

ci furono parecchie interlocuzioni, anche tra i partiti che sostenevano l'allora maggioranza, e tutti si lamentavano del fatto che tutte queste modifiche sostanzialmente non venivano portate all'attenzione del Parlamento, che di sei decreti ne votò cinque con la fiducia. fiducia. Capisco che sono dei nervi scoperti, ma anche rappresentanti del PD si lamentavano ai tempi del fatto che non c'erano queste verifiche puntuali che noi volevamo. Quindi, tutta questa trasparenza e questo coinvolgimento che noi reputiamo necessari e che sono scritti nella mozione di maggioranza, che certifica il fatto che il che il Governo relazionerà al Parlamento su tutti i cambiamenti necessari, avremmo voluto vederli anche allora, quando a comandare erano altri. *(Commenti).* La maggioranza relativa di quel Governo era giallorossa, me lo ricordo bene, non venite adesso a dire cose che non sono vere, anzi

nella sola Regione Lombardia, solo 2,1 miliardi sono gestiti dalla Regione, per il resto sono gestiti direttamente a livello centrale e questo è stato un errore madornale compiuto all'epoca, perché se si fanno piani centralisti,

Grazie a tutti

naturalmente tenuto conto che ci sono stati degli aspetti che sono cambiati come l'aumento dei costi, la scarsità dei materiali, alcuni investimenti percepiti come poco attrattivi e le difficoltà normative, amministrative e gestionali.

PNRR e sa benissimo che anche con un Governo diverso le difficoltà le avremmo incontrate. I tempi, le scadenze, le *milestone,* i *target* sono una battaglia di ogni giorno,

alla pandemia, ma per affrontare i nodi di fondo della competitività del nostro Paese rispetto ad altre aree territoriali. In parte avete anche riconosciuto questo, atteso che lo scrivete nel Documento di economia e finanza e in altri documenti importanti per

molto minore e l'Italia ci guadagna anche mettendo in campo delle procedure per portare avanti opere già in essere. Questo è quindi un passo in avanti che giudichiamo positivamente. La nostra impressione è che si sia perso tempo, perché voi stessi in campagna elettorale avevate insistito pesantemente sull'idea di modificare in radice il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ci saremmo quindi aspettati che voi vi poneste subito in queste Aule, in un pieno coinvolgimento con le Commissioni competenti, a discutere di quali progetti modificare; invece abbiamo assistito per mesi a una discussione sulla *governance,* su chi dovesse gestire e coordinare i progetti, se fosse meglio spostarla dal Ministero dell'economia e finanze alla Presidenza del Consiglio, se bisognasse spostare una parte delle risorse dai progetti del PNRR a quelli finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione. Così sono passati mesi.

settimane avete promesso un conflitto istituzionale fra Governo e Corte dei conti di cui nessuno avvertiva il bisogno, perché invece dovevamo concentrarci sui progetti da portare avanti e sulle modifiche da fare al Piano di ripresa e resilienza e questo non è stato fatto. Abbiamo perso tempo ulteriore e siamo arrivati alla fine, alla fine, all'ultimo momento, quando, il 31 agosto, magari con una serie di uffici chiusi, dovremo presentare, con il tempo che scade,

Perché si è aspettata la seconda metà di maggio, visto che dalla campagna elettorale dite di volerci spiegare e raccontare quali progetti verranno cambiati? Perché avete chiesto ai Ministeri solo a metà maggio, dopo che,

aperto un tavolo di confronto con i principali soggetti delle aziende partecipate dello Stato, Eni, Enel e Snam, per avere proposte di progetti? È vero non è vero che da tempo ve li hanno fatti avere? Perché non si è aperto formalmente un confronto con la Commissione, in cui discutere dei progetti per contrastare la povertà energetica, per spingere sulle energie rinnovabili, per promuovere a pieno l'attuazione e la possibilità di fare comunità energetiche su tutto il territorio nazionale? A queste domande ancora non ci avete risposto.

In qualche modo si dà l'idea che il sistema Italia non è in grado di affrontare fino in fondo la sfida del PNRR. Sappiamo che è una sfida complessa. Non ci nascondiamo i problemi. Parliamo il linguaggio della verità, come lei ha detto.

ne prendiamo atto e spostiamo una parte dei progetti, che sono finanziati con le risorse del PNRR, e li spostiamo sul fondo di sviluppo e coesione, su cui le Regioni hanno già altre idee e hanno già avviato un confronto un confronto con voi. Quei soldi, intanto, rimangono bloccati, quando invece, signor Ministro, li potrebbe

Noi abbiamo posto un obiettivo, molto chiaro, del 40 per cento di spesa al Sud. Se spostiamo una serie di progetti, che sono destinati al Sud, a valere sul fondo di sviluppo e coesione, saremo ancora in grado di rispettare quegli obiettivi? Oppure, alla fine, le risorse per il Sud diminuiranno? Su questo ancora non ci avete risposto. E noi vogliamo risposte chiare, perché lo meritano le comunità locali e le Regioni del Sud. Di grazia, poi, è possibile finalmente sapere di quanti miliardi stiamo parlando? Stiamo parlando di poche centinaia di migliaia di euro o di miliardi importanti, che noi spostiamo, ad esempio, dalla transizione ecologica per progetti che riguardano il Sud, sulle energie rinnovabili e su come noi accompagniamo questa difficile transizione? Sono investimenti? È il pezzo sulla rete ferroviaria? Non siamo in grado di tempo quelle opere attese da tempo? Magari facciamo partire il Ponte sullo Stretto, ma non siamo in grado di portare avanti progetti importanti per quelle comunità, sulla rete infrastrutturale o su quelle infrastrutture attese da tempo da quelle comunità. Su questo voi dovete darci delle risposte chiare. Noi non sappiamo di quanti miliardi si parli, di quali infrastrutture, di quali progetti e questo Parlamento merita di saperlo. Rinfreschiamo un po' la memoria anche al era in maggioranza nella passata legislatura. Vorrei leggere ciò che noi abbiamo chiesto insieme, perché c'era la sua firma, insieme a quella dei senatori Licheri, Bernini, Malpezzi, De Petris, Faraone e Unterberger. Si chiedeva, e l'abbiamo chiesto per tempo, di assicurare il pieno coinvolgimento del Parlamento, nonché la leale collaborazione con le Regioni e gli enti locali nelle fasi successive del PNRR, puntuale della necessaria documentazione relativa al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi intermedi contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, in modo da consentire al Parlamento di monitorare l'attuazione e l'impatto dei singoli interventi, il rispetto dei tempi

Da questo punto di vista, penso che noi dobbiamo mettere in campo una vera sessione in cui discutiamo di questo. Glielo dico perché

e il Governo del nostro stesso colore, abbiamo inchiodato il Governo precedente a venire qui, con la Commissione politiche dell'unione europea e con la Commissione bilancio, a discutere dei singoli progetti, delle missioni, in maniera dettagliata. Voi questo non l'avete mai fatto! *(Applausi)*. Di questo vi chiediamo conto e su questo vogliamo delle risposte precise. È questo il motivo per cui abbiamo presentato questa mozione. Voteremo chiaramente a favore della mozione presentata insieme dalle opposizioni, voteremo la proposta del Terzo polo, a cui chiediamo, per la prossima volta, se c'è la possibilità di fare delle battaglie insieme, di provare a farlo e di non distinguerci sul niente.

grazie per la presenza e l'ascolto costanti, non solo nei confronti di noi parlamentari, ma anche degli enti intermedi e dell'Unione europea. Grazie perché ci rende orgogliosi tutti, noi del Gruppo Fratelli d'Italia e la maggioranza. il suo tramite ringrazio anche la minoranza: sono per noi motivo di studio, ci insegnano sempre un metodo,

metodo? Ho dei dubbi e dopo questa giornata di interventi sul PNRR, i dubbi crescono. Andiamo per ordine, andiamo a fare chiarezza: è utile parlare di ieri,

Preciso che si tratta di prestiti sostitutivi e prestiti aggiuntivi. I prestiti sostitutivi sostituiscono coperture già disposte a legislazione vigente e gli aggiuntivi non sono dotati di autonoma copertura finanziaria. europea - finanzia progetti in essere, cioè progetti che già esistevano nelle pubbliche amministrazioni prima del 2019, del 2020, prima del PNRR, e di nuova progettazione. Questo lo avete voluto voi.

questa sigla, composta dalle iniziali di una frase in inglese, chiede di "non arrecare danno significativo". Occorreva cioè impostare tutti i progetti di investimento nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità. È il principio fondamentale su cui si dovrebbero basare il PNRR e tutte le sue rendicontazioni. È giusto, anzi giustissimo, ma è di difficile attuazione, non solo per la progettazione nuova, ma soprattutto per i progetti esistenti che avete scelto di inserire all'interno del PNRR, perché sono progetti che gli enti locali hanno progettato, ideato, pensato e messo a punto prima del 2019. Questa scelta, come tutte le altre sul PNRR, l'avete fatta voi, spero in maniera consapevole. Faccio due esempi di scelte consapevoli, a proposito dell'efficientamento energetico degli edifici scolastici e del dissesto idrogeologico. Nella maggior parte delle misure, su queste due voci,

grazie a voi, non sarà possibile. Ciò emergerà in maniera chiara dalle rendicontazioni.

Ormai il nostro tempo scorre a semestri. Il Governo Meloni si è insediato il 23 ottobre del 2022; il terzo semestre scadeva il 31 dicembre e il Governo Meloni Meloni ha inviato il tutto il 30 dicembre 2022. Come qualche collega ha detto, mi pare il collega Spagnolli, non vogliamo certo prenderci il merito della bravura di chi ci ha preceduto nel farci trovare 55 progetti e obiettivi realizzati. Assolutamente non vogliamo prenderci il merito del lavoro fatto dagli altri, ma neanche i controlli dell'Unione europea proprio sui 55 obiettivi del PNRR per cui l'Unione europea sta tardando a darci i soldi. Il 31 dicembre 2022 erano 30 gli obiettivi pronti, 55 quelli da raggiungere. A ottobre solo 25 pronti e lo voglio ricordare, perché da parte dell'Esecutivo Meloni nei primi due mesi c'è stato un lavoro incessante e, per

nel bene e nel male. Venendo alla quarta rata, 27 scadenze, di cui 7 obiettivi e 20 traguardi: 16 miliardi di euro. Dalla terza rata le rendicontazioni cambiano, sono più complesse; i *target* e le riforme richieste sono molto più articolati: sono scelte fatte da voi e la fase più delicata dell'attuazione è quella della realizzazione delle progettazioni e gli errori commessi nella redazione del PNRR si vedono tutti e sfortunatamente si vedono ora. Lo scenario economico mondiale cambia in maniera radicale. Gli enti intermedi hanno avuto difficoltà con la progettazione e ora ne hanno in fase di realizzazione per ciò che ho detto prima e per ciò che voi non avete fatto, per esempio, modificare e aiutare sulla mancanza di personale. Ben vengano i controlli, se questi se questi porteranno i nodi al pettine e tutti assieme potremmo risolvere il problema, se vogliamo. Il PNRR può essere cambiato e va fatto a beneficio dell'Italia, non contro il Paese: ben vengano, quindi, modifiche della *governance*, introdotta con il decreto- legge n. 13 del 2023, verifica della corrispondenza tra cronoprogrammi previsti e cronoprogrammi aggiornati. Ottimo è l'inserimento nel PNRR di un capitolo dedicato al REPowerEU, così come ottimo è l'utilizzo del REPowerEU per le piccole e medie imprese e le famiglie in difficoltà per le spese energetiche. La storia, però, va ricordata.

Occorreva evitare di avere fretta e di sbagliare per non ritrovarci al punto in cui ci ritroviamo, cioè dover mettere delle pezze. L'importante per alcuni, però, era prendere dei soldi, anche se questo avveniva presentando

ringraziando di nuovo il ministro Fitto per la grande opera di coinvolgimento che ha realizzato in questi otto mesi su tutti i livelli. Quante volte hai riferito tu, nessuno mai: si potrebbe scrivere una canzone, signor Ministro. Annuncio il nostro voto favorevole alla mozione Prima di passare alla votazione, avverto che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione. Vorrei richiamare l'attenzione in particolare dei Capigruppo, perché le richieste di votazione per parti separate, benché avanzate da un Gruppo per una mozione di un altro Gruppo, sono i presentatori

1 a 10. Sulla mozione che segue, della senatrice Paita, il Governo ha espresso parere favorevole

una richiesta di votazione per parti separate relativa al punto 2 del dispositivo, auspicata sia dal senatore Alfieri, sia dal senatore Patuanelli. Siamo riusciti a districarci in questo ginepraio.

Signor Presidente, intervengo a fine seduta per segnalare il fatto molto increscioso, direi scandaloso, che si sta verificando a Padova, dove la procura della Repubblica ha deciso di impugnare 33 atti di nascita di 33 bambini padovani, che erano stati registrati all'anagrafe come figli delle proprie famiglie. È un gesto che io non riesco a definire, per quanto risulti inumano, impietoso, gelido, distaccato e fondamentalmente contrario al senso di civiltà che ispira la nostra Carta costituzionale. *(Applausi)*. Il fatto che l'autorità giudiziaria entri nelle case di 33 famiglie per affermare che esse non sono tali è una cosa che ripugna al buon senso dei cittadini di un Paese civile. Signor Presidente, io le voglio ricordare che, quando i nostri Costituenti definirono la famiglia società naturale, lo dissero per spiegare che non può essere il legislatore o un giudice a stabilire cosa sia una famiglia. Una famiglia è ciò che è in natura, quello che si forma sulla base del progetto di vita delle persone. E se i Costituenti lo decisero, è perché nel regime precedente il legislatore decideva per esempio che un uomo cosiddetto ariano non poteva sposare una donna cosiddetta ebrea o viceversa e non volevano più che fosse la legge a stabilire cosa fosse una famiglia, ma che essa nascesse dall'amore, dalla volontà e dal progetto di vita delle persone. Qui ci sono 33 bambini a cui viene detto che devono cambiare cognome, a cui viene detto che la donna che chiamano mamma,

come legislatori, vi chiedo se sia tollerabile che questo Paese, nell'Europa occidentale di questo secolo, si possa permettere di violare la vita, il futuro, la stabilità, la sicurezza di 33 bambini e non avere ripugnanza di se stesso nel momento in cui lo fa. *(Applausi)*. Signor Presidente, mi scusi se stavamo discutendo animatamente, come si è visto. Intervengo per sollecitare la risposta a diversi atti di sindacato ispettivo, avendo presentato interrogazioni a risposta verbale

la quantità gigantesca di interrogazioni alle quali mi sono trovata a rispondere in rappresentanza e in sostituzione del ministro Speranza, anche durante l'epidemia da Covid, e non voglio scendere in polemiche in questa sede. La prego di rappresentare però la necessità, anche per rispetto dell'opposizione e diciamo della dinamica... Se lei, Presidente, ascoltasse sarebbe anche un bene. Potete forse parlare tra cinque minuti perché il mio intervento non durerà alcune ore. Rinviate un attimo il vostro confronto perché è questa una questione di rispetto anche dei diritti della democrazia e dell'opposizione. Credo che non si possa non aver avuto risposta a interrogazioni che sono ormai di quasi un anno fa o comunque dell'inizio della legislatura. La prego, Presidente, di volersi fare anche lei parte attiva affinché arrivi qualche segnale di vita da parte degli interrogati.

I viticoltori sono in allerta anche perché vedono andare in fumo un lavoro di un anno. Questo significa dover fare di tutto per riuscire a superare una grave criticità, soprattutto perché i trattamenti, che sono anche molto costosi, vanno fatti comunque anche se l'uva ormai è persa almeno per l'80 per cento, in alcuni casi. Quegli agricoltori, che devono sopportare il danno della perdita del guadagno derivato dal lavoro di un anno, devono anche sopportare queste spese.

Nella mia interrogazione pongo l'*alert* in modo che si possa

lavoro venga abbandonato. La Regione si deve esprimere per quanto riguarda la declaratoria delle eccezionali avversità atmosferiche e da lì il Governo deve assolutamente abbracciare questa istanza necessaria attivando anche tutto quello che è necessario, anche un altro fondo di solidarietà, e aiuti quali la sospensione di imposte, tasse e mutui per poter agevolare la sussistenza di quelle aziende. Potenziare studi e ricerche

Presidente, è con un po' di commozione, ma anche con grande orgoglio che in questi pochi attimi a disposizione ricordo l'amico senatore Stefano Bertacco.

con lo spirito di un guerriero e come uno che amava la vita. Credo che mai come in questa circostanza anche di combinazioni poc'anzi abbiamo ricordato il grande Silvio Berlusconi. In un modo diverso, il senatore Stefano Bertacco ha vissuto le cosiddette luci della ribalta, Limelight, per citare un famoso film

storie personali l'hanno messo duramente alla prova. Pensate che poco dopo la sua dipartita anche l'amato fratello Gigi lo lasciò

proprio per la sua dedizione nell'aiutare gli altri. Credo che questo sia un esempio per tutti noi, per chi fa politica. Quando una persona aveva bisogno,

in maniera clamorosa anche Fratelli d'Italia ebbe i suoi rappresentanti in Senato. Non mancava mai occasione di sentirci in questo percorso con Stefano. Era una persona molto concreta,

concluderei con una frase dello stesso quando dice che nulla finisce, cambia soltanto. Stefano è sempre qui con noi e vorrei ringraziarlo a nome di tutto il Gruppo. La Presidenza si associa al ricordo del senatore Bertacco. L'ho conosciuto e stimato. Pertanto, ringrazio il senatore Amidei per le parole che hanno interpretato un sentimento diffuso e doveroso.